Signor Presidente, purtroppo devo informarla e, con lei, devo informare l'Assemblea, che la Commissione che presiedo non è stata nelle condizioni di terminare l'esame del provvedimento. Anzi, se mi consente, vorrei sottolineare che non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di iniziare l'esame del provvedimento, visti i tempi ristrettissimi a nostra disposizione. A nome di tutta la Commissione, mi corre l'obbligo di auspicare che in futuro non si ripeta di nuovo questa situazione, che non mette la Commissione, e quindi il Parlamento, nelle condizioni di svolgere appieno il proprio ruolo e la propria funzione, per la quale abbiamo il mandato popolare. finestra"). La Presidenza condivide il suo auspicio e l'invito al Governo, affinché le Commissioni possano lavorare sempre meglio e con i tempi necessari. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 774, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

costruttiva, tenendo sempre una linea di confronto con il Governo. Quindi, ancora una volta, oggi appare davvero umiliante doversi confrontare con un testo che non abbiamo potuto esaminare in alcun modo. Ci viene chiesto l'ennesimo voto

proprio perché non ha alcun profilo di omogeneità, visto che dentro c'è di tutto (come dirò tra poco), è in palese contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. E, ancora di più, io chiedo al Governo e alla maggioranza come si possa continuare a lavorare così. Se andiamo ad esaminare rapidamente gli articoli, un po' per titoli e un po'

dell'istituto di credito sportivo, del PNRR, delle minoranze linguistiche (e potremmo continuare così), in palese violazione del dettato dell'articolo 77 della nostra Costituzione. Non ci sono - come dicevo - i criteri di urgenza e neanche ci sono dei criteri di valutazione solidaristica rispetto alle istanze e alle richieste dei cittadini italiani. Sappiamo che le urgenze sono altre, a cominciare dalla sanità e dal MES. Il 30 giugno è arrivato e vorremmo capire qual è la linea di questo Governo sul MES. Meloni ci deve venire a spiegare se si arriverà realmente a una ratifica. Abbiamo sentito che il ministro Giorgetti ha cambiato idea e questo è bene; ma vorremmo capire cosa intende fare la Presidente del Consiglio. Il MES è un atto importante di stabilità e di certezza, che andrebbe a migliorare certamente le tante urgenze urgenze che servono al Paese, come le liste d'attesa (due anni per le mammografie) e la carenza di medici e di infermieri. Queste sono le urgenze, questi sono i problemi di cui si dovrebbero occupare il Governo e il Parlamento.

il disastro del superbonus per le casse dello Stato. Ieri è emersa un'altra, ennesima truffa a Venezia, per 9 milioni e mezzo di euro; questo è successo nella città di Venezia, solo per ricordare l'ultimo episodio. inoltre ai crediti d'imposta: dopo otto mesi ci sono 33 miliardi di crediti incagliati e ancora non si trova una soluzione. soluzione. Noi continuiamo ad essere un'opposizione costruttiva e attenta; ci piace dialogare e confrontarci con il Governo, ma abbiamo messo in messo in piedi degli emendamenti importanti (penso alle colleghe e ai colleghi della Camera dei deputati), che ovviamente sono stati sonoramente bocciati. Penso anche a tutta la questione espressa dalla collega Bonetti sugli asili nido e sulle strutture per l'infanzia. E potrei continuare così. Ancora una volta sottoponete il voto di fiducia al Governo. Eppure lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto più volte, anche a fine maggio (poco meno di un mese fa). Ha convocato i Presidenti di Camera e Senato, richiamando l'attività legislativa di questo Governo e di questa Aula. Ancora una volta il Presidente chiedeva in maniera esplicita quale omogeneità ci fosse in questi decreti e quali fossero i criteri di urgenza. Io però posso ricordarvi - perché, ahimè, i numeri sono importanti - che il nostro sistema parlamentare si sta trasformando in un monocameralismo imperfetto. Dico imperfetto perché non è previsto nella nostra Costituzione, ma di fatto sta avvenendo, anche con il provvedimento al nostro esame, questo record di voti di fiducia.

dicendo, ancora una volta, che dovete rispondere delle urgenze, delle richieste e delle istanze espresse dai cittadini italiani. Noi vogliamo che il Governo ci venga a parlare di sanità, di PNRR, di infrastrutture, non andando soltanto alle inaugurazioni o ai tagli dei nastri, e che la stessa Presidente del Consiglio ci venga a riferire sul MES e sulla sua eventuale ratifica.

Chiediamo al Governo, riprendendo le parole del presidente Balboni a cui mi associo anche come Gruppo, di avere la possibilità di lavorare in maniera serena e rispettosa del Parlamento, prima di tutto facendo il nostro lavoro e il nostro dovere nelle Commissioni competenti. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

norme eterogenee. Nel mio intervento mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti che riguardano i temi che seguo maggiormente nella mia attività parlamentare. In particolare, sul tema della giustizia, ci sono sono alcune norme che vorrei sottolineare positivamente in quanto necessarie. In primo luogo, vi è la proroga dei termini per le notifiche via PEC previste per gli atti giudiziari della riforma Cartabia, che è assolutamente necessaria. Ci stiamo rendendo conto che le riforme ambiziose della scorsa legislatura necessitano di interventi strutturali all'interno degli uffici giudiziari e quindi questa proroga è assolutamente doverosa. Così come annoto con assoluto favore il ritorno, dopo il Covid, della prova scritta agli esami da avvocato. Viene lasciato Viene lasciato da parte l'orale rafforzato, che era uno strumento straordinario che è stato applicato nelle ultime sessioni di esame. Certamente, l'intervento normativo che stiamo discutendo riguarda la prossima sessione di esami, di esami, perché per quanto riguarda l'esame da avvocato bisogna fare anche una riforma più profonda, puntando soprattutto a risolvere due questioni: la necessità di una maggiore omogeneità di giudizio tra le commissioni di esame e la riduzione dei tempi. La parte più rilevante del mio intervento intendo dedicarla ad un altro tema che mi sta molto a cuore, che viene approfondito e risolto con questo decreto-legge: sto parlando del fondo indennizzo risparmiatori. che quello di oggi sia un giorno da cerchiare in blu sul calendario per i risparmiatori truffati dalle banche: mi riferisco in particolare all'articolo 4, commi 3-*bis* e *quater*, del provvedimento in esame.

poste in risoluzione qualche anno fa, in particolare la Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca, Carichieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria ed altre banche di credito cooperativo di minori dimensioni. una breve annotazione per ricordare come quelle banche, che furono poste in liquidazione coatta amministrativa, hanno pagato certamente la *mala gestio* degli amministratori, evidenziata poi in diverse condanne penali dai tribunali, ma certamente quei *crack* non furono dovuti soltanto alla *mala gestio* degli amministratori, ma anche a carenze e manchevolezze degli organi di controllo e vigilanza. Proprio tali manchevolezze hanno giustificato l'intervento legislativo di ristoro a favore di azionisti e obbligazionisti, previsto dalla legge di bilancio del 2019.

L'intervento di cui parlavo poc'anzi prevede che l'aumento dell'indennizzo per gli azionisti salga dal 30 al 40 per cento del costo di acquisto. Si tratta di un ammontare davvero ingente, per certi versi straordinario: a spanne sono circa 340 milioni - ripeto, 340 milioni, non un piatto di lenticchie

i truffati dalle banche hanno già percepito. Faccio un esempio semplice: se un'azionista ha ricevuto finora 1.000 euro, ora ne riceverà altri 333; e così tutti con la medesima proporzione. lo considero anche un successo personale, poiché l'aumento dell'indennizzo era stato l'impegno forse più solenne che avevo assunto nei confronti dei miei concittadini nella scorsa campagna elettorale, facendone tra l'altro oggetto di *spot* elettorali e interventi mediatici. L'aumento dell'indennizzo era stato anche oggetto di un ordine del giorno a mia prima firma, che l'intera Assemblea del Senato aveva condiviso nella seduta del 15 febbraio scorso. È quindi con mia grande personale soddisfazione che vedo quell'impegno tradursi oggi in legge. Tra l'altro, è una legge molto efficace che si applicherà in tempi assai ristretti: entro il 31 luglio indicare per i risparmiatori un nuovo IBAN, nel caso in cui avessero cambiato quello originario sul quale avevano ricevuto il primo bonifico, e seguiranno in tempi assai ristretti i bonifici del secondo indennizzo.

europei, ha accettato sul tema un confronto sereno e di merito, a conclusione del quale, gettato il cuore oltre l'ostacolo, ha dato semaforo verde a questo così significativo incremento dell'indennizzo. Questa giornata deve essere quindi di soddisfazione, di festa e di tributo alla politica, alla buona politica che si manifesta nella concretezza; non alla politica delle chiacchiere, ma dei risultati concreti che migliorano la vita delle persone. Dai nostri calcoli saranno circa 120.000 i risparmiatori che beneficeranno dell'incremento dell'indennizzo. In questo contesto vanno anche segnalate alcune criticità che permangono, che non vanno però enfatizzate

e il sistema telematico ad oggi non consente correzioni), alle difficoltà di provare le violazioni massive, alle domande prive di requisiti per l'accesso al regime forfettario che potrebbero essere valutate con quello ordinario, ad errori commessi da chi ha compilato le domande. Si tenga comunque conto che il fondo resta più che capiente, perché, anche al netto dell'incremento di indennizzo che oggi stiamo discutendo, restano a disposizione circa 150 milioni (è una cifra per difetto). Ciò premesso, attese le difficoltà interpretative, molti risparmiatori paiono essere decaduti dalle impugnazioni di questi rigetti. A mio giudizio - e mi rivolgo al Governo - si dovrà trovare un modo per consentire di poter ridiscutere le loro posizioni, permettendo a coloro che ne hanno i requisiti, e che hanno quindi commesso degli errori più o meno colpevoli ma comunque hanno i requisiti, di accedere al fondo che, come abbiamo già sottolineato, resta più che capiente. Qualche idea in proposito ce l'abbiamo e sarà nostra cura presentarla al Governo in altri provvedimenti prossimamente all'esame del Senato. Sono sicuro che le nostre proposte, come quella riguardante l'aumento dell'indennizzo, saranno adeguatamente vagliate dal Governo. Quindi, concludendo il mio intervento, non posso che riconfermare, a nome dell'intero Gruppo Forza Italia, la grande soddisfazione per l'approvazione dell'aumento dell'indennizzo a favore dei truffati dalle banche. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghi, siamo in uno Stato democratico. E in uno Stato democratico il potere va esercitato nel rispetto della popolazione e soprattutto nel rispetto delle persone. Ma come possiamo parlare di rispetto delle persone quando due figure apicali di enti come l'INPS e l'INAIL vengono cancellate dai loro ruoli con un colpo di penna? Come possiamo parlare di democrazia, quando viene utilizzato uno strumento, quello del commissariamento degli enti pubblici, in maniera strumentale, quando non ce ne sono le condizioni e soltanto per anticipare quella che era una scadenza naturale degli incarichi? Normalmente, lo strumento del commissariamento viene utilizzato se ci sono problemi di mafia, gravi crisi economiche dell'ente. Ma dov'è tutto questo? Chiediamocelo. Cosa ha fatto l'INPS per giustificare un attacco così forte, *ad personam*? Ha erogato, durante la pandemia, sessanta miliardi di euro ai cittadini. Ha chiuso l'ultimo bilancio con due miliardi di utile. utile. Ha raggiunto, addirittura, il 75 per cento degli obiettivi del PNRR. Capite che si tratta di un atteggiamento che vuole semplicemente mostrare forza, colpire, celebrare il proprio potere. È una questione di metodo. Osservando questa modalità di operare del Governo, a me viene in mente quella identificazione del potere con una parte della società che vuole, desidera e si fa coinvolgere dall'idea dell'uomo forte, dall'illusione dell'uomo forte. Ma il vero *leader* non è l'uomo che si impone e che non si interessa dei problemi degli altri: il vero *leader* è l'uomo che sa governare. È l'uomo che si sa confrontare, che sa piegarsi al rigore logico del ragionamento, che sa risolvere i problemi degli italiani, che si sa rendere conto che i problemi degli italiani, oggi, sono altri, che gli italiani hanno difficoltà a fare la spesa, che devono fronteggiare l'inflazione, che non possono pagare le bollette. L'uomo forte sa ascoltare, sa mettersi in discussione. Essenzialmente, si sa piegare al rigore logico del ragionamento e, soprattutto, sa trovare quelle soluzioni che devono essere democratiche e che devono rappresentare una orchestrazione delle differenze, anche nel rispetto di chi siede dall'altra parte, all'opposizione. Probabilmente, c'è una sorta di patto implicito, tra il Governo che vuole fare la voce grossa e chi ama farsi governare in questo modo. Il patto è che le glorie vanno condivise, ma per tutto il resto bisogna trovare un nemico e questo nemico va calpestato, così come vanno smantellate tutte le cose che ha fatto questo nemico. Quello che sta facendo questo Governo non è altro che fare un lavoro di smantellamento: e non parlo soltanto delle nomine, ma anche di quello che si sta facendo per il superbonus, con il reddito di cittadinanza: un lavoro per mettere fine a tutto ciò che ha fatto il vostro avversario. Almeno lasciate in pace due enti che hanno una funzione sociale importante. L'INAIL e l'INPS sono due enti che rappresentano un impegno dello Stato nei confronti dei cittadini. E se colpiamo questi due enti noi stiamo mettendo in discussione questo impegno. Vorrei fare ancora un'altra considerazione, colleghi, sempre su questo *modus operandi*.

Avete reso urgenti persino i provvedimenti sui *rave party*, creando una sorta di allarme sociale, come se ci fosse un proliferare di *rave party* a cui non si riuscisse a far fronte, come se non avessimo una normativa capace di intervenire in casi come quelli. Abbiamo perso tempo per i *rave party* e poi non avete tempo per occuparvi del PNRR e ci state facendo perdere i fondi che faticosamente il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto dall'Europa.

della forza. Come avete affrontato gli altri temi politici? Avete affrontato le politiche dell'immigrazione? No, non avete fatto politiche sull'immigrazione, avete fatto politiche contro gli immigrati, non avete fatto pianificazione,

Con la stessa modalità avete bloccato una misura di sviluppo che stava funzionando come quella del superbonus. Colleghi, fate una riflessione: state mettendo in difficoltà le imprese, quella misura creava occupazione, dunque andava stabilizzata, la potevate cambiare, ma non renderla completamente inefficace.

per come la state proponendo, state rischiando di condannare alla povertà intere Regioni italiane sulle quali non sono stati mai fatti investimenti infrastrutturali, Regioni sulle quali non è mai stato fatto alcun lavoro politico per metterle nelle condizioni di andare avanti e di creare sviluppo.

di Berlino ha fatto investimenti per evitare di mantenere quelle divergenze economiche tra due parti del Paese, oppure come la Spagna, che ha investito nelle infrastrutture, nella formazione, ha favorito investimenti esteri nelle aree economiche in maggiore difficoltà il Portogallo, che ha lanciato incentivi per chi investe nelle aree interne, perché ha capito che bisogna creare sviluppo e cercare di rimuovere le divergenze. Voi state andando nella direzione opposta.

il merito di alzare la voce, di accontentare quella parte della popolazione che vuole l'uomo forte, ma alzare la voce non risolve i problemi degli italiani, non li aiuterà a pagare le bollette a fine mese, non aiuterà quelle aree di crisi che ci sono in Italia, dove ci sono disoccupazione e povertà, dove bisogna fare sviluppo, che state abbandonando. Vi invito, colleghi, a fare una riflessione, perché nella politica non è importante solo alzare la voce, ma occuparsi dei problemi della gente. iscritta a parlare la senatrice Testor.

sentito l'ultima critica appena formulata sulla questione dell'autonomia differenziata. Vorrei ricordare che i fondi di coesione non vengono utilizzati e lasciatevi dire da una donna che viene da una terra dell'autonomia che autonomia significa responsabilità

ricordo qualcuno che da un balcone diceva di aver sconfitto la povertà, lasciando le persone alla ricerca del lavoro, senza mettere in atto politiche attive per il lavoro. Noi stiamo quindi

Un nostro emendamento dà ai responsabili del servizio finanziario dei Comuni la possibilità di rettificare i documenti allegati al bilancio 2022 e di adeguarli alla perdita di gettito connessa alla pandemia da Covid, riducendo i tempi burocratici e le lungaggini. È prorogata al 31 luglio la scadenza delle certificazioni di raggiungimento degli obiettivi riferiti ai servizi sociali, asili nido e trasporto pubblico scolastico per studenti con disabilità; viene prorogato al 15 agosto l'avvio degli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere

Grazie a un intervento del Governo, le Regioni che presentano un disavanzo *pro capite* superiore a 1.500 euro al 31 dicembre 2021 potranno ripianarlo in quote costanti nei nove esercizi successivi a decorrere dal 2023. Siamo intervenuti sul fondo di garanzia per la prima casa (anche in questo caso pensiamo ai giovani) estendendo la sua operatività fino al 30 settembre;

che sono state messe in campo non tenendo in considerazione le esigenze e i fiori all'occhiello del nostro Paese. Intanto, viene prorogato fino al 31 luglio il pagamento da parte delle aziende fornitrici, mentre si cerca di modificare questo sistema, dando tempo fino al 2026,

trovarsi a doversi rivolgere a forniture che arrivano dalla Cina o dai Paesi esteri. C'è stata l'introduzione del versamento di una quota del prezzo d'acquisto al Fondo sanitario

che potranno assumere a tempo indeterminato il personale per la ricerca sanitaria e le attività di supporto connesse, reclutato a tempo determinato, a condizione che abbia maturato al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio consecutivi, anche non continuativi, negli ultimi otto e che non abbia ottenuto due valutazioni negative dall'istituto che vuole procedere alla stabilizzazione. Anche in questo caso, si vogliono stabilizzare dei ricercatori. Con riguardo a questo punto, su cui le opposizioni il Governo ha dato una risposta, sono stati messi in campo 74 milioni per fare tale operazione e credo che vada riconosciuta al Governo la volontà di continuare di continuare a rimpinguare il sistema sanitario e la ricerca. È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per aderire alla rottamazione-*quater* dal 30 aprile al 30 giugno; slitta la scadenza per il pagamento della rata al 31 ottobre, mentre viene rinviata anche la scadenza fiscale con un meccanismo in due tempi, per cui si prevede un rinvio fino al 20 luglio senza alcuna maggiorazione, poi dal 21 al 31 luglio si potrà versare il dovuto con l'aggiunta di uno 0,40 Sono state fatte deroghe dei termini per quanto riguarda la materia fiscale. perché con un emendamento si sono voluti introdurre il riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua

da parte del Governo la sensibilità verso un'Italia che è diversa orograficamente, oltre che per storia e cultura,

Prima di concludere, vorrei aggiungere che con questo decreto è stato dato il via libera a 660 milioni di euro per gli alloggi universitari: sappiamo che è un tema molto importante, perché i nostri ragazzi

continua a lavorare, cercando di dare le risposte urgenti. Sicuramente, com'è stato evidenziato prima, avremmo voluto anche noi lavorare sul decreto-legge in esame, ma, come dicevo, i tempi sono stati ristretti,

come spesso accade, onestà intellettuale nel riconoscere i limiti a cui l'Assemblea e la nostra istituzione sono state sottoposte. Stiamo discutendo qualcosa - ringrazio anche la senatrice Testor per onestà intellettuale - di cui non abbiamo discusso nelle Commissioni e ci stiamo riferendo a ciò che i nostri colleghi hanno fatto

Questa discussione è diventata un rito, rispetto al quale, però, non possiamo non denunciare due cose. La prima è che siete diventati adulti e mi riferisco in particolare al Gruppo Fratelli d'Italia, la forza di maggioranza.

tanto ardore - si lanciava contro l'allora Presidente del Consiglio, per dire che il Parlamento veniva umiliato, perché si utilizzava la parola «urgenza» in pandemia, quando tutta quell'urgenza non c'era. Ciò

la senatrice Lorenzin sul punto), che era una riforma complessa, che era immotivato trattarla in quel provvedimento e che sarebbe stato opportuno discuterne. Oggi ce lo ritroviamo riprorogato, ma da voi.

Io apprezzo - lo dico anche alla Presidente, per il tramite del presidente La Russa - che dalle notizie di stampa nel Consiglio dei ministri di ieri sia stata

in questo avete superato anche chi vi ha preceduto. Vorrei però dire una cosa. Nella mia frustrazione di senatore della Commissione bilancio che voleva presentare emendamenti a questo decreto, parlando con i funzionari del servizio legislativo ho

con quello di incompletezza dell'attività amministrativa, che deriva dal fatto che, al di là dell'urgenza di alcune questioni, quando si fanno riforme,

analizzando quella che si chiama *evidence-based policy*, cioè l'impatto delle politiche esistenti, un'analisi degli obiettivi e come ci arriviamo. Allora, vedete, non ho nulla in contrario all'idea che magari l'INPS e l'INAIL possano essere ridisegnate come *governance*, ma prima vorrei capire perché, quali sono gli obiettivi, come ci arriviamo e quali sono i tempi congrui. Commissariare così, *d'emblée*, due o tre enti con un decreto, semplicemente rivela una cosa: l'occupazione del potere (*Applausi*). Questa sì che è urgente. L'occupazione del potere vostro è di un'urgenza enorme: INPS, INAIL, RAI, la stessa AIFA (con la modifica che è stata fatta). Cosa c'è dietro questa urgenza? C'è

che il regolamento del PNRR contiene una norma che è stata applicata alla Polonia e all'Ungheria, che si sono visti sospesi i finanziamenti del PNRR. Quando si viola lo Stato di diritto, la Commissione europea, come strumento sanzionatorio, può bloccare i fondi del PNRR. E si viola la *rule of law* (lo Stato di diritto) quando si minano l'indipendenza e l'autonomia di istituzioni che per legge devono averle e non possono essere commissariate dal Governo, soprattutto senza un disegno

guarda, ci chiede cosa faremo del PNRR, cerca di capire cosa succede sul MES, che è semplicemente uno strumento di ratifica, che possiamo utilizzare o no, ma soprattutto cerca di capire se, in questi anni così importanti, riusciamo a determinare una svolta che tutti ci auguriamo, perché è importante per il nostro Paese o - se vuole, Presidente - per la nostra Nazione. Ed è importante nella misura in cui riusciamo a incanalare una politica economica fatta di obiettivi e di strumenti chiari, per cui sappiamo cosa accadrà fra tre mesi e non stiamo a rincorrere i decreti di urgenza che di urgenza hanno semplicemente gli gli aspetti di errore e di controllo del potere. Ho iniziato dicendo che la fine è nota: è nota perché oggi siamo costretti a mettere la fiducia senza poter discutere nel merito un provvedimento. Proprio perché la fine è nota, vorrei concludere ricordando una frase del «Giulio Cesare» di Shakespeare, che recita «Se fosse dato all'uomo di conoscere la fine di questo giorno

basta che il tempo trascorra, che la fine di questi provvedimenti ci è già nota.

Grazie ringraziare il collega Nicita per avermi salutata, facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nasconderlo. Sto scherzando,

dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, avrà luogo nel pomeriggio di oggi a partire dalle ore 15,30.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore in data odierna di rivolgermi ai componenti di quest'Assemblea per relazionare in ordine alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge con il quale vengono introdotte misure urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Mi soffermerò solo su alcuni punti importanti del provvedimento. L'articolo 1, ai commi 1 e 5, introduce un complesso di modifiche rilevanti per gli istituti INAIL ed INPS: viene eliminata la figura del vice presidente per ciascuno dei due enti

prevista l'eventuale figura del commissario per entrambi gli istituti, ai commi 2 e 4, per ordinaria e straordinaria amministrazione. L'articolo 3 interviene sul sistema sanitario della Regione Calabria. I commi 1 e 2 prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del servizio sanitario della Regione Calabria. Si prevede inoltre che i commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L'articolo 3, comma 3, stabilisce che ai subcomissari delle Regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* Grazie a tutti la sospensione delle attività e dei procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pari a 100 euro, previste per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid. L'articolo 3-*ter* dispone norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per finalità di rafforzamento strutturale degli istituti. L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. Il comma 1 riapre i termini per aderire alla rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per aderire è posticipato al 30 giugno 2023. L'articolo 4, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e dunque di tassazione degli immobili ad uso produttivo e a destinazione speciale disposta dalla legge di stabilità 2016, individuando altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria. L'articolo 4-*ter* è volto a sospendere fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo per gli avvocati di effettuare con specifiche modalità le notificazioni degli atti nei procedimenti civili, nel caso in cui quella telematica non sia possibile o non abbia esito positivo. L'articolo 4-*quater* prevede la proroga della disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione forense per la sessione 2023. L'articolo 4-*quinquies* introduce la proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroalimentari colpite dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. L'articolo 4-*sexies* proroga i termini in materia di agevolazione per l'acquisto della casa di abitazione. prevede un finanziamento di 39 milioni di euro, per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. L'articolo 6-*bis* prevede la proroga dei termini dei contributi ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. L'articolo 6-*quater* prevede la proroga dei termini per l'accesso al fondo per l'utilizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva. L'articolo 7 differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, dev'essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e ai centri polifunzionali per i servizi della famiglia (risorse previste nel PNRR, missione 4). L'articolo 7-*ter* è volto a consentire che fino al 31 gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie ordinarie (professioni agrotecniche, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato). il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere da parte dei congiunti degli infoibati un'apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni - anziché venti, come attualmente previsto - dall'entrata in vigore della medesima legge. per il suo tramite vorrei condividere con i miei colleghi, soprattutto di minoranza, una semplice riflessione: ho svolto un'analisi dei vari articoli, proprio per dimostrare che anch'essi avrebbero potuto utilizzare il tempo a disposizione per approfondire l'utilità del contenuto di questo provvedimento. Ho fatto il sindaco per due mandati, quindi ho l'impostazione, ma anche la *forma mentis* dell'amministratore pubblico, che entra sempre nel merito dei provvedimenti, perché il fine ultimo, quando si fa politica, è dare risposte ai cittadini. Questo è un provvedimento che, per il rispetto delle tematiche e dei tempi, necessita dell'approvazione oggi,

Oggi, affinché possano essere efficaci da subito gli effetti di questo provvedimento, anche in ragione di alcune scadenze legate agli interventi del PNRR, è importante votarlo. Quindi, come Gruppo di maggioranza, lasciamo le polemiche pretestuose alla minoranza, che ha perso ancora una volta l'occasione per approfondire delle tematiche e dare risposte ai cittadini. Continuiamo a lavorare, con l'approvazione di tutti i provvedimenti necessari, con un alto senso di responsabilità e nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi,

Giorgio Napolitano rappresenta il testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione. La politica, in effetti, si fa cultura se si radica su idee e valori. E stare da una parte non significa essere necessariamente di parte. La cultura, peraltro, si fa istituzione se le procedure, le prassi, i leggendari precedenti e le convenzioni costituzionali sono sottratti alla casualità casualità e alla mera contingenza e si radicano sui principi, quantomeno sui propri princìpi. Per Giorgio Napolitano politica, cultura e istituzione sono vita, sono passione, ma anche razionalità e coerenza con la sua appartenenza politica. La ragione politica per Giorgio Napolitano è anche ragione storica,

Grazie a tutti

e, a un certo punto, il presidente Napolitano mi disse: «Ignazio, vedo più te che mia moglie, ultimamente». Non posso sapere se fosse un complimento o un'espressione

l'attenzione certosina con cui assolveva, oltre che al ruolo di Presidente della Repubblica, a quello che ne discendeva, ovvero il ruolo di Capo delle Forze armate. Non ho conosciuto, durante la mia permanenza nel Governo, altri Presidenti della Repubblica, ma dubito che altri siano stati così puntigliosi e così attenti nel tutelare le Forze armate, il loro onore, la loro qualità e la loro necessità di essere considerate uno dei momenti fondamentali della comunità

ricordo che persino nella maggioranza, o forse soprattutto nella maggioranza di Governo, vi era in quel momento qualche voce distonica, che voleva limitare al massimo quelle celebrazioni. Ricordo perfettamente

d'Italia venissero celebrati adeguatamente e per riuscire a vincere quella battaglia dal Consiglio dei ministri telefonai al presidente della Repubblica Napolitano e la sua parola fu decisiva affinché poi la celebrazione avvenisse con l'importanza con l'importanza con cui tutti ricorderete che avvenne, con la sua assidua partecipazione. Era un modo per ricordare a tutti che il Presidente della Repubblica rappresenta la storia d'Italia nella sua attualità, ma anche per tutti gli anni della nostra unità. Grazie, presidente Napolitano: spero di vederla ancora tra di noi in quest'Aula. Auguri, Presidente*.*

Signor Presidente, la ringrazio per le parole che, esprimendo il pensiero di tutti noi, ha appena rivolto all'Assemblea del Senato. Trovo estremamente significativo che il Senato abbia deciso di indirizzare i propri auguri al Presidente Giorgio Napolitano che domani compie novantotto anni. Lo trovo estremamente significativo perché stiamo parlando di una delle personalità politiche più insigni dell'Italia postbellica, un dirigente che ha iniziato il suo percorso politico partecipando alle battaglie civili e sociali più importanti della sinistra italiana. Egli fece il suo ingresso in Parlamento, come lei ha ricordato, esattamente settant'anni fa, nel giugno 1953, e nel corso della storia della Repubblica ha via via acquisito, da uomo di partito, lo spessore e l'autorevolezza tipici degli uomini delle istituzioni e degli statisti. Proprio nell'adempimento delle funzioni di alta garanzia, prima come Presidente della Camera per due anni, poi per nove anni come Presidente della Repubblica, ha offerto al nostro Paese prove non dimenticabili di equilibrio e coraggio nelle scelte, di rispetto e correttezza nel rapporto con i rappresentanti di posizioni politiche diverse dalle proprie, di attaccamento sincero e determinato all'interesse del Paese, di senso di responsabilità nazionale, di sobrietà e disciplina nell'adempimento delle cariche pubbliche, di dedizione assoluta alla causa europeista e di convinzione profonda - questo voglio sottolinearlo con forza della estrema importanza di lavorare sempre per accrescere il peso, la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel campo delle relazioni internazionali in generale e in particolare in quelle occidentali ed euroatlantiche. Ritengo che un modo adeguato di accompagnare i calorosi auguri del Senato a Giorgio Napolitano, per il ragguardevole traguardo che sta per tagliare, consista anche nel serbare memoria delle parole alte e illuminanti che, presiedendo quest'Assemblea come senatore anziano nel marzo 2018, egli rivolse con energia e garbo ai colleghi più giovani. Era l'inizio della XVIII legislatura ed io ebbi il non piccolo onore di essere tra costoro e posso assicurare che fu un momento - chi c'era lo ricorderà - di grande emozione e di grande valore politico e civile. Infine, pensando anche a molti dibattiti importanti che oggi sono in corso e che ci vedono tutti impegnati con passione, con grande attenzione alle nostre idee, non posso in questa sede non sottolineare il grande interesse Giorgio Napolitano ha sempre riservato alla materia delle riforme istituzionali, unendo l'apertura alle riforme necessarie, che in lui non è mai mancata, con una straordinaria fermezza nella difesa dei valori di fondo della nostra Costituzione, a partire dall'equilibrio tra i poteri che essa fissa indelebilmente e dalla coesione territoriale e sociale del Paese, che non può mai essere persa di vista in quanto principio essenziale e irrinunciabile, al quale Napolitano, da uomo di Stato e da uomo del Mezzogiorno, si è sempre mostrato legatissimo. Questa lezione è stata, e io credo resterà, preziosissima. Auguri di cuore Presidente.

Vorrei solo ricordare - visto che si tratta del riconoscimento di settant'anni di vita parlamentare di Giorgio Napolitano la grandissima attenzione che, nei rapporti che ho avuto occasione di avere con lui, gli ho sempre visto rivolgere al Parlamento; anzitutto al Parlamento europeo, nell'ambito del quale l'ho visto per la prima volta all'opera in anni ormai lontani, non solo come parlamentare esemplare, ma come Presidente della Commissione affari costituzionali, dove ha ricoperto un ruolo importantissimo. Devo anche dire che quando successivamente, nel novembre 2011, mi ha chiesto di formare e guidare un nuovo Governo in situazioni complicate, di fronte alla mia obiezione sulla mia inesperienza politica, la sua risposta fu che io, come commissario, quindi come membro del Governo europeo, avevo avuto per dieci anni un rapporto ottimo e profondo col Parlamento europeo. Ricordo infine che, nell'attività che per un anno mi vide molto vicino al Presidente e nella quale egli fu di uno scrupolo totale nel rispettare le prerogative del Governo e del Parlamento, pur essendo un Capo dello Stato che in quel momento aveva una particolarissima autorità nei confronti del Governo, in quel periodo una delle cose che lo resero particolarmente soddisfatto fu una legge che il Governo propose e il Parlamento approvò - quella del 24 dicembre 2012 2012 - legge che, tra l'altro, richiede al Presidente del Consiglio di recarsi in Parlamento prima di ogni Consiglio europeo. È una legge che da allora non è stata disattesa da alcun Capo del Governo e che e che cementa un rapporto molto profondo tra il Parlamento e l'Esecutivo nelle congiunture più rilevanti per le decisioni europee del resto oggi pomeriggio, quando ascolteremo la presidente Meloni, questo sarà nel solco di quella legge che il presidente Napolitano vide con particolare favore. Mi unisco agli auguri di tutti prego il professor Giulio Napolitano, presente in tribuna e che saluto, di portare al Presidente anche i miei particolarmente devoti e grati auguri per la fiducia che ha dato a me, ma soprattutto per la grandissima lezione che ha dato e sta dando a tutti noi.

e domani, come giustamente veniva ricordato, compirà novantotto anni. Nell'augurargli buon compleanno e nel

in questo momento una gratitudine enorme al presidente Giorgio Napolitano e vogliamo rendere onore ai suoi nove anni al Quirinale.

Ho avuto poi l'onore e la fortuna di poterlo votare come Presidente della Repubblica. Un fiero europeista, un riformista, che ha favorito le relazioni del nostro Paese con gli altri *partner* europei, mostrando però sempre vigore anche nei momenti di maggiore difficoltà, sia politica che economica. Tra le tante riflessioni che ha lasciato nel corso degli anni voglio ricordare anche quella puntuale e sempre attuale sulla giustizia. «La riforma della giustizia non è più rinviabile». Deve essere compito Deve essere compito del Parlamento «restituire efficienza a una macchina giudiziaria lenta e caotica, il cui funzionamento è largamente insoddisfacente»: queste le sue parole nel 2014. Intendo ringraziare ancora una volta in questa sede il presidente Napolitano per l'alto senso delle istituzioni che ha incarnato e incarna ancora oggi. Faccio riferimento, in particolare, al momento in cui ha accettato di continuare a rappresentare e a garantire il nostro Paese, da Presidente della Repubblica, anche dopo la scadenza del suo ordinario settennato, accettando di essere rieletto come Capo dello Stato. Una scelta, anche quella volta, di grande responsabilità, nell'esclusivo interesse del Paese, che viveva un grave momento di crisi, non solamente economica e sociale, ma anche e soprattutto politica.

bene - in quei giorni, rispetto ad alcune scelte di politica nazionale e internazionale che si andavano a compiere. Fu quindi un uomo di grande rigore, di responsabilità, ma sempre attento

di lavorare in questa sede, nell'esclusivo interesse del nostro Paese. Grazie, presidente Napolitano e grazie alla sua famiglia, a cui chiediamo di portare gli auguri, anche da parte del mio Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope.

Si deve, allora, procedere per titoli, e questi titoli sono: «un riformista» e «un uomo delle istituzioni». Il presidente Napolitano è stato un riformista, quando questa parola non andava di moda e, anzi, in alcuni ambienti politici veniva usata in senso dispregiativo. Meglio di altri, egli ha saputo dimostrare che il riformismo non è un cedimento, ma è la cultura politica di chi vuole davvero migliorare la vita delle persone. Da uomo delle istituzioni, la sua resta un'impronta indelebile. Un Presidente che ha dimostrato come, nei dettami costituzionali, nella forza delle istituzioni, il Paese ha le energie per uscire anche dalle crisi più drammatiche e minacciose. Giorgio Napolitano tornò in Senato dopo il periodo alla Presidenza della Repubblica, il 14 gennaio 2015. Quello stesso giorno aderì al Gruppo Per le Autonomie. In una pubblicazione del 2018 spiegava che la sua adesione al Gruppo Per le Autonomie è stata certamente motivata dal convinto apprezzamento per una rappresentanza plurale come quella garantita dal Gruppo e per lo sforzo di obiettività, senza spirito di fazione e senza rissosità, cui sono stati e sono tuttora improntanti l'orientamento e il comportamento del Gruppo. un fatto che ci ha sempre riempiti d'orgoglio e che segnala, tra le varie cose, lo storico legame tra senatori a vita, Presidenti emeriti della Repubblica, ex Presidenti del Consiglio e rappresentanti delle autonomie speciali. In questa antica consuetudine abbiamo sempre visto una volontà di segnalare all'arco parlamentare come il tema delle minoranze non fosse una questione secondaria, ma il termometro per misurare lo stato di salute delle istituzioni repubblicane, quelle istituzioni che il presidente Napolitano ci ha insegnato a rispettare e a valorizzare. Il suo impegno e la sua storia sono un grande esempio e lascito per le future generazioni. Buon compleanno, presidente Napolitano!

senatore Guidi onora sempre il Senato della sua presenza ed è di esempio a tanti per la sua assiduità in

non riesco a non aggiungere la mia voce un po' stonata su Giorgio Napolitano, perché ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie. Al di là delle leggi, dei dibattiti, dei conflitti, delle complicità, qualche volta anche un po' forzate, la conoscenza di persone straordinarie, non sempre famose e non sempre storiche, come il presidente Napolitano,

non solo Giorgio, ma Nilde Iotti e Giorgio Almirante, persone straordinarie, che coniugavano la forte scelta partitica, alla quale non hanno mai rinunciato, in qualche caso in maniera formidabile, al senso dello Stato. Mi ricordo Nilde Iotti che in occasione di una se non ce la faceva più a camminare, un po' come me oggi; lei sempre elegantissima, perché doveva dimostrare

stanchissima. La stessa cosa ha fatto Napolitano, coniugando un mistero, sul quale mi interrogo spesso, avendo avuto la fortuna - come lei ha detto, Presidente - di passare molti anni in Parlamento (molti dicono troppi, ma va bene così, sono felice di averlo fatto e di esserci ancora): il senso dello Stato e, nonostante tutto, di essere in parte grande di parte. Questo essere faziosi senza far torto alla democrazia e alla Costituzione credo che sia un miracolo che fa parte della forza e della volontà di questa scelta, io direi quasi santa, di essere tra noi per essere testimonianza di democrazia difficile, perché la democrazia non è mai facile. Non c'è giorno della mia vita nel quale in Parlamento io abbia vissuto un momento di scelta facile e non sofferta. Io feci un libro (scusate se mi cito, poi finisco, Presidente, glielo assicuro): il dolore in politica, la politica del dolore. Giorgio Napolitano ha saputo gestirla. Però mi deve permettere un ricordo. Subito dopo le elezioni del 1994, io diventai, forse inopinatamente, Ministro della famiglia, nell'anno della famiglia. Guarda un po', Silvio Berlusconi scelse una persona, non so se valida o no, ma certo con disabilità, facendo una scelta culturale della quale ancora oggi si hanno riflessi positivi al di là della Dovetti andare al convegno mondiale «Demografia e sviluppo» e feci conoscere alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato il mio discorso.

politicamente, le mie scelte, l'aver lasciato il sindacato per andare nella destra, ma di rispettare la mia scelta di vita. Scriveva: oggi le faranno un trabocchetto, lei resista, perché io sto con lei. Era una senatrice che diceva che non potevo andare al Cairo a rappresentare l'Italia per la mia disabilità e per altri tipi di scelte.

...anche un po' antipatico (perché no?), ma nonostante tutto intellettualmente onesto. Ecco, forse il mistero è svelato:

posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

oggi all'esame dell'Aula c'è un provvedimento sicuramente eterogeneo per materia nei suoi contenuti, ma ricco di elementi positivi che incidono concretamente su temi come sanità, piccoli Comuni, fisco, caro affitti, solo per fare alcuni esempi. In questo mio breve intervento mi limiterò ad evidenziare alcuni aspetti. In questi ultimi mesi questo Governo e questa maggioranza di centrodestra in Parlamento ha ascoltato, in maniera sempre costruttiva, chi - come i nostri giovani - protestavano giustamente, ad esempio, contro il cosiddetto caro affitti. Dal Governo e dal Parlamento arriva una prima risposta concreta: grazie al lavoro fatto sono state anticipate risorse europee per un primo intervento rapido sull'*housing* universitario sbloccati 660 milioni dei 990 previsti per costruire nuove residenze universitarie e creare nuove posti letti. Soprattutto sulla sanità e l'annosa carenza di medici e personale sanitario, c'è una dovuta premessa da fare, su cui vorrei che ci trovassimo tutti d'accordo: è un problema che questo Governo e questa maggioranza ereditano dal passato. La carenza di medici e di sanitari è un'emergenza nazionale, che va risolta in maniera seria con soluzioni strutturali. Con questo provvedimento abbiamo solo dato prime risposte, con un emendamento approvato che consente ai medici iscritti al secondo anno di specializzazione medica di partecipare a concorsi come dirigente medico, ad esempio. Sono convinto che nei Ministeri ci sia oggi la dimostrazione che c'è voglia di voltare pagina. Per uscire dalla logica dell'emergenza, infatti, bisogna programmare e per programmare - come sappiamo tutti noi - c'è bisogno di avere una visione. Ecco perché diventa importante l'impegno del Governo di aumentare i posti nelle facoltà di medicina per consentire a più studenti di intraprendere questo percorso formativo. Sarà poi il merito

il Paese dei mille campanili. A questa realtà vogliamo dare attenzione ed oggi lo facciamo concretamente prorogando i termini per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche, e ancora prorogando la data di avvio di lavori proprio per andare incontro alle amministrazioni più piccole che soffrono di carenza di personale. Quanto alla rottamazione fiscale, nella manovra approvata nello scorso dicembre è stata introdotta la cosiddetta tregua fiscale: parliamo di 140.000 cartelle coinvolte. Con questo provvedimento Con questo provvedimento la nostra maggioranza ha approvato un emendamento che sposta in avanti i termini per la presentazione delle domande al 30 giugno, e posticipa al 31 ottobre 2003 il pagamento della prima rata. Siamo per un fisco amico dei cittadini, alleato delle risorse delle famiglie e delle nostre imprese. Analogamente, siamo dalla parte dei giovani che credono nel futuro e nella possibilità di costruirsi un domani, e per fare questo serve sicuramente il lavoro. Vorrei commentare il dato positivo dell'Istat di ieri sulla disoccupazione giovanile, che cala di 1,4 punti nel 2023 rispetto allo scorso anno. È un segnale positivo del buon lavoro fin qui svolto dal Governo e dalla maggioranza in Parlamento. I nostri giovani vogliono lavorare e non restare a casa, e vogliono giustamente anche costruire una propria casa. Ecco perché, in questo contesto, diventa rilevante l'emendamento approvato dalla maggioranza in Commissione bilancio alla Camera, che interviene proprio sul fondo di garanzia per la prima casa. Tale fondo sarà operativo dal 30 settembre 2023 ed è uno strumento utile e importante per garantire ai giovani una possibilità in più, un sostegno rilevante nel momento in cui chiedono il mutuo per l'acquisto della prima casa. Tutto ciò basta? Certamente no, c'è moltissimo da fare. Siamo consapevoli che bisogna fare molto di più. Mi riferisco alla politica monetaria della BCE, tema che certamente non può essere approfondito in questa sede, ma che sta causando un incremento dei tassi e quindi il relativo incremento delle rate dei mutui. È un problema dai dai contorni sicuramente più ampi e che merita una giusta riflessione da parte di tutti. Va individuata una soluzione e va pensato, a nostro avviso, una sorta di scudo che possa proteggere le famiglie meno abbienti e le imprese, soprattutto quelle più piccole, dal rischio di una nuova pesante stretta sulla liquidità. Concludo con due note, concerne il fondo indennizzo dei risparmiatori. Grazie a un emendamento l'indennizzo è salito al 40 per cento, un importante segnale di concretezza e di sostegno per 140 famiglie di risparmiatori traditi. Un secondo importante traguardo riguarda, infine, 39 milioni di euro stanziati per i giochi olimpici di Cortina e Milano del 2026, perché comunque mettiamo l'Italia in vetrina. Si tratta di un investimento sull'Italia. Stando a uno studio, su 1 miliardo di investimenti, per l'Italia ci sarà una ricaduta positiva pari a circa 3 miliardi di euro. Altro che la politica dei no: con il centrodestra alla guida dell'Italia, la storia è cambiata e il vecchio registro è ormai un lontano ricordo. Per questo, annuncio il voto favorevole da parte del nostro Gruppo.

perché siamo di fronte ancora una volta a un Governo che rivendica, giustamente, di essere un Governo politico, ma che usa la decretazione

unica. Poiché, però, da sola non funziona, continuate a fare proroghe. Affrontiamo il problema. Un Governo, se non è un governo autoritario, dovrebbe essere un Governo politico e quindi venire in Parlamento a discutere di merito e trovare le soluzioni.

in modo corretto gli enti. Vengono sostituiti perché? Perché c'è una discussione tra di voi, che è pubblica, per cui non vi siete ancora messi d'accordo su come fare le spartizioni di tutti gli enti. Quindi, intanto fate il il commissariamento e poi trovate la soluzione. Ma questo non è un modo corretto di applicare lo *spoils system*. Questo è un modo per occupare il potere e, sostanzialmente, rispondere a chi comanda.

Sono neofita del Parlamento e non ho una lunga esperienza, ma avete già superato i limiti degli altri. Capisco che la decretazione si usi in un Governo cosiddetto tecnico, ma perché un Governo politico deve continuare a mortificare il ruolo dei senatori e delle senatrici o dei deputati e delle deputate

la maggioranza tenderà a non modificare nulla, ma allora si tratta sostanzialmente di un'imposizione, che è quello che state facendo. Ma se è questa la democrazia che avete in mente, francamente è una democrazia monca. Capisco che nel momento in cui si pensa che è necessario centralizzare molto, alla faccia di chi pensa all'autonomia differenziata che risolverà le sorti di questo Paese - da una parte avremo venti staterelli e dall'altra uno Stato centrale forte - si prospetta un Parlamento complessivamente debole. Se questo è il modello

Per questa ragione, voteremo contro questo provvedimento. rappresentante del Governo, mi riallaccio a quello che ha appena detto il senatore Magni ed esprimo una riflessione sull'intervento della collega Spinelli, che apprezzo perché dettato dalla sua esperienza di amministratrice, che è anche parallela alla mia, quindi l'ho ascoltata con attenzione. Credo che nessuno qui discuta sul fatto che ci siano in questo provvedimento anche disposizioni valide, ma il Senato, come ha detto il senatore Magni, dovrebbe essere un luogo di discussione e di concertazione, non di mera ratifica delle decisioni dell'Esecutivo, cosa che invece di fatto, in questo caso ma anche in altri, è. Sono già state espresse, nel dibattito generale, tante considerazioni relative alle diverse e numerose criticità conseguenti alle diverse modifiche e integrazioni apportate a più norme dal presente provvedimento. In gran parte le condivido e quindi evito di ripeterle. Mi soffermo, però, sul commissariamento di INPS e INAIL, di cui all'articolo 1, perché è indice della mancanza di attenzione istituzionale che caratterizza l'attuale compagine di Governo. Prendiamo l'esempio dell'INPS. È comprensibile che un Governo come quello in carica non veda di buon occhio un presidente scelto dal MoVimento 5 Stelle e un vice presidente scelto dal Partito Democratico e si faccia venire in mente di farli decadere anzitempo e di sostituirli abolendo la figura del ma prima di tutto dovrebbe stare a cuore a chi ci governa la continuità affinché la gestione dell'ente sia la più efficiente possibile. A tal fine, un comportamento adeguato sarebbe stato

Giulio Andreotti rispetto al pensar male, quindi non proseguo perché sapete come va a finire. Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo Per le Autonomie

che auspicava un maggior coinvolgimento del Parlamento ricordandoci che non ci sono state le condizioni per chiudere l'*iter* in Commissione del provvedimento

nemmeno di avviare una minima discussione e questo mi fa manifestare un personale imbarazzo a intervenire in dichiarazione di voto. L'imbarazzo parte dal nome che noi stiamo dando alle cose: decreto *omnibus.* Quella di decreto *omnibus*

tutto; è un ossimoro perché la decretazione, in quanto strumento eccezionale, dovrebbe fondarsi sulla necessità ed urgenza, ma se tutto è necessario ed urgente, niente è necessario ed urgente. Questa confusione semantica e giuridica tradisce un dato politico che mi preoccupa molto: la miopia di inseguire sempre ciò che è urgente, perché non si ha la chiarezza su ciò che è prioritario per l'azione politica. Così si sopravvive, non si governa un Paese come l'Italia; così si occupa il potere, non lo si esercita. Qui torna il mio imbarazzo. Poche settimane fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha interloquito con i Presidenti di Camera e Senato per ammonirci sull'abuso della decretazione d'urgenza. Io sono in imbarazzo per quando i Presidenti di Camera e Senato dovranno risalire al Colle e spiegare come sia stato possibile che questo Parlamento abbia approvato un decreto-legge definito *omnibus.*

o fossero entrate nel merito della discussione, avrebbero svolto il loro servizio al Paese. Anch'io sono stato un amministratore e la mia preoccupazione e il mio imbarazzo nascono dal fatto e anche le dichiarazioni di voto dei suoi colleghi *(Applausi)*. Per esempio, alla Camera, in una dichiarazione di voto, un suo collega ha detto che in realtà l'omogeneità nasce dal fatto che c'è un interesse pubblico. Colleghi, se l'omogeneità nasce dal fatto che l'interesse pubblico fascia provvedimenti così diversi, di che cosa stiamo parlando? di che cosa stiamo parlando? Non è così, altrimenti potremmo anche dire che l'articolo 77 della Costituzione non lo si utilizza più e andiamo avanti.

INPS, INAIL, RAI: sostanzialmente un modo con cui fare fuori Fuortes dalla RAI e piazzarlo in un altro ente pubblico diventa oggetto di un provvedimento.

conoscendo le difficoltà che i cittadini calabresi incontrano nella gestione del servizio sanitario in quella Regione. L'articolo 4 si occupa di fisco con la proroga dei termini in materia fiscale, riaprendo i termini per la cosiddetta rottamazione-*quater*. Dunque INPS, INAIL, RAI,

e vuole approvare alcune norme del provvedimento che ritiene utili - io, per esempio, ritengo che avere prorogato i termini in materia di agevolazione per i mutui degli *under* 36 sia una cosa giusta - ma come facciamo a votare a favore, se non ci mettete neanche nelle condizioni di potervi dare una mano nel sostenere questi provvedimenti?

L'articolo 6 è una perla: si differisce dal 31 marzo al 31 dicembre il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR. Vi ricordo che siamo partiti da INPS e INAIL, passando per la RAI. Infine, ce ne sono tanti, ma ne ne cito due. Prima la senatrice Testor ricordava un'altra misura, secondo me giusta e utile, vale a dire l'estensione dell'utilizzo della LIS, della lingua dei segni anche per le minoranze linguistiche: certo, avremmo voluto sostenerla. Peccato che non ci avete dato la possibilità di farlo.

State dando un mese di tempo. Pensate veramente che offrendo un mese di tempo si possa trovare una soluzione a un problema così strutturale? La verità è che ci ritroveremo da qui al prossimo mese con un altro decreto *omnibus*, perché ragioniamo di scadenza in scadenza. scadenza. Che cos'è urgente allora? È urgente aumentare, per esempio, il valore dei francobolli per poterli utilizzare a fini solidaristici o è urgente il fatto che il 30 giugno scade la ratifica del MES, su cui ancora non abbiamo capito quale sia la posizione del Governo? L'imbarazzo - e con questo concludo, annunciando ovviamente il voto contrario del Gruppo Azione-Italia è che, procedendo di decreto in decreto e di fiducia in fiducia, non solo si svuotano le prerogative della funzione parlamentare, ma si rincorre la scadenza dei singoli termini, senza determinare quello che dovrebbe fare un'azione di Governo, vale a dire indicare le priorità importanti per il Paese.

detto riguardo alle critiche sullo strumento della decretazione d'urgenza o sulla posizione della questione di fiducia, che ho sentito fare negli interventi precedenti, dal senatore Magni e da altri colleghi, anche in Commissione. È una critica sensata e anche il presidente Balboni, in Commissione,

così che quando si è in maggioranza si dica una cosa e quando si è all'opposizione se ne affermi un'altra. La verità è che il concetto di urgenza è divenuto totalmente diverso da quello immaginato dai nostri Padri costituenti, quando non c'era un'intrecciata pervasività tra finanza, economia, tessuto industriale e produttivo, esigenze sociali e, non ultimo, il diritto europeo e la sua osservanza. Oggi c'è una società veloce, immediata e interconnessa, in un assetto istituzionale ormai molto composito, con uno Stato frapposto tra Unione europea e Regioni. Tutto questo crea un nuovo tipo di urgenza, che non dipende, come alcuni hanno detto, da un difetto di programmazione,

l'esigenza immediata di tutelare il cittadino, nei confronti del quale si riverberano gli effetti delle norme in questione, sia quando lo riguardano direttamente, sia quando riguardano enti pubblici e aziende. Nel merito, il provvedimento riprende le fila di alcuni temi rimasti incompiuti e che necessitavano di essere portati a termine. Molte sono le norme per prorogare i differenti termini in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell'artigianato. Diverse sono state le proposte inserite nel testo, anche dopo gli emendamenti del nostro Gruppo alla Camera Durante l'esame sono state affrontate tante criticità e prorogate anche scadenze proposte per risolvere questioni e situazioni pendenti, relative anche all'attuazione di alcune parti del PNRR. La materia del PNRR si insinua in modo continuo, infatti, nelle disposizioni che regolano le norme della pubblica amministrazione, e quindi richiede continui affinamenti per arrivare a ottimizzarne i risultati. In questo modo si affinano anche i meccanismi con i quali la pubblica amministrazione può riuscire ad utilizzare al meglio gli investimenti pubblici. Sono misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che sono fondamentali anche per ottenere la quarta rata.

all'ordine del giorno dopo la crisi per l'emergenza sanitaria da Covid-19 - all'autorizzazione da parte della Commissione europea, in attuazione delle riforme del PNRR. In questo modo, gli impegni del Governo e del ministro dell'università e della ricerca Bernini possono essere rispettati. Sappiamo quanto sia diventato costante e centrale il tema degli alloggi per gli studenti. La strada intrapresa è quella giusta, per realizzare un *housing* studentesco sempre più sostenibile. Poi c'è un'altra norma, che differisce a fine giugno il termine per gli interventi infrastrutturali legati agli asili nido. È un'altra questione importantissima, perché si tratta di scuole per l'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, realizzati con i fondi del PNRR. Sono state introdotte norme anche a favore degli enti locali. Vengono semplificati i procedimenti per i piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti. Si tratta di realtà territoriali molto piccole, che spesso incontrano difficoltà per realizzare opere pubbliche e ricorrono a professionalità esterne all'amministrazione, non perdere i contributi, non avendo all'interno, appunto, tutte le figure richieste. Teniamo conto del fatto che sono quasi 2.000 i Comuni con meno di 1.000 abitanti, che sono chiamati a realizzare opere molto importanti per la loro comunità. Parliamo di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Capiamo appunto come queste attività possano riguardare direttamente la vita di molti cittadini. Si è affrontata poi con decisione l'emergenza del Servizio sanitario nazionale, a causa della carenza di medici e di personale sanitario. È un tema che ricorre in tutte le realtà territoriali, a causa del quale viene compromesso il livello di assistenza sanitaria dei cittadini. Ora vengono facilitati l'assunzione e l'utilizzo di medici specializzandi che siano iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica. Nel decreto poi sono anche presenti importanti disposizioni che riguardano il sistema sanitario calabrese. Le misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria adottate lo scorso anno vengono prorogate al 31 dicembre. Si tratta di un intervento straordinario, che ha bisogno ancora di un po' di tempo, considerata la disastrosa situazione iniziale, anche finanziaria, I programmi operativi proseguono molto bene verso i piani di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. Gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria potranno adottare il bilancio di di esercizio del 2022 entro la fine di giugno 2023 e potranno inoltre deliberare i bilanci pregressi, che non sono stati ancora adottati, entro la fine del 2024. Sono in corso attività di revisione contabile dei fornitori, ma anche il monitoraggio e la gestione del contenzioso; proseguono le procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture. Ecco perché si sono rese urgenti e necessarie queste ulteriori disposizioni, ora trasferite in questo decreto. Sono norme concrete e immediatamente operative, legate alla gestione dei bilanci; ma soprattutto queste disposizioni tecniche sono fondamentali, perché lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi connessi al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, che riguardano tutti i cittadini calabresi. Vengono inoltre riaperti i termini per l'adesione alla cosiddetta rottamazione *quater*, prevista la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole e agroindustriali nei territori colpiti dal sisma del 2012, è stata prevista l'estensione fino a settembre della garanzia massima dell'80 per cento sulla dei mutui destinati alle categorie che hanno determinati requisiti di età e di reddito. Mi sono limitato a citare solo alcune delle tante disposizioni introdotte, che incideranno concretamente sulla vita dei nostri concittadini e per cui c'era l'urgenza; ecco perché era necessario adottare questo decreto. Il complesso normativo del decreto va in direzione di semplificare nella sostanza la vita degli italiani e consentirà di raggiungere gli obiettivi in tempi ragionevoli. Sono queste le ragioni del voto favorevole dei senatori di Forza Italia al disegno di legge di conversione in esame.

ho ascoltato prima per esempio la senatrice Spinelli, che ha avviato il suo intervento in discussione generale come se fosse l'*incipit* della relazione all'Aula. Questa maggioranza è da settembre che ci dice che è pronta a governare, che sono preparati, che dimostreranno di saper governare il Paese per i prossimi cinque anni; dopo circa otto mesi dall'inizio della legislatura, non riusciamo ancora a far capire che, quando un provvedimento va in Aula senza relatore, non c'è una relazione all'Aula. Quindi magari lo *staff* della senatrice avrebbe potuto quanto meno cambiarle le prime due righe del discorso, per avere un impatto diverso su chi lo va ad ascoltare successivamente. Ma l'imbarazzo non finisce neanche quando ho sentito l'intervento della senatrice Testor, che criticava per l'ennesima volta - figurati, quando mai! - il reddito di cittadinanza, parlando delle mancate politiche attive e quindi del mancato avvio al lavoro dei percettori. Si dimentica però di dire anche in questo caso la senatrice di maggioranza che il problema sono stati i centri per l'impiego, quei centri per l'impiego gestiti dalle Regioni a guida centrodestra. Non vorrei sembrare complottista se affermo che magari c'è stato un po' di ostruzionismo da parte delle Regioni. Ma figuriamoci! il problema secondo me non è di ostruzionismo, ma è di palese incapacità, perché a dicembre nella legge di bilancio questa maggioranza ha scritto che entro luglio bisognava togliere il reddito di cittadinanza ai cosiddetti occupabili, perché nel frattempo avrebbero fatto mesi (non ricordo bene quanti) di corsi professionali per avviarli al lavoro. Siamo a fine giugno e di questi corsi che dovevano avviare le vostre Regioni non c'è neanche l'ombra *(Applausi)*, perché i percettori perché i percettori di reddito di cittadinanza - se va bene - stanno venendo chiamati in questi giorni per sottoscrivere i patti per il lavoro, seppur siano titolari del reddito da un anno o più. Perlomeno, queste sono le notizie che ci arrivano. Quindi, il problema non è il reddito di cittadinanza. Il problema sono le Regioni: ce lo vogliamo dire una volta per tutte che l'apparato dello Stato che funziona peggio e crea più problemi sono le Regioni? L'insegnamento della pandemia non vi è bastato? *(Applausi)*. Che cosa dobbiamo fare? Ma sì, andiamo avanti sull'autonomia differenziata; siccome ci sono due o tre Regioni su diciannove, più due Province autonome, che magari funzionicchiano, mandiamo a scatafascio l'intero Paese. Bello, mi sembra un ottimo programma per il Paese. Veniamo a questo decreto-legge, l'ennesimo di quella maggioranza che non ha fatto altro che sbraitare dai banchi dell'opposizione negli ultimi cinque anni sull'eccesso di decretazione d'urgenza e l'eccesso di fiducie poste dai governi precedenti e in otto mesi ha superato già tutti i record. Complimenti ancora una volta. Sulla pubblica amministrazione, vi state sbizzarrendo: vi è questo decreto-legge enti pubblici, un decreto pubblica amministrazione 1, un decreto pubblica amministrazione 2, tutti esaminati alla Camera dei deputati, perché sia mai che rispettiamo tutte e due le Camere del Parlamento. Qui va bene che veniamo solo a ratificare; non so se vi sta comodo questo aspetto, fossi in voi un po' protesterei, almeno per un po' di sana alternanza, ma evidentemente i commissari della maggioranza che siedono nelle Commissioni deputate ad esaminare questi provvedimenti non vengono reputati all'altezza dal loro stesso Governo se finisce tutto alla Camera dei Deputati. Comunque, proroghe, proroghe e ancora proroghe, ma su INPS e INAIL commissariamo i presidenti, perché sono stati inefficienti e non hanno fatto bene il loro lavoro? Parliamo semplicemente dell'INPS, che mi viene più facile (immagino che capiate): nel 2022 hanno avuto un avanzo finanziario di 23 miliardi, un pessimo risultato effettivamente; risultato di esercizio dell'anno +7 miliardi. Vi Vi sembra una bocciatura per commissariare il presidente? Hanno effettuato negli ultimi anni una enorme modernizzazione dei servizi e la produttività è aumentata del 9 sono state un po' di assunzioni per riparare al mancato *turnover* degli anni precedenti con concorsi (12.000 assunti) e sono stati stabilizzati 3.000 precari dei *call center* che erano stati esternalizzati. La conoscete la parola esternalizzazione? L'abbiamo derivata da un grosso errore fatto dopo il 1992, perché l'apparato dello Stato era pesante e i pubblici dipendenti fannulloni e incapaci. Vi è una frase che risuona spesso: abbiamo esternalizzato per risparmiare ed efficientare. Dopo trent'anni ci rendiamo conto che non abbiamo risparmiato il becco di un quattrino, non abbiamo efficientato niente e i servizi faremmo meglio a reinternalizzarli, partendo dai *call center* dell'INPS e arrivando arrivando - si spera - ai medici gettonisti che lavorano un giorno in Piemonte, un giorno in Lombardia, un giorno in Sardegna e rendono i nostri pronto soccorso inefficaci. Tornando all'INPS, durante la pandemia hanno erogato 60 miliardi di sussidi e altre provvigioni per i cittadini e le imprese in difficoltà, aumentando di 16 milioni il bacino dell'utenza a cui erogavano prestazioni. Devo dire che sono effettivamente un sacco di risultati negativi che giustificano il commissariamento. Oppure, semplicemente, volevate dare un segnale e accaparrarvi subito, nella vostra bulimia di potere e poltrone, altre due poltrone? Diciamocela, la verità. Avete fatto la stessa cosa con l'AIFA. A novembre vi siete affrettati a fare degli emendamenti per cambiare la *governance* e le commissioni della nostra Agenzia del farmaco, salvo poi prorogare per ben due volte anche in questo provvedimento l'esistenza in vita delle due commissioni precedenti che volevate cancellare e unificare: avrebbero dovuto essere unificate

del nostro Paese. Anche quando dovreste trovare le risorse per aiutare le imprese che creano lavoro e che fanno fatturato, quelle del Nord che tanto bene riuscite a coinvolgere, alla fine è un nulla di fatto e andiamo avanti a proroghe. Perché non affrontiamo seriamente tutti insieme il problema del *payback* dei dispositivi medici? Non solo quello: perché non affrontiamo finalmente il problema dei tetti di spesa e dei *silos* nella nostra sanità e lo risolviamo una volta per tutte? il perché: perché ci vogliono un po' di soldi. Ma nella sanità mettiamo sempre le briciole e la stiamo definanziando di nuovo. Qualcuno ha il coraggio di dire in questa maggioranza che hanno messo ben due miliardi quest'anno per aumentare il Fondo sanitario nazionale? Capperi, complimenti! Ne servivano 20 per ripianare

contenta. Finalmente avete stabilizzato il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS e IZS: almeno qualcosa di buono, in mezzo a un mare di catastrofi, riuscite a combinarlo anche voi. Un grazie da parte loro. Ovviamente l'avevamo proposto decine di volte, quindi finalmente avete capito che era necessario farlo. Insomma, anche da questo decreto si vede che siete in ritardo su tutto. esempio. Avete deciso a dicembre nella legge di bilancio di nominare un commissario per il Parco della salute di Torino. Dopo quattro mesi circa, finalmente è uscito un nome, con tanto di conferenza stampa per la nomina. Siamo al 28 giugno ma del decreto di ma del decreto di nomina non c'è ancora nessuna traccia. Quindi abbiamo il commissario, ma cosa deve fare non si sa, o meglio lo sapete solo voi, forse. Sarebbe bello che ci fosse un po' più di trasparenza per tutti. Ma non Ma non eravate pronti? A noi non sembra proprio. Per questo, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

Sappiamo che arriva dalla Camera, dove c'è stato un contributo fattivo e molto importante anche da parte delle opposizioni. Molti emendamenti delle opposizioni sono stati accolti e anche molti emendamenti della maggioranza, in particolare della Lega. Tutti questi contributi hanno fatto sì che il testo avesse anche dei miglioramenti importanti. Questo provvedimento risponde alla necessità di un'azione di Governo rapida, efficace e concreta, che dia risposte a cittadini, famiglie e imprese. La necessità e l'urgenza sono giustificate? Certo. Sappiamo che al suo interno ci sono norme che avevano come scadenza quella del 30 giugno per il PNRR, ma sappiamo anche che usciamo da una pandemia e il Paese deve iniziare assolutamente a correre.

Nel tempo sicuramente si potrà fare fronte anche a un modo di governare che dia ancora più centralità al Parlamento e dare anche quelle risposte invocate dal Parlamento già da molti anni prima che arrivasse questo nuovo Governo. Venendo al decreto-legge al nostro esame, le materie trattate sono moltissime, le risposte date sono moltissime. Cito: affari sociali, ambiente, attività produttive, cultura, finanze, giustizia, lavoro e previdenza Regioni e affari regionali, trasporti ed altre disposizioni. disposizioni. Prendo alcune delle norme che ritengo più importanti, avendo poco tempo a disposizione. Inizio dalla conferma, che decorre dal primo luglio, della soppressione dell'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altri misure di contrasto alla pandemia.

per le singole Regioni e Province autonome di elevare, portandolo fino a mille invece che a 850, il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale: misura importantissima per poter dare una risposta ai territori. Modifica, ampliando l'ambito dei soggetti interessati, della disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari e di informazione specialistica, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario, ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria proroga, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, della sospensione delle attività del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. inoltre, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia (e arriviamo, appunto, al *cashback* di cui abbiamo già parlato). Si dispongono norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e presso istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutati a tempo determinato (è la stabilizzazione dei nostri cervelli, che è fondamentale per il nostro Paese). Il decreto prevede poi l'applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana, della lingua dei segni italiana tattile e anche delle lingue dei segni e delle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche, come ricordato dalla collega Testor. C'è un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026 per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, relativi all'allestimento del Villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo per i quali bisogna assolutamente partire. modifica del codice dei contratti pubblici, volta a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna. proroga di un anno del termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE. C'è la previsione di una serie di proroghe di termini riguardanti i contributi erogati per l'anno 2023 dal Ministero dell'interno a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza, scuole strade, edifici pubblici, efficientamento energetico. C'è la proroga della scadenza delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche riferite ad impianti per la produzione di energia elettrica. C'è il differimento del termine per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia che rientrano nel PNRR. La normativa è poi volta a consentire gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni. C'è tutta la parte, importantissima, per implementare gli alloggi per gli studenti universitari. Un'altra parte importantissima è il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento e all'acquisto di impianti sportivi. questo Fondo possa erogare finanziamenti - non più solo mutui - sotto qualsiasi forma, ivi inclusi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma; concedere anche finanziamenti a favore di enti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, alla aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali. Questo, per il mondo dello sport, è un provvedimento molto importante. Si riaprono inoltre i termini per aderire alla rottamazione *quater*, si incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e dunque di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazioni speciali disposte dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa viene prorogato e viene estesa la garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, quindi è un intervento importantissimo per i nostri giovani *under* 36, soprattutto per il fatto che la garanzia sia aumentata addirittura all'80 Si proroga la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali più colpite dal sisma del 2012 nella Regione Emilia-Romagna. differisce il termine di utilizzabilità del contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. alle numerose norme in materia di giustizia, viene sospesa fino al 31 dicembre 2023 - essendo avvocato, so che è una norma particolarmente importante importante - l'efficacia della norma che prevede l'obbligo per gli avvocati di effettuare con specifiche modalità le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo. Viene prorogata, tra l'altro, la sospensione dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale.

quando in quest'Aula discutevamo del primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, è arrivata la notizia che il Governo si era riunito per esaminare un secondo decreto e abbiamo sperato che si recuperassero le tante lacune e i tanti problemi non risolti dal

Nulla di tutto questo, purtroppo. Siamo chiamati a discutere in tutta fretta di un disegno di legge sugli enti pubblici che in realtà raccoglie, senza alcun filo conduttore, una serie di misure *omnibus* ed è proprio il caso di definirle così. Questo decreto-legge, che questa Assemblea ha il compito di convertire, nonostante sia stato presentato come un provvedimento riguardante gli enti previdenziali, contiene in realtà tutto un insieme di proroghe di termini senza che sussista alcun requisito di necessità e di urgenza, una forzatura che sembra rispondere più alle esigenze della maggioranza parlamentare che non al buon funzionamento di questi enti, un provvedimento che rischia di essere dannoso per i precedenti che si creano sui commissariamenti degli enti e confuso perché contiene linee di indirizzo in contraddizione tra di loro. Dobbiamo guardarci in faccia e usare parole di verità: il decreto-legge in esame nasce per venire incontro alla vostra esigenza di commissariare INPS e INAIL. Lo avete fatto adducendo formalmente la necessità di mutare le modalità di nomina del direttore e di ridurre da cinque a quattro anni il suo Per legge, come sapete bene, il commissariamento di un ente pubblico avviene per motivi di particolare urgenza che ne impediscono il corretto funzionamento, in questo caso non è così: avete inventato una motivazione che prova a indurre una sorta di *spoils system* che in Italia è vietato. Avete però fatto di peggio, perché prima avete deciso di azzerare le presidenze di INPS e INAIL in anticipo rispetto alla loro naturale scadenza, poi siete stati incapaci di nominare i nuovi vertici, rispettando i venti giorni di tempo che voi vi eravate dati, lasciando a lungo due istituti fondamentali con i presidenti ormai delegittimati nel loro ruolo e diminuiti nelle loro capacità operative e di intervento. Detto in altri termini, si sono voluti azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali sono l'INPS e l'INAIL, giustificando la misura con una non meglio specificata esigenza di razionalizzazione e semplificazione, solo che poi nel testo generate altra conclusione. All'articolo 1, infatti, il testo dispone che tra le funzioni del direttore vi sia la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.

un'evidente sovrapposizione, che produrrà uno stallo gestionale, altro che semplificazione. *(Applausi)*. Con un ordine del giorno presentato insieme alle colleghe Zampa, Camusso e Zambito, abbiamo contestato questa soluzione normativa, che rischia di ingessare il processo decisionale degli enti, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzare e semplificare. Il provvedimento in esame rappresenta il punto più basso a cui siete arrivati in pochi mesi. Scegliete di commissariare l'INPS, il più grande istituto pubblico previdenziale d'Europa, non sottoposto normativamente a *spoils system,* in una delicatissima fase nella quale si sta discutendo di di come spendere le risorse provenienti dal PNRR e di come rilanciare l'azione della pubblica amministrazione, anche dell'INAIL. Siamo davanti a un commissariamento politico: non si può definire in altro modo una scelta di parte, che dimostra la vostra volontà di mettere le mani ovunque (INAIL, INPS e RAI). Tuttavia, se volevate correggere la *governance,* perché non avete proposto alle parti sociali, perché non avete proposto ai veri azionisti dell'INPS e dell'INAIL, che sono i lavoratori e sono i datori di lavoro, di entrare nella *governance*? Quella sarebbe stata la riforma importante, partecipativa, che chiamava i veri azionisti a decidere che cosa l'ente deve mettere nelle sue priorità di azione.

l'introduzione di un tetto all'età dei sovrintendenti lirici, in modo da far dimettere (oppure, se preferite, da eliminare dal campo) il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Anche in questo caso, siamo fuori dalle norme, perché c'è una sentenza della Corte costituzionale a confermarlo. Oltre che fuori dalle norme, siamo in un contesto di incoerenza totale, perché poi contemporaneamente aumentate l'età di altri dirigenti e funzionari dello Stato nella sanità e in tanti altri ambiti, con nessuna coerenza. D'altronde, il Servizio studi del Senato ha messo nero su bianco queste perplessità, segnalando proprio il precedente cui facevo riferimento: già nel 2017 la Consulta aveva sancito che azzerare in anticipo gli incarichi viola i principi di buon andamento e imparzialità; è un precedente che non lascia spazio ad alcun dubbio. Cara Presidente, non possiamo evitare di dire le cose come stanno. Non solo si stanno occupando tutti gli spazi in un modo poco democratico penso, ad esempio, a quanto sta succedendo in RAI - ma si fanno fuori dirigenti pubblici prima della fine del mandato con norme *contra personam*. Le esigenze della politica vengono prima dell'ordinamento e del buon funzionamento degli enti pubblici? È inaccettabile. Mi chiedo per chi siano urgenti le disposizioni urgenti cui fate riferimento nel nome del decreto: lo sono forse per lo Stato, per il buon governo degli enti pubblici oppure per la maggioranza che governa il Paese? La risposta è semplice da dare, purtroppo.

devono essere fissati e temporalmente collocati l'aggiornamento e l'aggiudicazione degli interventi da realizzare sugli edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. Siamo

perché diventata ormai senza governo e senza progettualità e non è più in grado di svolgere il suo ruolo, così delicato e importante per la salute dei cittadini.

dei carichi affidati all'agente di riscossione fino al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-*quater*, che era contenuta nella legge di bilancio 2023 e che viene in tal modo rinviata per la seconda volta, comportando lo slittamento delle relative entrate. Sarebbero tanti i casi da citare. Non avete mai tenuto conto dei nostri emendamenti e non abbiamo avuto tempo nemmeno di discutere. È per questo che il nostro voto sarà convintamente contrario.

Anche noi, come voi, abbiamo avuto poco tempo per leggere le norme, che sono tante. Parliamo di un provvedimento che si compone di 14 articoli, che trattano varie questioni e sottopongono alla nostra approvazione diverse misure. Anche noi abbiamo avuto poco tempo, però abbiamo letto il provvedimento, abbiamo cercato di entrare nel merito e di fare le nostre valutazioni. Il provvedimento che ci apprestiamo a convertire in legge reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale ed è stato emendato dalla Camera dei deputati, con modifiche anche sostanziali. Su questo voglio fare un inciso, ho sentito alcune considerazioni che miravano a contestare la velocità con la quale la maggioranza si appresta ad approvare il provvedimento. In effetti, non ci siamo mai sottratti al al dialogo parlamentare, né in Commissione, né in Aula, e non lo faremo neanche oggi. Se però aveste letto bene il provvedimento, avreste anche letto che ci sono alcuni termini che scadono il 30 giugno

tra le varie misure adottate, intervenendo sulla missione 4 del PNRR, differisce dal 31 maggio al 30 giugno il termine ultimo entro cui dev'essere fissata e temporalmente collocata l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per servizi alla famiglia. Questo è un termine fondamentale. Lo dico da sindaco di un piccolo Comune, che ha ricevuto 1,2

di un provvedimento - lo dirò in maniera sintetica - che agisce anche sulla sanità. Intanto agisce sulla sanità dei nostri amici calabresi, commissariata da tanti anni, anni, prevedendo un'ulteriore estensione delle misure in suo sostegno fino al 31 dicembre 2023 e disponendo inoltre che il personale tecnico-operativo fornito dall'Agenas possa essere prorogato, con riferimento ai contratti di lavoro flessibile risultanti in servizio. È prevista la decadenza dei commissari straordinari nominati, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. un breve inciso, concordando in parte con quello che ha detto il senatore Lombardo, per il tramite della Presidenza, perché anche io vengo da una Regione che, insieme alla Calabria, è commissariata dal punto di vista sanitario. Anche io ho visto i danni del commissariamento sanitario e sono d'accordo sul fatto che la politica debba mettere rimedio a questa situazione. C'è stata una sentenza della Corte costituzionale di qualche mese fa, del febbraio 2023, che, bocciando una norma della Regione Molise in tema di sanità, ha però fatto un inciso, che non gli era dovuto, e ha detto che, se una Regione è commissariata da quattordici anni e il commissariamento non produce effetti positivi, evidentemente c'è qualcosa che non va in quella procedura. La politica deve dunque prendere spunto da questo principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale e porre rimedio ai problemi che derivano dal commissariamento sanitario. La sanità deve tornare in mano alla politica, a una politica e a dirigenti ovviamente responsabili, non può essere lasciata ai freddi numeri, perché si tratta della vita delle persone *(Applausi)*. Si stabiliscono inoltre misure economicamente compensative per i sub-commissari delle Regioni in disavanzo, nonché la soppressione, a decorrere dal 1o luglio 2023, delle unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima. Particolare rilievo assume poi l'articolo 3, al comma 5-*bis*, che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario, ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. Non meno importanti appaiono le previsioni legislative del comma 5-*ter* dell'articolo 3, che proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023, delle singole Regioni o Province autonome, di elevare da 850 a 1.000 il numero massimo di assistiti a carico dei medici di medicina generale, aventi anche un incarico ad attività oraria di ventiquattr'ore settimanali. Il comma 6 dispone la proroga, fino al 30 giugno 2024, della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pari a 100 euro) prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid.

che modifica l'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, un'apposita insegna metallica con relativo diploma *(Applausi)*

intervenendo sul credito d'imposta a loro favore. Si tratta quindi di un provvedimento utile; ripeto che, se lo aveste letto perbene, probabilmente oggi lo avreste approvato insieme a noi.

Ci avete definito come quelli che affamano la loro gente, che non riesce neanche a pagare le bollette. Dimenticate spesso però, anche in quest'Aula, che per dieci anni avete governato voi questo Paese, che, se oggi è alla fame, è per colpa vostra. *(Applausi)*. Questo Governo da pochi mesi a questa parte ha dato importanti risorse per famiglie e imprese, proprio per contrastare la crisi energetica. Ci avete accusato di aver dato solo due miliardi per la sanità pubblica (ma già è un dato confermare che abbiamo dato questi due miliardi), quando ne servirebbero 20 e quando voi avete distratto risorse importanti (centinaia di milioni di euro) per l'acquisto di mascherine fasulle, banchi a rotelle e monopattini.

un'istanza non solo carente di ogni presupposto giuridico, ma che dimostra ancora una volta il fatto che voi siete contro l'Italia e gli italiani (i quali però se lo ricordano e ogni volta che vanno in cabina elettorale ve lo dimostrano)?

Non ci limiteremo però a trattarvi come voi trattate noi, che siamo avulsi dalla cattiveria e dall'astio. Vorrei concludere dicendovi che non tratteremo la cattiveria come un vento gelido

nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 774, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Ciascun senatore Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. senatrice Pirovano).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pirovano.

Onorevoli colleghi, su richiesta e intesa unanime dei Presidenti di Gruppo, *nemine contradicente*, come si suol dire, l'ordine del giorno è integrato con la discussione immediata di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

primo comma, della Costituzione, nell'ambito di una procedura di mediazione civile e di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti***

2021 presso l'organismo di mediazione civile ExAequo a.d.r. di Potenza, e per il quale è altresì pendente un procedimento penale dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Giarrusso, che è parte di un procedimento civile e di un procedimento penale per gli stessi fatti, che naturalmente la Giunta ha la Giunta ha trattato congiuntamente. Si tratta sostanzialmente di dichiarazioni rilasciate dall'ex senatore in un'intervista che è stata rilasciata il 27 maggio

- e altre accuse ancora più gravi di una potenziale trattativa Stato-mafia della quale il dottor Basentini sarebbe stato protagonista, addirittura con incontri con pregiudicati e condannati per reati gravissimi in prigione, al fine di risolvere turbolenze che si stavano verificando negli istituti penitenziari. colleghi e colleghe, non è però il tenore delle dichiarazioni dell'ex senatore Giarrusso, ma è comprendere se quelle dichiarazioni possono essere considerate opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, cioè se nel formulare le accuse che il senatore di Giarrusso formulò in quell'intervista stesse in realtà esercitando il suo mandato parlamentare. Questa è la valutazione che la Giunta ha fatto all'unanimità, sulla base in particolare di un atto di sindacato ispettivo di identico contenuto, con il quale il senatore Giarrusso interrogava l'allora ministro della giustizia, utilizzando praticamente le stesse parole che aveva poi condiviso con il giornalista e che erano state rese pubbliche. Ora, a strettissimo rigore di logica, si cerca sempre di avere una coincidenza di tempi

del 27 e del 28 maggio 2020, i giorni erano esattamente gli stessi. Andare a ricostruire se l'interrogazione sia stata depositata il 27 o il 28, è veramente questione di ore; potrebbe essere stata consegnata il 27 e poi protocollata il 28, ma di fatto, a nostro avviso, si ha una sostanziale coincidenza di tempi. di tempi. Io non starei neanche a usare il bilancino del farmacista, nel senso che se un parlamentare si è occupato di una certa materia, lo ha fatto storicamente nella sua attività e in in quel periodo si stava esattamente occupando di quello. Si può essere d'accordo o no con le cose che ha detto, ma è fuori discussione che stava esprimendo delle opinioni, seppur opinabili, discutibili e censurabili e seppure possano aver ferito l'oggetto di quell'intervista. È fuori discussione che quando i nostri Costituenti hanno stabilito Grazie a tutti l'insindacabilità di quelle espressioni ed è per questo che, in qualità di relatore, chiedo a questa Assemblea di votare conformemente alle decisioni della Giunta.

nel quale le opinioni espresse fuori dall'Aula sono state riversate anche in atti tipici

è un caso classico nel quale noi riteniamo assolutamente applicabili le prerogative di cui all'articolo 68. Voteremo pertanto coerentemente con quello che abbiamo fatto in sede simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale l'ex senatore Mario Michele Giarrusso ha ricevuto l'istanza di mediazione presentata in data 19 febbraio 2021 presso l'organismo di mediazione civile ExAequo a.d.r. di Potenza, e per il quale è altresì pendente un procedimento penale dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Pacifico,

per il punto di fatto, in particolare la domanda dell'autorità giudiziaria riguarda la possibilità di acquisire i *file* di *log* relativi al profilo Instagram e all'*account* di posta elettronica dell'onorevole Pacifico, che sono stati oggetto di indebito accesso, ed è quindi rivolta al fine di identificare l'autore dei reati descritti in danno della stessa ex senatrice. Nella seduta del 14 febbraio 2023, in cui è stata esaminata la richiesta in discorso, la relatrice evidenziava che la stessa era stata formulata ai sensi della legge del 20 giugno n. 140, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione e, come più volte ricordato dalla stessa giurisprudenza costituzionale e dalla Corte di cassazione, anche laddove il parlamentare si configuri come persona offesa del reato è necessario in ogni caso l'autorizzazione della Camera di appartenenza dello stesso, non essendo tali prerogative rinunciabili da parte dell'interessato. La relatrice inoltre aggiungeva che ai fini istruttori si reputasse opportuno acquisire l'avviso dell'ex senatrice Pacifico rispetto alla richiesta dell'autorità giudiziaria di accedere ai propri dati di *account* e del profilo personale, in considerazione appunto del fatto che la stessa ex senatrice è in tal caso vittima stessa del reato e non presunta autrice di reati come avviene ordinariamente, e tuttavia avrebbe potuto avere riserve rispetto all'accesso ai propri dati informatici. L'acquisizione dell'opinione dell'interessata sarebbe stata anche finalizzata ad escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* a suo danno, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere. Quindi, la relatrice proponeva di fissare un breve termine all'interessata, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, per presentare le proprie memorie scritte o eventualmente per chiedere di essere audita. La Giunta conveniva sulla proposta e, con nota del 21 febbraio, l'interessata ha manifestato il consenso all'accesso ai propri dati informatici a tutela della sua persona e delle istituzioni rappresentate, invitando quindi la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere. Nella successiva seduta del 28 febbraio 2023 la Giunta prendeva atto della citata nota e approvava la proposta della relatrice di concedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Per il punto di diritto, come evidenziato in punto di fatto i Presidenti delle Camere e della giurisprudenza evidenziano che, anche laddove il parlamentare sia persona offesa del reato, il procedimento previsto dal Regolamento di ciascuna Camera innanzi alla rispettiva Giunta e all'Assemblea deve essere comunque esperito a tutela della persona del parlamentare e delle prerogative del Parlamento. In particolare, nel caso specifico, deve potersi escludere ogni possibilità

Quindi, eravamo al punto di diritto. In particolare, nel caso specifico, deve potersi escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* in danno dell'ex senatrice. Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole alla relazione del Gruppo Partito Democratico, per la ragione evidente, che è emersa anche dalla relazione, che si tratta di una richiesta di autorizzazione che viene dalla stessa senatrice Pacifico, in qualità di persona offesa in un procedimento in cui c'è stata una illegittima intromissione nei propri dati personali. Quindi, evidentemente non si poteva che accogliere la richiesta. scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione)*.

di cui agli articoli 81 e 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale per aver offeso la reputazione di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, con riferimento alla missione con soccorso in mare di 53 persone nella cosiddetta zona SAR libica del 12 giugno 2019. In particolare, il senatore Salvini è accusato di aver proferito nei confronti di Carola Rackete, tra il 15 giugno e il 19 luglio 2019, diverse frasi offensive il cui contenuto integrale è riportato nella relazione già depositata, a cui si rinvia, in dirette o *post* su Facebook e Twitter, nonché nel corso di un'intervista durante la trasmissione televisiva «Fuori dal coro». In punto di diritto, va osservato che la giurisprudenza costante della Consulta - vedi tra tutte le sentenze del Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011 ritiene che le dichiarazioni rese *extramoenia*, cioè in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio, da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le dichiarazioni espresse all'esterno delle Aule parlamentari o quelle pronunciate all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica fra i due atti (cioè *extramoenia* o *intramoenia*) essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale. secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima. La corrispondenza contenutistica fra dichiarazioni *extra moenia* e quelle *intra moenia*, nonché il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna appare sussistente nel caso di specie. Per alcune delle attività *intra moenia* tale corrispondenza è testuale e contemporanea. Sul punto si rinvia, per i dettagli, alla relazione depositata. In conclusione, la Giunta propone quindi all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

del Governo e del Parlamento, perché l'articolo 68 della Costituzione dice che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il tema, però, si pone quando un parlamentare sia anche membro del Governo, perché la Costituzione non prevede per i membri del Governo una simile guarentigia e quindi il tema che ci troviamo ad affrontare in questo caso è: nel momento in cu il ministro dell'interno Salvini fa delle dichiarazioni che sono considerate diffamatorie da una terza persona, è coperto in quanto parlamentare o sta esercitando la sua funzione di Ministro per il quale questa copertura non è prevista, ma è previsto eventualmente che ci siano i reati ministeriali e il tribunale dei Ministri? Ministri? Dato che questo interrogativo non viene risolto, noi preferiamo astenerci, in quanto a nostro avviso in questo caso il ministro Salvini parlava come Ministro e sicuramente non come parlamentare. La dimostrazione - ce ne sono due - è che vengono indicati alcuni atti *intra moenia,* cioè alcune dichiarazioni fatte in Aula prima del 19 marzo e poi successivamente. Nel primo caso si dice che il ministro Salvini si alza e va a parlare dal suo scranno di senatore per specificare che sta parlando come senatore. Al di là del fatto che secondo me la qualità di Ministro non cambia se ci si siede da una parte o dall'altra, o dall'altra, nel momento in cui si è titolari delle politiche nazionali sui temi che riguardano il Ministero dell'interno, ovunque ci si siede si è Ministro, tant'è che il ministro Salvini, pur seduto nel suo scranno di senatore affermava, come leggiamo dal Resoconto stenografico: «Desidero confermare a quest'Aula, in conclusione, che il Governo di cui mi onoro di essere Vice Presidente e Ministro dell'interno ha sviluppato, eccetera..». Lui stesso, pertanto, si accorge che, nonostante si sia seduto da un'altra parte, evidentemente era ancora Ministro dell'interno.

fare interrogazioni parlamentari, perché il Governo non può interrogare sé stesso. Ricordo che i membri del Governo non possono nemmeno presentare disegni di legge, perché il Governo è un organo collegiale e quando il Governo vuole presentare un disegno di legge, deve farlo collegialmente. Pertanto il relatore afferma che il ministro Salvini non poteva presentare l'interrogazione, ma poteva rispondere all'interrogazione e questo sarebbe l'atto *intra moenia* che egli svolse come parlamentare. tutti noi e in particolare chi ha avuto incarichi di Governo, sappiamo benissimo che la risposta alle interrogazioni parlamentari è l'atto di Governo *par excellence,* nel senso che viene scritto dagli uffici del Governo, viene stampato sulla carta intestata del Governo e quindi è sicuramente un atto del Governo. Io credo che in questo caso, parlando strettamente, dobbiamo riconoscere che in quel momento il ministro Salvini stava intervenendo come Ministro dell'interno, cioè se avesse parlato di agricoltura o di salute e di sanità, probabilmente avremmo potuto dire che stava facendo facendo politica, nel senso che stava facendo politica generale in quanto parlamentare. Tuttavia, nel momento in cui le sue dichiarazioni sono strettamente sono strettamente connesse alla responsabilità di Ministro dell'interno, dobbiamo considerare che quelle sono le dichiarazioni di un qualsiasi Ministro, altrimenti dovremmo considerare due categorie di membri di Governo: quelli che possono dire qualsiasi cosa perché sono coperti dall'articolo 68 della Costituzione e quelli che, non essendo parlamentari, invece rischiano il reato ministeriale in quanto non parlamentari. Io credo che questo sia un elemento sul quale la Giunta dovrà riflettere. Desidererei inoltre che il voto odierno non fosse considerato un precedente, perché credo che dal punto di vista tecnico-giuridico il problema resti aperto e meriti una definizione. Non so se più avanti nel tempo capiteranno sentenze della Corte costituzionale su questo argomento, ma di certo, stanti così stanti così le cose, noi riteniamo che non sia possibile prendere una posizione definitiva e pertanto il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEuropeper questi motivi si asterrà.

essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese *extra moenia,* soltanto quando queste presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette interne. Questo è il ragionamento seguito dalla Cassazione con la sentenza n. 32862 del 2019; ci sono poi i precedenti conformi del 2010 del 2014. Vengono fatte rientrare altresì nell'alveo delle immunità anche le dichiarazioni rese in forma o in sede non tipica, ma che siano da ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare. Non è a tal fine sufficiente, né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate. Alla base del ragionamento tecnico - preciso, tecnico e non politico - da parte della Corte ci sono due elementi: innanzitutto, il legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; in secondo luogo, la corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e degli atti esterni al di là delle forme letterali usate. Il legame temporale non sembra sussistere. Infatti, gli atti richiamati dalla relazione conclusiva della Giunta rispetto a quelli per i quali il senatore Salvini è chiamato a rispondere di diffamazione aggravata, datati 15 giugno 2019, non sembrano suscettibili di assorbimento rispetto alle Si fa riferimento a due diversi atti *intra moenia*. Il primo, svoltosi il 20 marzo 2019, è riconducibile alla discussione del documento inerente alla questione della nave Diciotti. Si tratta di un tema che solo in via generale e astratta può essere sussunto a quello relativo al caso di specie. Infatti, a ogni buon conto, non potrebbe assicurare la guarentigia dell'insindacabilità a un atto *intra moenia* che, pur avendo ad oggetto il macro-tema del contrasto alle questioni dei flussi irregolari e del *business* del traffico degli esseri umani nel Mediterraneo, non abbia requisiti ulteriori rispetto alla semplice comunanza di argomento. Il *post* diffamatorio pubblicato sembrerebbe scoperto dei requisiti, in ragione del fatto che trattasi solo di uno sconnesso elenco di insulti resi dal senatore Salvini nei confronti della comandante della Sea Watch 3 quali: criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca. Sono insulti sicuramente estranei rispetto alla citata finalità divulgativa necessaria ai fini dell'applicabilità della guarentigia. Il secondo atto *intra moenia*, citato nella relazione conclusiva e datato 14 giugno 2019, ha del surreale. Si fa riferimento a un decreto-legge in quanto - e cito testualmente «viene presentato in Parlamento per la conversione e conseguentemente non può non rilevare come atto parlamentare». Se tale assunto rispondesse al vero, ciascun parlamentare avrebbe potuto beatamente diffamare la comandante della nave senza nessun timore di ipotetici procedimenti, perché ricadente nell'ipotesi di insindacabilità delle opinioni espresse espresse esclusivamente per avere partecipato al procedimento di conversione di un decreto-legge in materia. Per me è assurdo. La relazione conclusiva fa riferimento anche all'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, nella specie del diritto di critica politica. Sul punto occorre segnalare che il diritto di critica assurge a causa di giustificazione all'avverarsi di determinate circostanze: innanzitutto, ove siano rispettati i limiti di veridicità dei fatti narrati, nonché della pertinenza, ossia dell'oggettivo interesse dei fatti per l'opinione pubblica, nonché della correttezza formale - cosiddetta continenza - che nella competizione politica è caratterizzata da maggior elasticità in ragione dei toni aspri ed elevati che contraddistinguono tale ambito. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, pur potendo sopportare toni duri e di disapprovazione, la condotta non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto di altri all'integrità morale. Infatti, se non si rispettano tali limiti, la competizione politica diventa solo un'occasione per aggredire la reputazione altrui. Concludo, signor Presidente. Le dichiarazioni espresse dal senatore Salvini non sembrerebbero ricadere nell'ipotesi di cui l'articolo 68, comma primo, della Costituzione per i motivi esposti in premessa. Il voto favorevole alla richiesta di insindacabilità creerebbe un precedente difficilmente giustificabile, essendo le affermazioni del senatore Salvini configurabili esclusivamente come attacco personale. Qualsiasi valutazione che esuli rispetto ad un voto contrario si porrebbe in distonia con la consolidata giurisprudenza sul tema. Per queste ragioni dichiaro il voto contrario alla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

come ho detto e come abbiamo avuto modo di dire in Giunta, apprezziamo lo sforzo del relatore di trovare degli appigli giuridici per giustificare la richiesta di insindacabilità del senatore Salvini. Tuttavia, c'è parso di sentire il classico rumore delle dita sugli specchi, di chi si arrampica sui vetri, per cercare di giustificare l'ingiustificabile. Vorrei ricordare all'Assemblea di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una querela che è stata presentata da una cittadina tedesca, Carola Rackete, nei confronti del senatore Salvini, per le seguenti frasi, che cito: «Chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati» (26 giugno 2019). «Nel mezzo, la decisione del giudice sulla conferma o la revoca degli arresti per la criminale tedesca» (1° luglio 2019). «Nessun problema: per la comandante criminale (...) è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese» (2 luglio 2019). «Sono semplicemente incazzato per una sentenza che libera una delinquente» (3 luglio 2019). «Questa ricca tedesca fuorilegge...la liberazione di una criminale, che in questo momento è libera di mangiarsi spaghetti aglio, olio e peperoncino e di andare in giro per l'Italia, magari tornando a provare a delinquere». «La ricca e viziata fuorilegge tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino». «La capitana è una fuorilegge». «Quella povera donna, che ha solo provato ad ammazzare cinque militari italiani». «Questi non sono soccorritori, questi sono complici, questi sono potenziali assassini. Questi sono criminali» (3 luglio 2019). «Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini, non con le delinquenti» (3 luglio 2019). «La nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i finanzieri italiani... Una nave di pirati» «Non è colpa della comandante fuorilegge». (4 luglio 2019). «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca». (5 luglio 2019). i colleghi a non interrompere e a non commentare: è una dichiarazione di voto e ognuno esprime la propria opinione. In questi casi, la calma è sempre più utile. Prego, prosegua senatore Bazoli. è curioso che si discuta senza neanche sapere di cosa stiamo discutendo. Quindi, cito esattamente le parole *(Applausi)*. «Carola, voglio dire, uno basta che la guardi in faccia». «Pure Carola mi ha denunciato. Cioè, tra le tante denunce, pure la zecca tedesca mi ha denunciato» (18 luglio 2019). «Non vedo l'ora di espellere questa viziata comunista tedesca!». «Hanno rischiato la vita per colpa della comandante criminale». (19 luglio 2019) Quindi, stiamo parlando di un Ministro della Repubblica che ha detto a una cittadina tedesca cinque volte «criminale», quattro volte «fuorilegge», due volte «viziata comunista tedesca», due volte «delinquente», una volta «sbruffoncella», una volta «zecca tedesca», una volta «povera donna», in un mese e mezzo. di un mese e mezzo che è stata addotta dal relatore per giustificare la richiesta di insindacabilità è che il Ministro era insieme Ministro e senatore, perché sappiamo che i Ministri non sono coperti dalla guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione, ma hanno un altro percorso, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, che tutela i Ministri. I Ministri, di per sé, non sono tutelati dall'articolo 68 della Costituzione, che riguarda solo i parlamentari e la difesa della libertà del Parlamento, non riguarda i Ministri. Quindi, si è cercato di dire che in realtà, quando interveniva in il ministro Salvini interveniva non come Ministro, ma come parlamentare, anche qui arrampicandosi sugli specchi. Sostiene il senatore Scalfarotto che questa è una questione tecnica su cui bisogna avere chiarezza. Voglio fare chiarezza, citando le parole di una sentenza della Corte costituzionale del 2007. Le cito, perché forse sono più chiare di come potrei essere chiaro io: «La coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di Ministro non giustifica in alcun modo l'applicazione estensiva al Ministro della garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proprio del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo». Quindi non è applicabile l'articolo 68 *(Applausi)*, perché il ministro Salvini in quest'Aula interveniva in qualità di Ministro, non di parlamentare.

stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che ora vi leggo, così ce lo ricordiamo tutti *(Commenti)*: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

ce lo dice la Corte costituzionale, se non ci arriviamo noi con il buon senso. La Corte costituzionale ci dice che la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. parlamentari. Perché non possono essere ricompresi gli insulti? Perché giustamente i Regolamenti parlamentari stessi negano l'ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti, quindi *a fortiori* - dice la Corte - le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse. In ogni caso, anche a fregarsene delle risultanze della Corte costituzionale sul fatto che l'articolo 68 non può essere applicato ai Ministri, non potremmo giustificare le le espressioni utilizzate dal ministro Salvini, perché non si tratta di opinioni, ma si tratta di insulti, tra l'altro pronunciati nell'arco di un mese e mezzo, cosa che non era mai capitata.

Non è mai capitato; sono episodi singoli di solito. Non possiamo ora introdurre un precedente in base al quale basta depositare un atto in quest'Aula per essere per essere autorizzati a insultare per due mesi una persona. È assurdo, è illogico, è inconcepibile, è inaccettabile.

La Giunta si è attenuta, in merito alla questione dell'applicabilità dell'articolo 68 ai Ministri parlamentari e ai Ministri non parlamentari, ai suoi precedenti. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in merito al senatore Candiani, nella XVIII legislatura, documento 4-*ter*, n. 7-A, proposto al voto dell'Assemblea il 19 maggio 2021, e anche la Giunta per le autorizzazioni

secondo me, tra la posizione di un ministro parlamentare e non parlamentare è ragionevole, atteso che lo *status* di parlamentare non cessa con il conferimento dell'incarico di governo. *(Applausi)*. mi preme sottolinearlo perché è un aspetto tecnico, si ribadisce che, nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo 2019 il senatore Salvini, spostandosi sullo scranno di senatore, come appunto precisato espressamente dal Resoconto stenografico d'Assemblea, quindi intervenendo in qualità di parlamentare e non di Ministro, si soffermava sul profilo inerente all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani che tale fenomeno alimentava. Ricordo anche che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non è richiesta una corrispondenza letterale, ma contenutistica delle dichiarazioni. Se vogliamo discutere di frasi sicuramente che teoricamente possono costituire un reato di diffamazione o costituiscono reato di diffamazione, allora dobbiamo discutere dell'applicazione o dell'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione. Dobbiamo fare un disegno di legge costituzionale in cui abroghiamo l'articolo 68 della Costituzione, se siamo del parere che frasi offensive, che in teoria possono costituire anche reato di diffamazione, debbano essere perseguite. Ricordo che anche il Partito Democratico, in votazioni precedenti, anche di fronte a delle dichiarazioni pesanti, ha votato a favore di un'immunità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, mentre devo riconoscere la linearità del MoVimento 5 Stelle sulla questione, anche di fronte a propri colleghi senatori in quest'Aula. Quindi, volevo tecnicamente rispondere e confermo la relazione già depositata agli atti.

simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione)*.

di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

che dichiarava, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, di non doversi procedere nei confronti della senatrice Barbara Lezzi. Il giudice di pace dichiarò infatti l'improcedibilità dell'azione, affermando di doversi applicare il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, posto che tali espressioni erano state proferite dalla senatrice Lezzi in un discorso pubblico inerente al suo ufficio di parlamentare. a tale pronuncia venivano presentati dei ricorsi e con sentenza n. 309 da parte della Corte di cassazione nel gennaio 2021, dopo aver respinto la censura proposta dalla parte civile sulla tardività dell'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata, si riteneva che nella sentenza impugnata mancasse la verifica - da parte del giudice - della sussistenza del nesso fra la funzione di parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia* dalla senatrice. Quindi, in punto di diritto, si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare basato sulla corrispondenza

quando si parla davanti a un gruppo di persone del proprio partito, di fatto si sta svolgendo un'attività che è quella politica dei partiti e che in Parlamento diventa quella del Gruppo parlamentare. Lo dico perché, secondo me, bisogna bisogna rifuggire da interpretazioni meccanicistiche per le quali se non c'è proprio la parola scritta esatta negli atti parlamentari non si possa invocare l'articolo 68. Credo che l'articolo 68 sia stato scritto dai nostri Padri costituenti costituenti con un preciso obiettivo in mente, che era quello di fare in modo che i parlamentari potessero liberamente fare politica, quindi potessero esprimersi senza il timore di essere perseguiti per le proprie opinioni. Ed è ovvio che, nel caso della senatrice Lezzi, quelle opinioni espresse davanti a un gruppo di militanti erano certamente delle opinioni politiche e, come tali, necessitavano di essere

del Parlamento, perché non dimentichiamo che le guarentigie dei parlamentari non sono date *ad personam* per creare una casta di privilegiati, come qualcuno potrebbe pensare anche in quest'Aula, ma servono a garantire la libertà di tutta l'Assemblea. Quindi dobbiamo avere sempre un atteggiamento estensivo rispetto all'articolo 68 e non dobbiamo entrare in una sorta di bilancino del farmacista che ci dice che questa parola va bene e quell'altra non va bene. Ovviamente, se uno parla di qualcosa che non ha nulla a che fare con la sua storia politica e con la sua attività politica, è evidente che non può essere coperta. Se ci fosse, però, un parlamentare che ha un modo di esprimersi un po' colorito - e non è che non ce ne siano ne siano - noi dovremmo fare in modo di ricordare che nessuno può utilizzare questo strumento per limitare la libertà del Parlamento. Io provengo da una cultura garantista e questo mi sento di dire. I colleghi del Partito Democratico potranno anche essere ma questo è il modo con il quale noi interpretiamo l'articolo 68 e questo è il modo nel quale in questa legislatura voteremo quando si presenteranno casi di questo genere.

la reputiamo un'accusa molto grave. A noi fa ancora un certo effetto essere o non essere delinquenti. *(Applausi)*. Detto questo, questo è il classico caso in non si tratta di applicare in modo meccanicistico la norma oppure no. Si tratta di applicare le norme, le sentenze della Corte costituzionale che diventano norma, ma soprattutto applicare la Costituzione. infatti, non bisogna avere un approccio ideologico - e devo dire che nella giurisprudenza della Giunta, purtroppo, è sempre molto più raro trovare un approccio non di parte o non ideologico e di questo mi dolgo, perché ciò umilia le funzioni del Parlamento e l'autonomia della Giunta però l'ideale della Costituzione. L'articolo 68 infatti, è nato all'indomani dell'uscita da un regime autoritario, in cui il Parlamento era stato umiliato, la libertà dei parlamentari non era solo minacciata, ma addirittura a costo della vita, e dove l'autorità giudiziaria era completamente sottomessa all'Esecutivo. Di questo stiamo parlando

molto pacificati rispetto al fatto che si tutela la libertà del parlamentare. Diverso è quando sul piatto della bilancia c'è la tutela di un diritto. A proposito di garantismo, dico con affetto al senatore Scalfarotto che il garantismo nasce a tutela dei più deboli, non dei più forti *(Applausi).* Il garantismo è la tutela dei deboli, perché, quando sei in un processo penale, sei la parte debole, nei confronti sicuramente dello Stato (tant'è vero che, quando guardiamo oltreoceano, l'accezione è sempre: lo Stato contro), ma anche se si chiede la tutela di un diritto. Perché noi dobbiamo richiamarci alla Costituzione? Perché Perché nella Costituzione c'è una continua ricerca di equilibrio tra le libertà individuali e il potere. È chiaro È chiaro che in questa legislatura ci troveremo molto spesso a discutere di che cos'è questo equilibrio e come interpretiamo il potere, perché è evidente che non la pensiamo allo stesso modo. è evidente che non la pensiamo allo stesso modo. Il caso di cui abbiamo trattato prima lo dimostra. L'autonomia della politica, che noi rivendichiamo, la nobile autonomia della politica, non è esercizio indiscriminato di un potere a discapito della tutela dei singoli cittadini, non è il potere per il potere, non è il fine che giustifica i mezzi. La politica è uno strumento, è l'esercizio del potere in senso virtuoso, ma, attenzione, noi non faremo un solo passo indietro sulla questione dell'autonomia della politica, che rivendichiamo. Attenzione, però, a non confonderla con qualcos'altro, perché la separazione tra i poteri, i poteri di controllo, l'autonomia delle autorità indipendenti nascono esattamente da questo, a tutela del Parlamento. Distinguere il Parlamento dall'Esecutivo è l'ABC

o di là. Capiamo come farle funzionare meglio, ma spingere continuamente perché ci sia un potere senza controllo, a discapito dei diritti dei cittadini, è fuori dalla Costituzione.

proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023: sulla

luogo, partendo dalla riforma del Patto di stabilità e crescita, siamo tutti d'accordo sulla necessità di una sua revisione mirata, dato che oggi è sospeso, ma esso non può, nel 2024, tornare a essere solo di stabilità e non di crescita. e non di crescita. Abbiamo bisogno di una politica europea industriale, visionaria e futuristica, con una sua autonomia strategica e un suo potenziale indipendente dalle altre potenze globali. ci stiamo impegnando nell'attuazione del PNRR e delle reti TEN, con i fondi strutturali e con gli investimenti legati al clima e nella difesa comune europea. Servono percorsi credibili e sostenibili, per diminuire il debito e controllare la spesa, e dev'essere concesso un uso flessibile dei fondi europei per per la crescita economica e lo sviluppo industriale, specialmente per le piccole e medie imprese, che coprono il 99 per cento del tessuto industriale europeo, non solo italiano. Si è deciso che gli investimenti nel clima, nel digitale, nel PNRR e nella sanità europea qualificano l'Europa del XXI secolo rispetto agli altri attori dello scenario globale, quindi dobbiamo essere conseguenti anche nel valutarli sul piano della disciplina fiscale, che dev'essere comune e non avere *dumping* fiscali e concorrenza nello stesso mercato europeo. secondo luogo, vorrei dunque parlare del mercato interno, creato nel 1993, con l'idea di armonizzare le legislazioni nazionali, per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale e non per farci concorrenza tra noi, con il *dumping* fiscale e salariale, come avviene in questo momento. Gli oneri delle direttive europee, specialmente del Fit for 55, che vanno a gravare sulle nostre aziende, sulle nostre famiglie e sulle nostre amministrazioni pubbliche, devono essere ridotti al minimo e dobbiamo vigilare sul loro rispetto. Lo stesso vale anche sulle politiche europee, specialmente quelle di contrasto all'inflazione. L'aumento continuo degli interessi dei mutui sicuramente non fa bene all'economia, alle famiglie e ai cittadini. 19 aprile abbiamo contestato, con un parere motivato, la recente proposta di regolamento degli imballaggi. Lo faremo anche per la direttiva sulle case *green* e lo abbiamo fatto in Europa con la direttiva sulle auto

di Stato, in modo che le aziende non abbiano problemi ad accumulare più aiuti contemporaneamente, specialmente per le piccole e medie imprese, verso un *green deal* europeo. Come ultimo punto intervengo sul tema dei rapporti dell'Unione europea con la Cina. Dobbiamo avere una visione strategica comune comune sulla Cina e non avere rapporti bilaterali, come talvolta si ritiene di fare, anche nel raggiungimento del *green deal* europeo, che si vuole imporre alle nostre aziende e ai nostri cittadini, facendo poi accordi con Paesi come la Cina, che non hanno gli stessi criteri, obiettivi e restrizioni sulla transizione ecologica. La riduzione della dipendenza strategica dalle fonti fossili russe dovrebbe quindi indurci, come Unione europea, a ridurre anche la dipendenza strategica dalle produzioni cinesi, spostando in Europa quelle tecnologiche tecnologiche strategiche. Mi riferisco direttamente al settore delle telecomunicazioni, dove le minacce cibernetiche possono essere contrastate solo evitando di utilizzare materiali di grandi fornitori cinesi. La stessa cosa avviene nell'ambito dei semiconduttori, che sono una risorsa importante. L'Italia è strategica in questo: lo hanno capito direttamente anche le imprese straniere, come quelle di Taiwan, che hanno investito nel nostro Paese. Abbiamo sicuramente università, centri di ricerca e piccole e medie imprese È per questo che ritengo che il Governo faccia bene a investire sul tema. Proprio perché ho toccato direttamente il tema di Taiwan, vorrei concludere parlando di questo argomento. Le politiche assertive di Pechino si manifestano in modo crescente nei confronti di Taiwan e dell'Indopacifico, intendono consolidare un allineamento strategico tra Cina e Russia, che mira revisionare il sistema internazionale. È fondamentale invece mantenere lo *status quo* nello stretto. Dobbiamo impegnarci a conservare la pace e la sicurezza in quell'area, non solo per i cittadini, ma anche per le economie internazionali, dato che, secondo gli esperti, un possibile conflitto nell'area avrebbe ripercussioni tre volte superiori rispetto alla pandemia. Quindi ci affidiamo a lei direttamente, *premier* Meloni, proprio perché abbiamo sicuramente la trattazione...

Signor Presidente, la riforma delle regole di *governance* economiche è sicuramente uno dei temi più importanti in discussione nel prossimo Consiglio europeo. Il commissario Gentiloni ha fatto un lavoro importante per cambiare queste regole. Il vecchio Patto di stabilità e crescita aveva dei limiti, che sono stati via via riconosciuti da tutti: l'ottica di breve periodo, il fatto che fosse fondato su variabili non osservabili regole rigide e complicate, che poi alla fine sono rimaste spesso non applicate. Ora la proposta della Commissione supera parecchi di questi limiti: prevede piani di medio termine termine e la spesa primaria netta, quindi una variabile osservabile come unico indicatore operativo, e rafforza la titolarità nazionale delle politiche di bilancio. Certo, nel negoziato i Paesi cosiddetti frugali hanno ottenuto alcune clausole di salvaguardia valide per tutti, ma i passi in avanti sono innegabili. Detto questo, ci sono cose che mancano nella proposta delle Commissioni e noi condividiamo alcune delle valutazioni fatte dal Governo. Manca una *golden rule*, una regola aurea che escluda gli investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale e per la trasformazione del nostro modello di sviluppo che saranno richiesti per i prossimi anni. Manca una capacità fiscale comune dell'Unione europea,

è importante che il Governo italiano si batta per conseguire quegli obiettivi e per migliorare ulteriormente la proposta della Commissione, due convitati di pietra che pesano sulla capacità negoziale del Governo: il primo è la sorte del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Badate: la nostra capacità di attuare il Piano italiano è fondamentale non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, ed è anche per questo che ci preoccupano i ritardi che si sono accumulati nell'attuazione del Piano: sono passati nove mesi dall'insediamento di questo Governo e ne avevate annunciato una revisione, ma

due giorni fa la Commissione europea ha approvato le revisioni proposte da Francia e Malta e nei mesi passati sono state approvate quelle del piano tedesco e di quello del Lussemburgo. Altri sei Paesi quelle carte le hanno ufficialmente presentate. In Italia tutto tace: non c'è nessuna novità e i soldi che dovevano arrivare non sono ancora arrivati nel nostro Paese. Presidente, l'attuazione di quel Piano non è un inciampo fastidioso da derubricare e mettere nel dimenticatoio. Se l'Italia fallisce - e noi rischiamo di fallire, se continuerete ad accumulare ritardi

Con che faccia l'Italia potrà andare in Europa a chiedere maggiore flessibilità, se non dimostreremo di aver speso bene e nei tempi previsti i 200 miliardi di euro che i nostri Governi hanno conquistato in Europa? C'è un secondo convitato di pietra, il meccanismo europeo di stabilità Presidente, la *premier* Meloni ci ha invitato oggi alla Camera a non fare polemiche. È curioso che la Presidente del Consiglio dica all'opposizione quello che può dire o non può dire. Non funziona così, anche perché noi non stiamo facendo polemiche sul MES, stiamo cercando di dire la realtà per quella che è. La realtà è che sul MES la maggioranza sta facendo melina. La realtà è che avete disertato i lavori della Commissione esteri della Camera pur di non votare; la realtà è che vi apprestate a rinviare il voto in Aula alla Camera,

Sarebbe assolutamente controproducente. Credo che siate consapevoli, perché lo ha detto il vostro Ministero dell'economia, che il nuovo meccanismo europeo di stabilità conviene all'Italia. Presidente, la *premier* Meloni ha parlato di un approccio a pacchetto. Traduco: si tiene fermo il MES per negoziare su altro.

Se decidete di dividere i dieci minuti in più parti, non si può pretendere che ciascuna parte vada verso i dieci minuti. È iscritto

siamo alla vigilia di un nuovo Consiglio europeo, che ha molti punti fondamentali su cui discutere, ma che sottolineano soprattutto, per quello che ci riguarda, una grande discontinuità rispetto al passato e di cui siamo particolarmente orgogliosi.

abbiamo portato anche la voce dell'Italia e del Governo italiano. Abbiamo ricordato proprio l'intervento del Presidente del Consiglio al vertice di Reykjavík del Consiglio d'Europa, in cui si diceva che il popolo ucraino con la sua eroica resistenza all'invasione non sta difendendo solamente la sua Patria, ma i valori fondanti dell'identità europea, la libertà, la democrazia, la giustizia e l'uguaglianza tra gli uomini. Se l'Ucraina fosse capitolata, noi vivremmo in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte: è tutta qui la vicenda dell'Ucraina ed è tutto qui il motivo per cui noi siamo e continuiamo ad essere accanto a questo Paese in lotta. Se oggi si può parlare di pace è perché esiste l'Ucraina. E l'Ucraina esiste perché le diverse organizzazioni, l'Unione europea, la NATO e i Paesi occidentali hanno via via fornito armi per resistere, hanno accolto i profughi per solidarietà e hanno fornito risorse economiche e sostegno diplomatico. L'Italia è stata in prima fila con orgoglio e con determinazione. Se oggi l'Ucraina c'è è anche perché l'Italia c'è stata e ha tenuto un comportamento trasparente, chiaro e coerente nel tempo. Non è più quella "Italietta" che balbetta e trova ogni motivo per non impegnarsi, per stare con tutti per non stare con nessuno. negli anni Ottanta, durante la Prima Repubblica, quando i Paesi occidentali ci invitarono a boicottare le Olimpiadi di Mosca, perché c'era stata l'invasione dell'Afghanistan? I russi hanno sempre fatto un po' di queste cose, mandando carri armati di qua e di là. il Governo in quel momento decise di non mandare gli atleti militari, ma di mandare quelli civili, come a dire: stiamo con tutti e con nessuno. Quando sono venuti recentemente alcuni Ministri del Governo iraniano, per non suscitare la loro sensibilità, abbiamo coperto alcune statue, onde evitare di sembrare poco ospitali, mentre quei Ministri nel loro Paese torturavano e ammazzavano gli oppositori politici. *(Applausi)*. Ecco, non è più quest'Italia. Abbiamo scelto l'Ucraina perché l'Ucraina ha scelto noi, perché si trovava in un'area geopolitica a cui era stata assegnata un'influenza particolare dopo la Seconda guerra mondiale, quella sovietica ed ex sovietica; ma poi invece il popolo ucraino ha scelto liberamente di guardare da un'altra parte, di guardare verso di noi e verso quello che noi rappresentiamo, perché abbiamo una concezione dello Stato di diritto che dall'altra parte non c'è, ossia la concezione di chi non fa sconti sul tema della libertà e della democrazia, che vengono prima di ogni cosa. Non potevamo e non volevamo

C'è anche un altro tema, quello dell'immigrazione, sul quale si sta avendo una grande discontinuità rispetto al passato. Il Consiglio europeo finalmente scrive che quello dell'immigrazione è un tema europeo e non è più demandato agli Stati nazionali e soprattutto a quelli come quelli come l'Italia, i cui confini nazionali coincidono con i cosiddetti confini esterni dell'Unione. Siamo soddisfatti, perché la Commissione europea ci ascolta e ci segue. Basta vedere la vicenda tunisina, che ne è un esempio (sì, è proprio un esempio). bastate poche ore, non pochi giorni: di fronte ad un'annunciata tragedia a causa di una situazione molto difficile in Tunisia, che poteva travolgere quel Paese ed avere conseguenze catastrofiche anche sull'Italia e sull'Europa, c'è stato un Governo, con il Presidente del Consiglio in prima persona, che in poche ore ha preso la Presidente della Commissione europea - non un funzionario della Commissione, ma la Presidente - e l'ha portata in Tunisia per risolvere il problema tunisino e per mettere in sicurezza l'Italia e l'Europa. Questa è la differenza di questa nuova Italia che portiamo avanti con grande orgoglio. *(Applausi)*.

pensare alle tante tragedie che accadono nel nostro mare, in particolar nel Mar Mediterraneo, cui non sappiamo rassegnarci e cui non vogliamo abituarci. Allora, se per queste tragedie, come per quelle del Mar Egeo, purtroppo ogni volta abbiamo dovuto commemorare vite che si sono perse nel nostro mare

Davvero possiamo immaginare di aprire le nostre porte non solo alle persone protette dalle convenzioni internazionali, quindi dalle Nazioni Unite e dalle regole dell'Unione europea, ma a tutti quanti? Possiamo cioè accogliere quelle persone che molte volte partono con la voglia di avere un futuro migliore e una speranza,

ulteriormente raccontato oggi alla Camera, quello che viene definito il piano Mattei, per restituire una centralità e una cooperazione vera tra Italia, Europa e Paesi africani, per non cadere nello sfruttamento e creare cooperazione e possibilità di sviluppo. Anche qui, non ci rassegniamo a pensare che l'Africa debba essere la culla della povertà. Non ci rassegniamo a pensare che lo sradicamento e la fuga da quel Paese siano il destino per tutte le persone che lì vivono e crescono, diritto di ogni persona è quello di vivere e di realizzarsi nel proprio Paese d'origine, non quello di scappare. L'emigrazione poi può essere una scelta, ma non dev'essere una scelta obbligata. Presidente, questo è il cambio di paradigma e questa è la discontinuità che abbiamo creato e che stiamo creando con questo Governo. Ecco perché l'appuntamento del prossimo 29 e 30 giugno diventa fondamentale, non tanto e non solo per i risultati che ne scaturiranno, ma per ribadire, ancora una volta, la nuova identità della nostra Italia. Rispetto a chi mi ha preceduto e che, come al solito, ha fatto un po' il menagramo e raccontato sciagure, dico che sono le stesse che raccontavate anche in campagna elettorale. I risultati sono diversi: sappiamo qual è stato il nostro successo e sappiamo qual è l'accredito di cui oggi godiamo in Italia e nel resto del mondo.

non significa inanellare compromessi continui, ma scegliere. E noi abbiamo scelto, scegliamo e sceglieremo sempre ciò che è giusto per il bene del nostro popolo. Buon lavoro, presidente

Signor Presidente, colleghi, nel mio breve intervento vorrei soffermarmi su uno dei temi principali che verrà affrontato nel prossimo Consiglio europeo, vale a dire il conflitto in Ucraina, anche in relazione agli ultimi avvenimenti che sono accaduti in territorio russo. La ribellione di Prigozhin nei confronti del Governo russo e la marcia dei suoi mercenari verso Mosca ha evidenziato a livello internazionale la portata della crisi in atto in Russia, costringendo Putin a fare i conti con il fuoco amico del gruppo Wagner, la spietata milizia privata che ha fatto per lui il lavoro sporco, non solo in Ucraina, ma anche in molteplici scenari, come quello africano. non si è scoperto nel *weekend* appena trascorso che il *leader* del gruppo Wagner fosse fortemente deluso e amareggiato dall'andamento dell'invasione russa in Ucraina, ma il sentore di un vero e proprio ammutinamento contro il Cremlino non era assolutamente percepito a livello generale. I servizi segreti occidentali pare avessero notizie in tal senso, ma nell'elaborazione politica del nostro, come di altri Paesi, non si pensava certo a un possibile *golpe*. Questo fatto ha innescato una serie di problematiche non previste, le cui conseguenze non sono oggi determinabili. Tuttavia, la gravità della posta in gioco deve indurre tutti noi a non scartare alcuna ipotesi e ad agire di conseguenza, con grande fermezza, ma anche grande prudenza. La Russia infatti è un Paese complesso, che nella sua storia non ha mai conosciuto vere forme di Governo pienamente democratico come da noi intese o conosciute. Sarebbe perciò sbagliato e pericoloso, come invece avvenuto in passato per altre situazioni di crisi, leggere gli avvenimenti e muovere le azioni dei nostri Governi secondo i canoni interpretativi occidentali, che, giusto per fare degli esempi, nel caso dell'evoluzione delle cosiddette primavere arabe, hanno dimostrato di non essere adeguati alla comprensione di realtà storiche, sociali e culturali così diverse dalla nostra, aggiungendo - non dimentichiamolo - che la Russia mantiene il più vasto arsenale nucleare del mondo. Nell'immediatezza degli avvenimenti, in questo senso, bene ha fatto il nostro Governo, di cui la Lega fa orgogliosamente parte, a ribadire la posizione italiana, che, da un lato, è di sostegno al popolo ucraino, ma al contempo, con saggezza e misura, è volta a non entrare nel merito degli accadimenti riguardanti la Federazione Russa, al fine di evitare una pericolosa *escalation* derivante da una disordinata destabilizzazione di quel Paese, che metterebbe seriamente a rischio la sicurezza mondiale, con evoluzioni che al momento non appaiono prevedibili. Mentre il mondo tira un sospiro di sollievo per non essere passati dalla padella alla brace, lasciatemi registrare la piccolezza e, per certi versi, il provincialismo di alcuni organi di stampa italiani, che passano la giornata a disquisire se il presidente Biden abbia o non abbia chiamato la presidente Meloni, per poi scoprire che la telefonata c'è stata, e allora si lanciano in uno *slalom* gigante su quanto sarebbe durata la chiamata: troppo corta, troppo lunga, di pura cortesia e così via.

sta presentando il conto a Putin, con tutto quello che ne consegue in termini di morti, distruzione e orrore che lui stesso ha innescato e messo in atto, dall'altro lato la storia sta nuovamente bussando alla porta di noi occidentali che abbiamo il privilegio di vivere in società libere e aperte. Oltre al privilegio, la storia ci impone però anche l'onere di muovere i nostri pensieri e le nostre azioni con saggezza e lungimiranza per il bene dell'umanità ed è in questa direzione che tutti insieme dobbiamo pensare ed agire. Sono certo che che il Governo che lei presiede sarà pienamente all'altezza del compito gravoso che ci aspetta. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, il cosiddetto Patto europeo sui migranti raggiunto l'8 giugno scorso, pur prevedendo un meccanismo diverso dal precedente, si sta rivelando una farsa, che però diventa

Paesi di primo ingresso, un accordo, cioè, che non supera minimamente l'impianto e le stesse problematiche del Regolamento di Dublino, perché non garantisce una diffusa solidarietà a livello europeo dei ricollocamenti. Ancora una volta, si è trattato di un'occasione mancata, è mancata una visione europea e nazionale delle politiche da perseguire sul versante immigrazione. Dopo i tragici e ancora non chiariti fatti di Cutro, due settimane fa abbiamo assistito a un'altra tragedia terribile nel Mediterraneo. La Grecia, in piena campagna elettorale,

Il Partito Democratico, facendosi anche portavoce di molte associazioni e di molti cittadini, chiede l'istituzione di corridoi umanitari che potrebbero garantire a chi arriva in Europa un viaggio senza rischi e a chi arriva lo *status* di rifugiato e non più di richiedente asilo: è l'unica via di accesso legale per soggetti vulnerabili,

Lo dice un sindaco di Fratelli d'Italia, come quello di Pordenone, che ieri al giornale «Il Gazzettino» ha dichiarato che siamo tornati al 2016, tornano i bivacchi, le attese sono per un'estate ancora più pesante. Ecco, ricordiamo bene come ci attaccavate in quel 2016; ma la rotta balcanica è un fiume che si ingrossa, e il tempo della propaganda, quando si governa, finisce. Tocca a voi governare un fenomeno strutturale come le grandi migrazioni, e non ci state riuscendo. Infine, proprio perché provengo da una realtà vicina ai Balcani e abbiamo interesse specifico affinché Europa e Italia assicurino stabilità nell'area balcanica, vorrei ricordare a lei a quest'Assemblea che i sei Paesi dei Balcani occidentali ancora non UE sono al centro del processo di integrazione dell'area. Quei Paesi costituiscono costituiscono diretto e strategico interesse dell'Italia e, come dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, bisogna avvicinarli al mercato unico dell'UE, approfondire l'integrazione economica regionale, accelerare le riforme fondamentali e aumentare i fondi di preadesione. Pensiamo che una loro rapida e solida adesione sia nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, al fine di produrre una maggiore sicurezza per l'intero continente e al contempo limitare l'attività della criminalità organizzata, le minacce terroristiche, gli stessi fenomeni migratori. Pensiamo che vada ancora più più intensificata - anche in coordinamento con i Paesi UE dell'area - l'azione dell'Italia sui punti più caldi a rischio di crisi, a cominciare dal rapporto tra Kosovo e Serbia. Si deve favorire un compromesso a un accordo globale fino alla normalizzazione delle relazioni, dedicando uguale impegno politico ed economico alla Grazie a tutti focalizzato sui trasporti e le reti energetiche. Questo alla luce del ruolo cruciale che sta giocando il Mar Adriatico in questo momento storico dal punto di vista logistico e geopolitico. Vorremmo, dunque, che il Governo italiano si impegnasse su queste questioni invece di inseguire obiettivi rivelatisi per lo più propagandistici.

Signor Presidente, illustre Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nei prossimi giorni vivremo un appuntamento europeo molto importante che ci proietterà verso gli ultimi passaggi di una legislatura europea che ha dovuto attraversare molte difficoltà: la crisi economica, la pandemia del Covid, la crisi migratoria, la guerra in Ucraina. In tutti questi momenti, il nostro partito - sotto la guida del presidente Meloni si è fatto trovare sempre pronto, quando era all'opposizione e ancora di più oggi che è il primo partito della coalizione e guida il Governo della Nazione. Si è fatto trovare pronto, quindi, per dare una risposta seria ai cittadini italiani ed europei. Colgo l'occasione, presidente Meloni, per farle gli auguri per la riconferma alla guida del Partito dei Conservatori e

del Consiglio ci sarà la questione ucraina e il perdurante conflitto bellico con la Russia. Nelle scorse ore abbiamo assistito al tentativo di colpo di Stato dei mercenari del gruppo Wagner, che non è riuscito nel suo intento, e quindi oggi la Russia è ancora nelle mani di Putin. Sarà compito del Consiglio europeo rivolgere molta attenzione a quanto sta accadendo e ai riflessi che tale azione avrà sul conflitto in Ucraina e sullo scenario globale. Tutti gli Stati europei, tutti gli Stati membri della NATO sono pienamente impegnati a garantire il pieno e incondizionato sostegno finanziario, economico, umanitario e diplomatico alla sovranità dell'Ucraina. Si parla molto del cessate il fuoco e di una prospettiva di pace; vogliamo ribadire la necessità di arrivare alla pace, ma che sia una pace giusta e duratura, basata sul pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, riconoscendo a Kiev la libertà di aderire alla NATO e di diventare membro della Comunità europea. Bisognerà poi affrontare il tema della ricostruzione; sul punto l'Unione europea ha già stanziato 18 miliardi di euro e altri 50 sino al 2027 sono previsti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale. caso avremo un modello che assomiglia molto al *recovery plan,* con 33 miliardi di prestiti e 17 di sovvenzioni e un sistema di controlli per bilanciare le erogazioni con specifiche riforme che lo Stato ucraino si dovrà impegnare a fare.

Il 31 dicembre, dopo ben quattro anni, sarà disattivata la clausola di sospensione del Patto e si dovrà quindi tornare all'applicazione delle regole fiscali europee. L'Italia lavorerà incessantemente perché queste regole siano nuove, più moderne e finalmente associate a programmi di sviluppo e di investimenti per la crescita. È fondamentale che questo nuovo assetto di regole eviti il ritorno ad un quadro che imporrerebbe obblighi non più sostenibili per il nostro Paese e per molti altri. Come Italia siamo fortemente impegnati e lavoriamo per ottenere una riforma della *governance* economica in grado di assicurare adeguato sostegno agli investimenti pubblici, quelli per la transizione verde e digitale, quelli per la difesa e quelli in adempimento dei programmi europei. In buona sostanza, ci si dovrà attivare affinché queste spese siano escluse dal meccanismo di calcolo del nuovo Patto di stabilità e crescita, perché è utile, ad esempio, raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione, ridurre la dipendenza strutturale dalle energie fossili e così via. Vogliamo che l'Europa torni ad essere un gigante politico e mai più solo un nano burocratico. Sui temi dell'economia desidero portare la nostra attenzione anche sul tema delle materie prime, sulle quali l'Europa sta lavorando ad un piano per ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti da fornitori terzi. L'altra materia sicuramente affrontata domani a Bruxelles sarà quella migratoria. Si tratta di una sfida dell'Unione europea che richiede una risposta europea: le frontiere italiane sono frontiere europee e l'Europa è chiamata a difenderle. Il tema è dibattuto da anni, soprattutto in Italia, Paese di primo approdo e porta del Mediterraneo che da anni si fa carico di una solidarietà europea troppo spesso declamata a parole, ma poco praticata nei fatti. di fronte a flussi migratori con numeri così importanti, è mancata proprio la solidarietà tra gli Stati. Su questo punto, come forza politica siamo fieri di aver posto per primi la questione, rendendola una priorità ormai non più rinviabile per l'intera comunità europea. Non possiamo attendere inermi il prossimo naufragio a causa di viaggi irregolari organizzati da trafficanti di esseri umani. A proposito, tutti ci uniamo, signor presidente del Consiglio Meloni, al cordoglio che lei ha espresso per la recente tragedia al largo delle coste greche.

a favore di soluzioni a lungo termine sia in Tunisia che negli altri Paesi, con strategie mirate sulle rotte seguite dai migranti. A proposito, è del 25 giugno la lettera del presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen che fa riferimento a ciò che è stato fatto in Tunisia e lo indica come modello da seguire. In soli pochi mesi l'Esecutivo ha portato avanti un lavoro encomiabile, sia per le tematiche macroeconomiche di interesse internazionale, sia per quanto sta facendo in Italia. Il Paese inizia a respirare un'aria nuova e, nonostante le tante difficoltà, stiamo portando avanti la nostra agenda politica, nel solco di una netta posizione atlantista e filo-occidentale e lavorando con l'Europa, grazie anche agli incessanti sforzi del ministro Fitto affinché le risorse del PNRR vengano spese correttamente e nei tempi stabiliti, in ogni caso usando sempre i criteri del buon senso e della ragionevolezza. Fondi del PNRR, che, ove ci fosse ancora bisogno di ribadirlo - lo ha detto più volte il Ministro e lo ha ribadito stamane il Presidente del Consiglio saranno utilizzati per gli investimenti e non per le armi. Insomma, in pochi mesi il lavoro dell'Esecutivo e del presidente Meloni può essere riassunto in tre parole: chiarezza, coerenza e coraggio. La chiarezza di chi in campagna elettorale ha raccontato il suo programma e ora dai banchi del Governo sta onorando il patto con gli italiani, il mandato affidatogli dagli elettori, rappresentando con orgoglio la propria visione del mondo. La coerenza, sì, quella di chi non ha mai rinunciato alle sue idee, a prescindere dalle poltrone e anche a costo di sacrifici e rinunce, come testimonia il percorso di opposizione nella scorsa legislatura. Infine, il coraggio il coraggio di chi non ha avuto paura di mettersi in gioco, di chi ha lottato e combattuto, gettando il cuore oltre l'ostacolo prima di raggiungere la cima e la vetta. Voglio ricordare le parole del presidente Meloni - presumo che me lo consenta - che ha usato in occasione della Conferenza programmatica di Milano: saliremo e più porteremo con noi ciò da cui proveniamo. Più saranno i sogni che avremo e più sarà nostra responsabilità ancorarli alla realtà. Più avanzeremo e più tenderemo la mano a chi è rimasto indietro. Ma, soprattutto, si sappia, l'unica ragione per la quale vogliamo arrivare in vetta è perché sappiamo che da lì possiamo guardare più lontano». Grazie, presidente Meloni, aveva proprio ragione.*(Applausi)*. Mi avvio dunque alla conclusione, signor Presidente.

Gli indicatori statistici indicano un raddoppio delle stime sul PIL, smentendo le previsioni dei detrattori e consegnandoci una Nazione in cui i consumi crescono trimestre su trimestre. Possiamo dire - e chiudo, signor Presidente - che il lavoro fatto dal Governo in pochi mesi viene apprezzato da chiunque, tranne che dalle opposizioni, forse nostalgiche del servilismo nei confronti della Merkel e abituate per decenni supinamente a subire le imposizioni esterne. Siamo stanchi di assistere a polemiche su tutto

quando invece l'interesse dell'Italia in questo momento è affrontare il negoziato sulla *governance* europea. Chi polemizza a tutti i costi comunque non ha a cuore il bene della Nazione...

*(Misto)*. Signora Presidente del Consiglio, ho trovato le sue comunicazioni nel complesso convincenti e, a mio parere, meritevoli dell'appoggio del Parlamento. Sottolineo tre punti. Il primo è una sua affermazione presentata in modo incidentale, ma della quale può e deve essere fiera - e lo è - e che per il suo Governo rappresenta un impegno. riferisco a quando lei dice: «Senza venir meno a quella disciplina di bilancio sulla quale il Governo italiano ha dimostrato serietà fin dalla manovra finanziaria con buona pace dei gufi che preconizzavano catastrofi di ogni sorta» (e non mi riferisco tanto a quest'ultimo dettaglio). dettaglio). Su questo punto, signora Presidente, non rivendica l'interesse nazionale, ma lo ha fatto, forse su questo punto più che su qualsiasi altro. È proprio con questa linea che lei fa gli interessi dell'Italia e ha acquistato credibilità in Europa. Ha avuto la capacità - non lo voglio dire a voce troppo alta, per non determinare reazioni che a lei non gioverebbero non gioverebbero - di portare con sé, finora, anche componenti della sua maggioranza tradizionalmente riluttanti alla disciplina di bilancio. Questo, per l'Italia e per l'Europa, è un tema enormemente più rilevante, nella sostanza, di quello chiamato MES. Il secondo punto su cui voglio soffermarmi, sperando di avere la sua attenzione, signor Presidente, è proprio quello del MES. Non pensavo di parlarne oggi, ma lei lo ha fatto in modo così nitido, nella sua comunicazione, che mi sento in dovere di farlo. Sulle cose che lei ha detto sul MES, per metà sono d'accordo, per metà no. La metà su cui sono d'accordo è quando lei dice: «Per questa ragione voglio dire con serenità, ma anche con chiarezza, che non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES». Sono totalmente d'accordo con lei. Sono meno d'accordo su quanto segue: «L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova *governance* europea con un approccio a pacchetto, nel quale le regole del Patto di stabilità, il completamento dell'unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutano nel loro complesso». Mi permetto di osservare che spesso la prospettiva dei pacchetti è utilissima e cruciale, ma dipende. In questo pacchetto ci sono due cose, come il completamento dell'unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria su cui gli altri al tavolo europeo potranno dirle: il MES è stato concepito il pacchetto tra l'Italia e l'Europa, che non è determinato solo da lei, ma anche dagli altri, ha un nuovo petalo nella rosa, davvero molto importante. la posizione finora occupata dal membro italiano del comitato esecutivo della Banca centrale europea potrà essere o meno ancora occupata da un italiano, dopo la partenza del futuro governatore Panetta. Quindi, affidarsi a questo pacchetto lo considero sinceramente un po' periglioso.

ma farebbe anche l'interesse europeo e quello dell'economia europea di fronte alle sfide geopolitiche ed economiche di Stati Uniti e Cina. L'Italia, in un momento in cui Francia e Germania - io dico «purtroppo» - sembrano aver trovato come unico comune denominatore la larghezza negli aiuti di Stato,

che preservi il mercato unico è inseparabile da un approccio europeo alla competitività; è sotto gli occhi di tutti come, senza finanziamenti europei erogati indipendentemente da capacità fiscali nazionali, si rischi solo di aumentare le disparità, favorendo alcuni Paesi a discapito di altri». Ebbene, credo che sarebbe un grande paradosso se l'Europa, volendo

dicesse questo a parole, ma nei fatti mandasse a Washington e a Pechino tutt'altro messaggio, magari in latino: *divide et impera.* Se ci dividessimo tra noi, come le politiche franco-tedesche, spesso preziose, questa volta rischiano di fare, allora non sarebbe quello che né l'Italia, né l'Europa devono volere.

è una grande soddisfazione politica prendere atto del cambio di passo a 180 gradi effettuato dal suo Governo rispetto alle affermazioni del recente passato. L'ostilità per l'Europa più volte manifestata dalla sua parte politica, fino alla campagna elettorale dello scorso settembre, con la volontà espressa più volte di uscire dall'euro, la simpatia per Putin e l'antipatia per gli Stati Uniti hanno ceduto il passo a una fedeltà quasi incondizionata all'Unione europea e alla peraltro condivisibilissima, a mio avviso, scelta di campo inequivocabile a favore dell'Ucraina. Machiavelli diceva, nel "Principe", che chi governa deve avere due paure, una da *drento* e una da *fuora*. Allora però il regnante era tale per motivi dinastici, mentre ora viene eletto, ed è giusto così; ma per essere eletto deve ingraziarsi quelli da *drento*, che poi dovrà temere nel momento in cui invece essi potranno creargli dei problemi di Governo. Da qui ovviamente nasce la capovolta a 180 gradi. Capita a tutti, ma voi lo fate meglio di tutti quelli che vi hanno preceduto, perché lei, Presidente, è dotata di un eccellente *team* di comunicazione, che ha elaborato delle espressioni straordinarie che ogni rappresentante della maggioranza di Governo continua a ripetere. Per esempio: chi c'era prima ha lasciato solo macerie, che noi abbiamo ereditato, e ci vuole tempo per ricostruirci sopra. È vero, ma ormai sono passati nove mesi e qualcosa dovrebbe essere stato ricostruito; in ogni caso, non potrete continuare a dirlo per cinque anni (e io mi auguro che governiate per cinque anni). È cambiato il vento, mentre il vento ha sempre soffiato; diversa è stata ed è la capacità di manovrare le vele, però bisogna anche dimostrare di saperlo fare. E poi: il popolo ci vuole. Certo, è vero; ma, se facciamo i conti dei voti espressi a settembre, il centrodestra non aveva la maggioranza dei voti. Ha vinto perché era unito, ha corso unito e continuando a correre unito vincerà sempre, perché, se ha degli avversari che si dividono, non c'è verso e finirà sempre così. Il centrosinistra non è mai stato capace di fare una perenne campagna elettorale con la stessa compattezza del centrodestra. Quindi siete bravissimi, vi ammiro, ma alla fine la storia vi misurerà per i mattoncini che avrete portato nella costruzione del Paese del futuro. Tra le diverse affermazioni contenute nel suo intervento, Presidente, mi permetta di segnalargliene alcune. A pagina 1 lei dice che nel Consiglio europeo straordinario di febbraio scorso, grazie all'azione dell'Italia, è stato finalmente riconosciuto da tutti i 27 Stati membri e dalle istituzioni europee che la migrazione è una sfida europea e richiede risposte europee. Siamo d'accordo, ma questa considerazione era già espressa in almeno tre risoluzioni europee, nel 2009, nel 2016 e nel 2018; quindi già altri ci avevano pensato. A pagina 2 lei parla del piano Mattei per l'Africa; io sono d'accordissimo che venga fatto, ma le ricordo che il problema dell'Africa non è solo energia, ma anche acqua, cibo e pace sociale. Per quanto riguarda i migranti, divisi tra migranti economici e migranti con diritto di protezione internazionale, gli Stati Uniti non sarebbero quello che sono se allora ci avessero accolto in questo modo. In realtà il problema è fare selezione e cercare di fermare da noi quelli che sanno fare delle cose, come succede in Germania e in Francia. Bene la fermezza sull'Ucraina e il ringraziamento delle Forze armate. Sono dell'avviso che l'opposizione sia presente e, per quanto riguarda le misure da adottare contro l'inflazione, se avete bisogno ci siamo. *(Applausi)*. finestra") *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, nel Novecento c'era chi diceva che i fatti hanno la testa dura. Allora potremmo tradurre questa allocuzione in numeri. I numeri dei migranti che, nello stesso periodo in cui lei è arrivata al Governo, si sono triplicati rispetto all'anno precedente: 61.268 arrivi, rispetto ai 27.346 dello stesso periodo dell'anno precedente, come le può confermare il Ministro dell'interno che è lì vicino a lei. Questo denota che sono state inefficaci tutte le misure sin qui assunte, che sono state configurabili al livello della propaganda. Le ricordiamo: lo stato d'emergenza, la lotta ai trafficanti sull'intero globo terracqueo e lo stesso accordo europeo, che non lascia sul campo la soluzione delle due questioni chiave, la volontarietà della redistribuzione e il tema dei Paesi di primo approdo contenuti all'interno del Trattato di Dublino. Insomma, lei sa che questo dell'immigrazione, insieme col PNRR, signora Presidente, è la vera potenziale pietra di inciampo del suo Governo. È per questo che serve un salto di qualità, ad iniziare dalla Tunisia. Lei ci ha parlato di approccio "a pacchetto" sulla Tunisia e sul MES: non ironizziamo su cosa potrebbe lessicalmente trasformarsi il pacchetto, ma guardiamo ai fatti. Al di là della retorica, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione europea sono andati a Tunisi e appena sono decollati il Presidente tunisino ha sbattuto la porta, perché evidentemente non accettava un approccio sulla base del quale, per poche decine di milioni, avrebbe dovuto fare il poliziotto per conto dell'Europa. *(Applausi)*. Serve un salto di qualità politico, che non è la rincorsa ad una banca. È la capacità di mettere in campo un'azione specifica. Guardi, le soccorre un precedente: nel 2016, quando l'Europa era nelle condizioni peggiori rispetto alla questione della Tunisia sulla vicenda siriana, si misero sul campo 3 miliardi in un accordo anche contestato per molte sue parti con il presidente Erdogan, che vide però un protagonismo. Faccia questo: vada in Europa a chiedere un intervento politico che porti in Tunisia una vera capacità di investimenti su quel Paese. Altrimenti, lo sa meglio di me: entrerà la Cina con tutte le conseguenze del caso. Allora, su questo noi le chiediamo di essere coerente e conseguente e l'abbiamo scritto nella nostra mozione. Denunci fin d'ora che il nostro Paese non prorogherà l'adesione alla Belt and road initiative, alla Via della Seta, perché diversamente si rischia di essere in contraddizione dei termini. In conclusione, tra un fervore retorico di antica memoria, signora Presidente, che le abbiamo visto fare anche questa mattina, e la rotondità dorotea di chi ambisce al ruolo di nuova Merkel europea che butta la palla in *corner* rispetto ai nodi, noi preferiremmo che lei seguisse la frase di un suo predecessore molto autorevole, che diceva che la politica - ho concluso, Presidente - vuol dire realizzare. Ecco, ci eviti i comizi, ci eviti i rinvii e realizzi, a cominciare dal MES.

colleghi, Presidente del Consiglio, alla vigilia del Consiglio europeo bene ha fatto, Presidente, a riportare nelle nostre Aule parlamentari, riordinandoli, i temi ai quali siamo chiamati a dare risposte adeguate come Paese e come Europa. Il Consiglio europeo del 29-30 giugno avrà ancora al primo posto la questione ucraina. L'Unione europea continua il proprio sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico alla controffensiva ucraina ed è bene che sia così. Certamente, gli ultimi eventi, l'ammutinamento di buona parte dei combattenti sul campo della milizia Wagner e prima di questo la distruzione della diga hanno segnato delle importanti novità su quel campo. La crisi Ucraina ha avuto anche un forte impatto sull'economia del vecchio continente e del nostro Paese in particolare: questo è bene ricordarlo anche ai nostri alleati europei. Sulla politica industriale ha evidenziato come sia necessario ridurre le dipendenze strategiche, in particolare in quelle aree che sono più sensibili e per quei materiali da cui dipendiamo di più. Ebbene, la riflessione sta avvenendo sia nel nostro Paese, per iniziativa del ministro Urso, sia a livello europeo, sui materiali rari, sui materiali preziosi per la nostra indipendenza tecnologica. Noi confermiamo la nostra posizione, cioè un atlantismo maturo e convinto e un europeismo concreto che disdegni i proclami senza avere i contenuti. quindi il nostro totale appoggio all'Ucraina, sia con gli aiuti economici (quindi continueremo su questa strada), con quelli militari, al di là di tante anime belle che vorrebbero distinguere i due elementi. E questo lo dobbiamo fare senza esitazioni. Si tratta però, signor Presidente, anche di ricostruire un approccio adeguato con i nostri *partner* europei, come dicevo prima. Non può essere che se l'Italia affronta il tema migrazione con una certa rigidità veniamo subito accusati di razzismo, mentre se la stessa cosa la fa la Francia è invece nazionalismo. Da questo equivoco dobbiamo uscire, perché non possiamo continuare anche in quest'Aula a doverci sentire contare il numero degli sbarchi da chi, fino a poco tempo fa, ci diceva che invece andava bene così. *(Applausi)*. È evidente che servono degli accordi internazionali, soprattutto nel Mediterraneo, però è anche evidente che indeboliamo la nostra posizione continuando ad attaccare qualsiasi tentativo venga fatto in questa direzione. Non può essere che se la Germania pone un problema economico è un fatto politico assolutamente rispettabile, mentre se lo facciamo noi invece è un ricatto. No, non può essere così e su questo dobbiamo essere chiari.

riportare l'Europa alla sua vera vocazione, cosa che non si fa da troppo tempo; costruire l'Europa dei popoli, che oggi ancora non c'è, ponendo al centro i valori che l'hanno costruita, sui quali è fondata e che la costituiscono ancora oggi, altrimenti non ci sarebbe un'Europa. Anche su questi valori dobbiamo essere concreti e realisti. MES, Patto di

diventa un tema unico che merita un accordo complessivo, non per trattare con le tre, quattro carte o che dir si voglia, ma è un accordo complessivo ed è necessario che sia così, perché l'uno influenza l'altro: non nascondiamocelo, e chi dice il contrario sa di mentire. Possiamo avere dei dubbi sul fatto che il MES, così come è stato pensato, possa non dare adeguate garanzie non solo all'Italia, ma a tutti i Paesi che aderiscono, e che possa non dare adeguate garanzie calato nell'attualità, nell'oggi? Lo strumento MES è assolutamente condivisibile e credo sia un'invenzione assolutamente appropriata ai tempi, ma la modalità di accesso e, ancora di più, le garanzie che non ci sono sul controllo di questo istituto credo che siano determinanti per valutare lo strumento nel suo complesso. Giustamente il Governo sta sollevando questo problema, perché questo strumento deve rientrare in un controllo un controllo degli Stati dell'Europa che ci deve essere. Non possiamo pensare di attivare uno strumento che non ha più nessun controllo, ma vive in autonomia, avendo responsabilità diretta e influenza diretta sull'economia dei singoli Paesi. Un comportamento come questo, che chiede garanzie e controllo, credo che rientri assolutamente in un comportamento responsabile, doveroso da parte del nostro Paese. Quindi è bene che il Governo abbia intrapreso questa strada e che chieda anche agli altri Paesi una conferma rispetto a tali temi. Su questo dobbiamo chiedere, esigere ed avere risposte; senza risposte non ci sono le condizioni, e non è che non ci sono per un capriccio o per un ricatto: non ci sono perché non ci sono. Su questo dobbiamo essere chiari. L'Italia deve recuperare un ruolo anche trainante, come diceva il senatore Monti. Vale con la Francia e con la Germania, ma dobbiamo essere in grado di portare dei temi ad un tavolo autorevole che possa vedere l'Europa recuperare la propria iniziativa. Quindi, bene ha fatto il Governo, e forse dovevamo farlo prima, a sollevare dei dubbi sull'utilità dell'ennesimo rialzo dei tassi preannunciato, perché pone la domanda a chi serva: non certo ai cittadini e non certo al nostro debito pubblico. Non ci possiamo permettere di passare direttamente dall'inflazione alla recessione e questo credo che sia chiaro a tutti.

Meloni, lei ha davvero il compito di richiamare l'Europa ai propri doveri, di riprendere un ruolo da protagonista e richiamare l'Europa ad un approccio maturo e responsabile, non nel solco della sola rigidità, ma che sappia guardare alle diverse esigenze degli Stati e dei cittadini. Quindi, più attenta agli effetti, prima ancora che ai soli principi, senza guardare dove questi ci portano. Insomma, è necessario un approccio costitutivo di una nuova responsabilità europea. E noi siamo certi, presidente Meloni, che lei saprà bene interpretare questo ruolo.

torniamo ai temi di interesse dell'Unione europea. Presidente Meloni, vedo che lei è molto attenta e che ha preso un bel po' di appunti. Spero di fornirle ulteriori spunti da portare, per conto della nostra Nazione, all'interno dell'Unione europea. Iniziamo dalla guerra: dal vile, vigliacco attentato, l'invasione, da parte dei russi di Putin, al popolo ucraino. Palese violazione di diritti internazionali: lo voglio sottolineare, affinché nessuno possa avere dubbi su come il MoVimento 5 Stelle definisca questo atto. Ribadisco: vile attacco in violazione di diritti internazionali. Su questo non ci devono essere dubbi e nessuno ne deve avere. Provo ora ad agganciarmi alle vicende legate

cambiato rotta, andando verso Mosca. Ora le farò capire dove voglio andare a puntare. Parliamo della Russia, una delle Nazioni più potenti al mondo, anche dal punto di vista militare, con un arsenale nucleare che ha pochi pari. Si parla di oltre 6.000 testate nucleari: quindi, stiamo parlando di un ingente contingente militare. Ora, io voglio parlare di stabilità di grandi aree, di stabilità degli Stati, che possono essere messi in crisi anche da rivolte interne, non so se autoalimentate o alimentate dall'esterno. Invito alla riflessione, facendo un piccolo parallelismo. Nel 2011, noi abbiamo appoggiato la destabilizzazione della Libia. Abbiamo visto come un piccolo Stato, destabilizzato su iniziativa di Regno Unito e Francia, con l'appoggio dell'Italia (lei era Ministro a quei tempi), creato grandissimi danni, con riverberi diretti sull'Italia, perciò sul confine meridionale dell'Unione europea. Lascio a lei concludere cosa potrebbe capitare in caso di destabilizzazione di una Nazione come la Russia, in presenza di un personaggio che non è proprio da può definire equilibrato come Putin. Pertanto, io la invito, anche nel nel foro dell'Unione europea, in quel contesto internazionale, a far capire anche agli altri Stati che continuare a soffiare e a spingere sull'idea che noi dobbiamo battere militarmente la Russia, non è proprio la soluzione che ci può portare il massimo dei vantaggi, come non lo è la destabilizzazione di quello Stato. Lo lancio come monito, ne faccia ne faccia il miglior uso possibile. Noi siamo contrari, l'abbiamo detto in maniera chiara. Oggi in dichiarazione di voto un membro del suo partito politico

vogliamo una Nazione che continui, nel solco della propria storia, a mantenere l'equilibrio. La nostra è una Nazione che all'interno della propria Carta ha scritto in maniera chiara che è per la pace e affinché la pace venga

mettendosi al fianco di Regno Unito e Stati Uniti, spingendo sul bellicismo estremo, rilanciando l'azione o la richiesta ucraina di carri armati

facendosi capofila di un gruppo di Stati per la mediazione. Ora non ci rimane che riporre speranza nello Stato Pontificio, nell'opera del cardinal Zuppi e nel Padreterno.

allo scorporo dal Patto di stabilità e crescita di tutti gli investimenti per la transizione verde, per le energie pulite, per la sanità, per gli equilibri sociali, ma sicuramente non di quelli per le fabbriche di morte.

continua a essere uno dei Paesi di primo approdo, perciò è fra quelli più impattati insieme a Spagna e Grecia, ma non è cambiato nulla da quel punto di vista. Su di noi è rimasto sempre l'onere

non abbiamo raggiunto l'obiettivo, pertanto ci faccia capire per cosa stiamo esultando: forse per il fatto che nel caso in cui gli altri Stati

Abbiamo fallito su tutta la linea e dico "noi" perché quando chiediamo a lei di rappresentarci in Europa, ci sentiamo parte di questa Nazione, non vogliamo sicuramente essere detrattori

questi signori ci stanno prendendo in giro, oppure lei, siccome è blindata e costretta in un perimetro insieme ai suoi amici e colleghi sovranisti, si ritrova a non poter fare più di quanto ha fatto. *(Applausi)*. Ce lo dica: non vuole scontentare Orban o gli amici polacchi?

prendono la briga di dire che anche voi tenete tantissimo alla lotta ai cambiamenti climatici, che avete a cuore la biodiversità,

quando lei e i suoi Ministri continuate a bloccare quel processo a livello di Unione europea. È di qualche giorno fa un ulteriore stop dell'Italia; parlando di tutela di ecosistemi. Avete addotto giustificazioni false: non è vero che bloccando la legge sulla biodiversità e sulla protezione degli ecosistemi andrete a difendere

con dati tangibili; pertanto utilizziamo questi dati. Bloccare quel tipo di azioni è una follia. Vi invito a tornare sui vostri passi perché il pianeta non può più attendere.

i quali ci chiedono soprattutto una cosa, quando si tratta di rapporti internazionali: essere rispettati. Questo era ciò che chiedevo io da elettore ai miei rappresentanti e mai lo ottenevo, perché storicamente il punto di vista dei nostri rappresentanti in Europa era permeato dall'idea del Partito Democratico, che è sempre stata solo una, e Conte è andato in continuità con quell'approccio: dobbiamo dire sempre di sì e saremo rispettati. Ma questo è il rispetto del servo! Come si fa a pensare che il rispetto che i nostri cittadini chiedono sia quello dell'inchino costante, sperando che poi caschi qualcosa dalla tavola dei signori per poterlo mangiare nella nostra ciotola? Questo è un aspetto che personalmente non ho mai tollerato, e adesso che arriviamo a decisioni importanti dobbiamo ricordare che in Unione europea il rispetto - e ce lo insegnano proprio quei signori che noi, nel nostro complesso di inferiorità, abbiamo sempre guardato dal basso in alto - tante volte si ottiene dicendo no, quando si va contro l'interesse nazionale. Se l'interesse nazionale dice che bisogna dire di no, si dice di no, anche da soli. il simbolo della Lega è Alberto da Giussano, che era un combattente per la libertà, leggendario; qualcuno dice che non sia mai esistito, certi combattenti per la servitù, mi viene da pensare che effettivamente è difficile trovarne uno. Ad ogni modo, lui era uno di quelli, almeno nell'idea dell'italiano, un combattente per la libertà, interesse nazionale, che riusciva a mettere assieme tutti coloro che normalmente erano nemici l'uno con l'altro, di solito sempre abituati, come nella storia d'Italia, a preferire la sventura del vicino piuttosto che la servitù straniera.

infatti ha detto: vergogna, dobbiamo essere pronti a combattere per la nostra libertà, per non essere sotto una dittatura, anche a costo della vita, altrimenti non ci sarebbe Falcone, non ci sarebbe Borsellino, non ci sarebbero tanti degli eroi della nostra storia. Io sono d'accordissimo,

si aggirino i cauti, quelli che arrivano e dicono che bisogna stare attenti perché abbiamo tanti titoli di Stato da collocare, perché poi ci attaccano, perché poi non ci danno quello che vogliamo. Colleghi, sull'economia vorrei ricordare sempre che nell'Unione europea siamo quelli che pagano, quindi non abbiamo nessun bisogno di aspettare soldi dall'Unione europea e anche quelli del PNRR sono soldi nostri.

risparmiatori arrivano e comprano tutto quello che c'è da comprare e lo faranno ancora, perché il risparmio degli italiani ammonta, solo in conti, a circa 2.000 miliardi. Figurarsi che problema c'è per comprare le emissioni di quest'anno, che sono pari a 300 miliardi. Signor

consenta ai futuri studenti che studieranno questo periodo, invece di essere umiliati come al solito, di essere orgogliosi dei loro cittadini e dei loro rappresentanti. *(Applausi)*.

siamo rimasti piuttosto perplessi. Intanto desidero garantire al Governo (non c'è la Presidente del Consiglio, ma ci sono autorevoli esponenti del Governo) che l'opposizione non intende fare la guerra all'Italia nel Consiglio europeo; l'opposizione vuole che l'Italia faccia bene e faccia il suo dovere, perché - signor Presidente, tramite lei lo vorrei dire al senatore Claudio Borghi - il rispetto non lo si ottiene solo dicendo dei no, ma anche facendo il proprio dovere, facendo quello che si deve, rispettando gli obblighi internazionali ed essendo seri. *(Applausi)*. Il rispetto si ottiene essendo seri. Non è vero che l'opposizione sta sminuendo l'azione del Governo italiano, voglio rassicurarvi. Noi non stiamo facendo nulla, state facendo tutto da soli, perché siete voi che sulla crisi russa siete stati chiamati il giorno dopo, non siamo noi che vi abbiamo delegittimato. *(Applausi)*. Siete voi che sul MES parlate di pacchetto, non capendo, come vi ha spiegato benissimo il presidente Monti, che il MES fa parte di un percorso verso l'unione bancaria. Come fate, quindi, a chiedere l'unione bancaria e a non ratificare uno strumento che peraltro potrete anche non usare? È questo che mina la credibilità dell'Italia, non l'azione dell'opposizione. *(Applausi)*. Per favore, siamo seri.

portarci il PNRR; non è l'opposizione a dire di presentare REPowerEU; è l'Europa a farlo. È chiaro che è una raccomandazione. Noi tifiamo perché il ministro Fitto lo faccia il prima possibile, ma ancora non è stato fatto. Ministro Fitto, attendiamo l'esito del suo lavoro con pazienza, ma, scusate, non stiamo minando la vostra credibilità dicendo cose che sono scritte nei documenti ufficiali dell'Unione europea. Da ultimo, credo che mini la credibilità

non avete avuto la maggioranza in Commissione sul decreto lavoro; ci sono stati un po' di infortuni mediatici, per cui capisco che ci sia bisogno di caricare un po' la maggioranza. Bisogna però fare attenzione, perché caricare la maggioranza è un problema per tutti noi: non abbiamo bisogno, infatti, che la Presidente del Consiglio si presenti in una veste da capo partito o capo popolo. Sinceramente, presidente Meloni, non mi aspettavo che lei oggi dicesse che finalmente avete cambiato la direzione e avete evitato che qualcheduno, come era in passato, cancellasse i confini nazionali. Non troverà mai nessuna dichiarazione dei Governi precedenti in cui c'è scritto che volevamo cancellare i confini nazionali. *(Applausi)*. Lei non troverà nessuna dichiarazione sul fatto che qualcheduno volesse far entrare soggetti irregolari nell'Unione europea senza nessuna distinzione: questo è ciò che lei ha detto oggi e questa è una caduta di stile senza precedenti da parte di un Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. Nessuno ha mai detto

avete votato persino sulla nipote di Mubarak *(Applausi)*, quindi figuratevi se mi stupisco che abbiate votato l'immunità per Salvini. Non vi preoccupate, lasciate perdere. Mi stupisco molto, però, che lei parli di speronamento - lo ha detto ha detto lei - di una nave italiana. I tribunali italiani l'hanno smentita. Vorrei che lei rispettasse le sentenze dei tribunali italiani, perché nei tribunali italiani questa versione dei fatti è stata smentita *(Applausi)*. Quindi rispettiamo la legge, il Presidente del Consiglio rispetti la legge.

Il nostro vero compito, l'unico modo che abbiamo per dare sollievo al Paese è che venga modificato... Questo è l'impegno che noi chiediamo perché tutto il resto, quello che avete fatto fino a oggi, ce lo dicono i numeri. Quando c'erano 60.000 immigrati irregolari che sbarcavano sulle coste italiane,

le vostre politiche sull'immigrazione. Non è servito il decreto sulle ONG e non sono serviti tutti questi decreti che cancellano la protezione speciale e la protezione umanitaria.

Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, signore e signori Ministri, onorevoli colleghi, è stato estremamente interessante per me ascoltare questo dibattito, perché avevo auspicato che nella risoluzione di maggioranza ci fossero alcuni punti fermi, su aspetti che ritengo imprescindibili, per portare non solo pace e sicurezza in Europa e per superare la tragedia del conflitto in Ucraina, di questa guerra vergognosa, vile, di aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina

presentato - una serie di punti fondamentali, che riguardano il sostegno per tutto il tempo necessario a questo grande popolo, che è il popolo ucraino: un sostegno economico, di ricostruzione, politico e militare; tutto il tempo necessario per creare le condizioni per aprire un tavolo di trattative, in modo serio, obbligando se necessario la controparte, l'aggressore, a sedersi al tavolo delle trattative. Ho ascoltato questo dibattito, aspettando che da parte degli autorevoli colleghi dell'opposizione emergessero anche alcuni timidi accenni ai problemi della giustizia, al problema della deportazione dei minori ucraini, dei bambini ucraini deportati in Russia *(Applausi)*, che emergessero delle voci chiare e forti su alcuni temi che vengono sempre mantenuti quasi in sordina, o di cui quasi si ha pudore a parlare, che invece bisogna denunciare. Sono i temi della congiunzione di intenti fra Russia e Cina, e Cina, della presenza delle forze iraniane e dei droni iraniani contro le popolazioni civili sul teatro di guerra ucraino e della necessità di aiutare l'Ucraina, in base anche a quell'articolo 11 della Costituzione, che viene sempre invocato, giustamente, ma in base al quale siamo un Paese contrario alla guerra per negare per negare la libertà degli altri popoli, non certo per un uso legittimo della forza, come prevede l'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite.

dagli altri Gruppi dell'opposizione. Nella risoluzione della maggioranza c'è una chiara affermazione della necessità della giustizia, non soltanto quella della Corte penale internazionale, che sicuramente è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda però i crimini di aggressione, ci vogliono anche altri sistemi, come probabilmente un tribunale *ad hoc* o un riconoscimento della giurisdizione universale, come il Governo italiano ha cominciato a considerare e a proporre. voglio iniziare ringraziando il presidente Meloni e il Governo, per lo straordinario lavoro fatto a livello internazionale, a tutto campo, in sede europea e in tutti i *forum* multilaterali, per ottenere stima, credibilità e fiducia dai nostri interlocutori. Questa stima, credibilità e fiducia le stiamo ottenendo con la chiave della coerenza. È stato sorprendente ascoltare alcune voci che ci ci criticano per non essere coerenti. Ma come non siamo coerenti? Siamo il partito, la forza politica, la coalizione che nel suo programma elettorale ha detto quello che avrebbe fatto e che ha continuato a farlo anche nei momenti più duri della

della maggioranza, prova ne siano la visita e l'incontro del presidente Meloni con il presidente Macron e addirittura i commenti sui giornali francesi, che non sono necessariamente dalla stessa parte o schierati politicamente a favore dell'Italia. «Le Figaro» e a «Le Monde», per esempio, che hanno dato delle descrizioni molto positive di quello che è avvenuto e dei risultati concreti. Credo che queste cose debbano essere dette chiaramente. È stato riferito prima della necessità di saper dialogare senza complessi, senza sensi di sottomissione, senza paure e cedimenti, quando sono

sia una forma di protezione dell'infanzia, che sradicare la cultura ucraina e russificare l'Ucraina significa integrare ed educare. Ci sono purtroppo, anche in Europa e anche nel nostro mondo politico italiano, delle voci che sembrano riflettere questi elementi di disinformazione e di propaganda. Vorrei menzionare due cose in particolare: la prospettiva dell'Ucraina nell'UE e l'avvicinamento e l'ancoraggio dell'Ucraina alla NATO. La prima dimensione è di estrema importanza ed è stata sottolineata dal presidente Meloni anche in recenti occasioni, nell'affermare la necessità dell'impegno dell'Italia per favorire questo percorso in tempi ragionevolmente rapidi, naturalmente riferiti anche ad altri Paesi che sono in attesa di avere il riconoscimento di membro a parte intera dell'Unione europea.

quando ha ricordato che, dei sette capitoli aperti in tema di riforme fra Unione europea ed Ucraina, due sono stati risolti e cinque stanno progredendo. Devo dire che su questi temi, anche come parte della Commissione politiche dell'Unione europea, riscontro negli interlocutori diversi altri Stati membri un grande apprezzamento per il lavoro dell'Italia, a tutto campo, sui temi economici, sui temi della *governance*, ma anche e soprattutto sui temi della sicurezza e del superamento di questa congiuntura. Devo ringraziare, per parte del del lavoro parlamentare che stiamo facendo, il sostegno e l'attenzione che il ministro Fitto riserva al lavoro delle Commissioni parlamentari

di negazione di quello che avviene da parte di alcuni settori delle nostre forze politiche, gli sbagli che sono stati fatti nel rapporto con la Cina.

di anni fa, chiamata «Lo Xinjiang è una terra meravigliosa», promossa dall'ambasciata cinese a Roma, con il vice governatore dello Xinjiang Manlik Siyit e autorevoli esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. L'obiettivo della conferenza era spiegare la corretta strategia del governo cinese in Xinjiang, nonché le sue politiche a beneficio del popolo. È stata una disinformazione puntuale e voluta, alla quale hanno presenziato autorevoli esponenti delle forze politiche dell'opposizione Qui viene da pensare, quando si parla di armonia, solidarietà e stabilità della Cina e dello Xinjiang, ai problemi del lavoro forzato e alle violazioni pesanti dei diritti umani. Viene veramente da pensare

sempre più problematico proprio per l'apporto pesante che sta dando alle operazioni militari russe in Ucraina.

come molte materie e di rilevante complessità riguarderà il Consiglio europeo di domani e di dopodomani. Ovviamente ringrazio per i numerosi spunti e mi limiterò, come sempre evitando di ripetermi, alle questioni sulle quali posso fornire un punto di vista ulteriore e a quelle che non condivido. Ho sentito molti interventi

È ricorrente la questione della riforma della *governance*, il Patto di stabilità e crescita, è ricorrente il tema del PNRR ed è ricorrente il tema del MES. In particolare, il senatore Misiani mette insieme giustamente le tre cose, dicendosi d'accordo - come anch'io credo - sul fatto che non si possa e non si debba tornare alle regole del vecchio Patto di stabilità. Dicevo stamattina e sono convinta che quella sulla riforma della *governance* europea in tema di stabilità e crescita sia una di quelle materie sulle quali ragionevolmente, anche in passato, le posizioni del Parlamento sono state più ampie di quelle delle singole maggioranze. Spero che sarà così anche in questo caso. Ovviamente tutti ci rendiamo conto di come le future regole della *governance* debbano essere orientate soprattutto a garantire la crescita, senza la quale - come dicevo - è anche molto più difficile

degli investimenti che siamo chiamati a fare, particolarmente noi italiani, particolarmente con il PNRR, particolarmente sulle grandi scelte strategiche che l'Europa si è data: transizione verde, transizione digitale (poi tornerò anche sul tema della difesa), che vengono in qualche maniera protette dalla *governance*. Su questo siamo d'accordo. Dopodiché, però, il senatore Misiani ci dice che ci sono due convitati di pietra che rendono sostanzialmente difficile per l'Italia portare avanti questa trattativa, che sono la lentezza e i ritardi sul PNRR e la mancata ratifica del trattato di modifica del MES. Non sono d'accordo ovviamente, senatore Misiani. Non sono d'accordo, intanto perché - mi perdoni il senatore Misiani - a monte c'è un racconto che non corrisponde a verità. Ci si dice che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta. Temo che non si sia molto preparati, perché sono molti e copiosi i documenti che noi abbiamo prodotto per la Commissione europea, per essere precisi rispetto ai tempi di attuazione di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che non avevamo scritto noi e rispetto al quale le contestazioni che vengono fatte dalla Commissione non sono riferibili a noi. Potrei citarle lo stadio di Firenze, che la Commissione dice che non ritiene debba essere finanziato con i soldi del Piano nazionale di ripresa resilienza, ma non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. *(Applausi)*. Semmai, noi stiamo producendo molte carte cercando ovviamente di dare continuità, per quello che possiamo fare, a un Piano del quale non avevamo la responsabilità. Questo per quello che riguarda il passato. Senatore Misiani, anche sul tema della trasparenza

Anche sulla modifica del REPower EU chiaramente vogliamo coinvolgere il Parlamento, poiché sono materie strategiche sulle quali è giusto che ci sia una convergenza. Sono contenta che oggi vogliate il Parlamento centrale rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché ricordo quando il Piano fu approvato dal Parlamento: un documento di 370 pagine che era stato consegnato alle Camere un'ora prima dell'inizio della discussione. Sono cose che non abbiamo condiviso in passato e che non intendiamo ripetere. Dopodiché, lei, senatore, dice che siamo in ritardo sul futuro e cita la Germania e il Lussemburgo, che hanno già presentato i loro progetti, nonché la Francia e Malta. e Malta. Il senatore Misiani è una persona molto preparata e conosce la differenza tra quello di cui ha parlato e il caso italiano, quindi sa benissimo che, per ciò che concerne Germania e Lussemburgo, parliamo solamente di una modifica di Piani nazionali che sono infinitamente più piccoli del nostro: il Piano tedesco, se non vado errata, si aggira intorno ai 27 miliardi e non devo ricordare io a questo Parlamento che il Piano italiano investe complessivamente 190 miliardi, più i 30 italiani; insomma è un Piano un tantino più corposo. Malta e Francia sono le due Nazioni che finora hanno presentato una modifica che coinvolge il REPower EU, che è un Piano nuovo: anche questo dovremmo saperlo, così come dovremmo sapere che la scadenza per la presentazione di quel Piano è il 31 agosto. Essendo il Piano italiano il più complesso di tutti, anche per non dover poi ritrovarci a modificare in corsa le cose che erano state inserite nel PNRR, è bene che questo lavoro si faccia con serietà. Quindi non ci sono ritardi, ma c'è semplicemente un lavoro serio che stiamo cercando di fare. Lo dico senza fare polemica, colleghi; avremmo potuto fare polemica, invece non abbiamo fatto polemiche, ci siamo messi ai remi e abbiamo cominciato a lavorare per mandare avanti un Piano che è importante per l'Italia anche sugli aspetti che potevamo non condividere complessivamente, perché quando si tratta di interesse nazionale noi

e che, in alcuni casi, richiede da parte della Commissione europea delle modifiche, siano anche quelli che se la prendono con l'attuale Governo. Mi fa specie, come pure - e lo dico - mi fa specie che lo faccia il commissario Gentiloni, che immagino quel Piano lo abbia letto prima e oggi chiama in causa il Governo italiano, dicendo che bisogna correre e fare di più. Insomma, se si fosse vigilato un po' di più in passato, probabilmente oggi si farebbe più velocemente. Per quello che riguarda il MES, così rispondo anche al senatore Monti, che ringrazio, sul tema della logica di pacchetto, torno su quello che diceva sempre il senatore Misiani:

Il meccanismo europeo di stabilità richiama però i parametri del precedente Patto di stabilità al suo interno, quindi, da una parte, si dice che non dobbiamo tornare ai vecchi parametri del Patto di stabilità, e, dall'altra, si chiede, prima di vedere quali siano i nuovi parametri del Patto di stabilità, di ratificare un trattato che prevede i vecchi parametri del Patto di stabilità. Temo che questo sia uno dei tanti elementi che dimostrano come le cose vadano valutate nella loro interezza, nella loro interezza, anche per una questione di equilibrio e di maggiore chiarezza su quello che si sta approvando. Dopodiché, la collega Rojc parlava di immigrazione e di corridoi umanitari. Collega Rojc, temo che il tema dei corridoi umanitari sia un tantino in contrapposizione con la politica delle porte aperte che si è fatta in questi anni. È proprio questo il tema che cerco di segnalare, così come un'immigrazione regolare, purtroppo, è più difficilmente compatibile con la politica delle porte aperte; tant'è che, negli anni nei quali c'erano altri al Governo, i decreti flussi, con i quali si normano

secondo la protezione internazionale, la convenzione di Ginevra e la protezione sussidiaria dell'Unione europea, e chi non vi ha diritto, perché migrante economico e dunque va gestito e affrontato in maniera completamente diversa, noi non aiuteremo davvero chi ha maggiore bisogno e diritto a essere aiutato. È esattamente questa distinzione che stiamo cercando

di fortuna persone che troppo spesso periscono nel Mediterraneo.

apriamo il nostro dibattito e la nostra attenzione, per esempio, alla Moldova o ad altre Nazioni, non dobbiamo dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimanga indietro. Non ci sono corsie preferenziali, né ovviamente trattamenti diversi e non ci devono essere, soprattutto per rispetto ai Balcani occidentali, materia che - insisto - l'Italia è forse una delle Nazioni che in Europa

e prudenza, perché considero la fermezza come la principale forma di prudenza che si possa mettere in campo. Su questo voglio citare diversi interventi che ho sentito. Ribadisco che, quando si parla di pace, immagino che nessuno in cuor proprio, in quest'Aula, pensi che la guerra piaccia o piaccia o voglia alimentare la guerra perché si diverte in un conflitto. Siamo tutti d'accordo sulla pace, il punto sul quale non siamo d'accordo e come ci si arrivi. a questo che non capisco alcuni interventi e non mi riferisco, ovviamente, a quello del senatore Paganella, che ho condiviso, ma a quello del senatore Lorefice. Ho detto e ribadisco, quando mi si chiede di lavorare sulla pace, che ad oggi, a condizioni date, il modo più efficace di favorire la fine del conflitto e l'apertura di un tavolo negoziale è sostenere l'Ucraina è sostenere l'Ucraina e questo, colleghi, perché - l'ho detto e ribadito cento volte - l'unico elemento che può costringere in un conflitto le parti a mettersi intorno a un tavolo è l'equilibrio delle forze in campo, lo stallo. Se non avessimo sostenuto gli ucraini, non avremmo avuto bisogno di parlare di niente, ma non perché avremmo avuto la pace, bensì perché avremmo avuto un'invasione.

nella risoluzione del MoVimento 5 Stelle c'è scritto che non bisogna mandare armi all'Ucraina e questo è un fatto. E allora il tema non è più la pace, perché, collega Lorefice - lo chiedo a lei e spero che mi risponda chi farà la dichiarazione di voto - se dovessimo smettere di sostenere l'Ucraina - ammesso che ci seguissero anche i nostri *partner*, che non ci seguirebbero - sa dirmi che cosa accadrebbe? Lei pensa che si aprirebbe un tavolo negoziale, nel momento in cui l'Ucraina fosse più debole?

Purtroppo questo è il pensiero che il generico riferimento alla pace sottintende. L'ho detto stamattina e lo ripeto anche a voi, perché spero che almeno in questa dichiarazione di voto del MoVimento 5 Stelle qualcuno mi risponda. Ho visto un'intervista del professor De Masi, filosofo di riferimento del MoVimento 5 Stelle, che diceva che è meglio vivere sotto una dittatura, piuttosto che morire. Posso sapere da chi interviene in dichiarazione di voto se condivide queste parole? Voi capite bene come questa sorta di esegesi della vigliaccheria di fatto faccia strage di secoli di civiltà europea e di battaglie di gente che ha dato la vita per difendere la libertà, la democrazia e i valori che sono della nostra civiltà. Voglio sapere se siete d'accordo o meno. Voglio sapere se ritenete che Paolo Borsellino dovesse preferire vivere piegandosi alla mafia piuttosto che fare le battaglie che ha combattuto. Non si può sostenere in coscienza una frase del genere. *(Applausi)*. E se non siete d'accordo, sono contenta e mi aspetto che lo diciate. *(Applausi)*. Mi aspetto che lo diciate, perché le cose vanno chiamate con il loro nome, signori; non vanno chiamate in un altro modo. Io sono una persona da sempre abituata ad assumersi le proprie responsabilità, anche quando c'erano da dire cose scomode, che si possono dire, basta che si metta la faccia.

che vuol dire rafforzare le proprie catene di approvvigionamento, quando si vuole fare la transizione verde, per non passare da una dipendenza dalla Russia a una dalla Cina, e vuol dire rafforzare la propria tecnologia digitale e la propria difesa.

Sa che cosa mi colpisce? Che solitamente coloro che si scagliano contro gli investimenti sulla difesa sono anche quelli che poi denunciano un'eccessiva ingerenza - per esempio, degli Stati Uniti - nelle scelte di politica estera europea. Le due cose non stanno insieme, collega Lorefice *(Applausi)*, perché se chiedi a qualcun altro di difenderti devi anche sapere che probabilmente non lo farà gratis e avrai maggiori difficoltà a difendere i tuoi interessi. Quindi, sì, autonomia strategica: quello nella difesa è un investimento nell'autonomia politica della Nazione e dell'Europa.

Collega Monti, nel ringraziarla, al netto della vicenda del MES e della questione del pacchetto, ho qualcosa da dire. Sul tema dell'equilibrio di bilancio la ringrazio, ma non credo che si possa dire davvero che ci sono componenti della maggioranza riluttanti rispetto a una seria politica di bilancio. Sono riluttanti, lo sono stati come sono come sono stata critica anch'io si sa - verso le politiche di austerità, ma sono due cose diverse, tant'è che stamattina dicevo che sono finite le politiche di austerità, ma questo non vuol dire non essere seri anche rispetto al modo in cui ci si pone all'estero. Anche da grande contestatrice dell'austerità, mi sono ritrovata in passato a segnalare che alcuni provvedimenti che i Governi avevano adottato, di spesa molto allegra e poco produttiva, non ci hanno aiutato nelle nelle contrattazioni che andavano fatte. Condivido invece pienamente il tema del rapporto, all'interno del mercato unico, con gli interessi delle altre Nazioni europee.

nel quale però c'è una cosa che questo Governo ha chiesto con forza in risposta a chi chiedeva un allentamento degli aiuti di Stato per rispondere all'*inflation reduction act*, senza porsi sufficientemente il problema che questo avrebbe creato una disparità tra Paesi che avevano un maggiore spazio fiscale e Paesi che non ne avevano, né il problema si poteva risolvere a monte con il fondo sovrano, perché conosciamo il tema un fondo sovrano richiede molti mesi di contrattazione, se non anni, quindi non saremmo stati in grado di competere nel momento in cui si allentavano le norme sugli aiuti di Stato. Come tutti sanno, abbiamo chiesto piena flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti,

a essere assertivi sui tavoli competenti, ma mi sembra che in questa fase il Governo abbia lavorato per difendere l'interesse italiano e fare del suo meglio anche per garantire il mercato unico

Non è vero che la Tunisia ci ha sbattuto la porta in faccia; è vero che c'è una trattativa in corso; è vero che è già stata firmata una dichiarazione congiunta, obiettivo che non era scontato; è vero che adesso si sta lavorando per arrivare a una iniziativa a una iniziativa più sostanziosa. Io non voglio dare tempi rispetto a quando questo accadrà, ma continuiamo a lavorare e mi sembra che si facciano passi in avanti molto significativi. Desidero anche dire che non è vero che noi abbiamo chiesto al presidente Saïed di fare in buona sostanza il gendarme dei migranti per qualche milione di euro; non è questo l'approccio che si vedrà, quando questo lavoro dovesse andare avanti. L'approccio che si vedrà è proprio quello sul quale stiamo lavorando con la Commissione e ovviamente, da una parte, affronta la questione dei migranti, ma dall'altra parla soprattutto di investimenti, di sviluppo e di aiutare

vada dato atto al lavoro che il Governo italiano ha fatto da questo punto di vista, dal suo arrivo ad oggi, nel riaprire anche un dialogo che sta diventando quotidiano

sono venuti con me in Tunisia in una missione che era europea è perché tutti si rendano conto di un tema che è molto strategico. Dico con garbo e sottovoce che, a mio avviso, il Governo italiano in questo ha avuto un ruolo non secondario.

in Africa, di cui ho parlato lungamente, debba essere strutturale e debba richiedere risorse adeguate. È esattamente il lavoro che stiamo facendo, colleghi. Adesso si apre il tema del bilancio pluriennale dell'Unione europea, l'Italia ha mandato il suo documento di posizionamento e stamattina

con i Paesi africani, che secondo me può essere strategica - come dicevo - con il piano Mattei per l'Africa. Mi dispiace che in questa sede si riesca a fare polemica anche su un progetto

Ci sarà una ragione per la quale noi, in questi anni, abbiamo speso moltissime risorse per la cooperazione, in centinaia o in migliaia di microprogetti, e quelle risorse non sono riuscite a rendere adeguatamente in termini di stabilità, di crescita e di sviluppo dei Paesi africani. Forse bisogna concentrarsi su un progetto strategico e ci sono alcune questioni strategiche che possono mettere in collegamento gli interessi europei con quelli africani. La cooperazione seria si fa così: la cooperazione seria si fa da pari a pari, si fa quando le Nazioni condividono scelte strategiche e si legano grazie a progetti che non sono uno *spot*, ma diventano strutturali. È esattamente quello che tentiamo di fare con il tema del piano Mattei per l'Africa, che non è una cosa che possiamo o vogliamo fare da soli. Si un progetto pionieristico, sul quale cerchiamo di coinvolgere l'intera Unione europea, perché, per esempio, come ho detto anche in questa sede diverse volte, l'Africa è potenzialmente un enorme produttore di energia e, segnatamente, di energia pulita. L'Europa oggi ha un problema di approvvigionamento energetico non irrilevante. Le due cose possono essere messe insieme in un progetto strategico? Assolutamente sì. Possiamo, con adeguati investimenti, con un po' di intelligenza, con un po' di visione e con progetti che non si fermano dopo tre o sei mesi, aiutare finalmente l'Africa a vivere delle risorse delle quali dispone,

può far crescere i suoi interessi strategici, la sua economia e il suo benessere. Noi possiamo, per la parte che non serve all'Africa, approvvigionarci, perché abbiamo un problema di approvvigionamento, che in particolare c'è nel Centro-Nord L'Italia può essere particolarmente interessata, banalmente, perché è la porta. E allora, piano Mattei per l'Africa sia! Lo dicevo stamattina: c'è una serie di progetti che è già sul campo. Li presenteremo in autunno, definitivamente:

collegamento elettrico con la Tunisia, per cui sono stati sbloccati i finanziamenti, o come il SoutH2 Corridor. Ci sono diverse questioni infrastrutturali sulle quali lavoriamo, perché senza le infrastrutture di collegamento tutto questo funziona e non si realizza. Poi, certamente, se si pensa che un progetto del genere possa essere realizzato in sei mesi, si capisce la differenza, tra me e chi lo sostiene, su cosa sia un progetto strategico.

vinciamo solo perché siamo uniti, mentre gli avversari sono divisi. In Molise non mi è sembrato che sia andata così, onorevole

alla Belt and road initiative, collega Borghi, lei sa bene che l'adesione alla Nuova via della seta non è stata una decisione dell'attuale Governo e credo ricordi anche quale fosse, al tempo, la posizione della sottoscritta. Ritengo che, come ho affermato e come ribadisco, si possano avere ottime relazioni con la Cina senza per questo partecipare a un progetto e far parte di un piano strategico. Del resto, una cosa che mi ha colpito molto è che, per paradosso, noi siamo l'unica Nazione l'unica Nazione in Europa che sta all'interno della via della seta, ma non siamo affatto la Nazione che ha il maggiore ritorno nel commercio e nei rapporti con la Cina. Questo è davvero un paradosso. le valutazioni sono in corso e c'è ancora tempo per modificare la decisione; credo la questione vada maneggiata con delicatezza, con cura e con rispetto,

ma per trovare soluzioni che siano le più valide possibili nella difesa dei nostri interessi nazionali. Qualcuno - mi dispiace, non ho segnato il nome e non lo ricordo relativamente al patto di migrazione e asilo, del quale ho ampiamente parlato questa mattina, diceva che in realtà è un compromesso al ribasso e che la ragione per la quale non abbiamo potuto fare di più è che - tema ricorrente - siamo collegati e amici dell'Ungheria di Orban. Mi corre l'obbligo di segnalare ai colleghi che l'Ungheria ha votato contro il patto di migrazione e asilo, mentre noi abbiamo votato a favore, perché in questa Nazione oggi c'è qualcuno che non decide in base a quello che gli viene indicato da altre Nazioni, ma al proprio interesse nazionale. *(Applausi)*. Se io sono d'accordo, sono d'accordo; se non sono d'accordo, non sono d'accordo. degli Stati nazionali non si legge con una lente così schematica. Del resto, chi conosce un po' la politica europea ed è abituato a conoscere il tema più di quanto la propaganda a volte imponga sa benissimo che all'interno del Consiglio europeo le alleanze sono variabili,

di perseguire la politica a livello internazionale. Per questo oggi così faccio e per questo ieri contestavo chi mi sembrava che facesse più quello che dicevano i suoi alleati politici che non quello che fosse di interesse per la propria Nazione; non ero d'accordo e l'ho detto tante volte. *(Applausi)*. Dopodiché - e con questo mi pare di aver concluso

che vengono discusse al Consiglio europeo e che vengono discusse in Europa, cioè che c'è una preminenza della difesa dell'interesse nazionale rispetto al nostro legittimo dibattito politico interno. Però, guardi, le voglio citare una cosa che accadeva qui questa mattina, che mi aveva dato della vecchia: com'era? Nicita. No, scherzo, collega: era una battuta, ma avevo letto la cosa politica. Gli avevo promesso una risposta, perché il collega Nicita stamattina, parlando di altro (non era in questo dibattito, ma, insomma,

ammetto che nel merito, se la Commissione europea non è intervenuta fino a adesso sulla RAI, difficilmente interverrà. Cioè, se non è intervenuta quando, per la prima volta nella storia d'Italia, nel consiglio di amministrazione della RAI non era rappresentata l'unica opposizione esistente al Governo della Nazione *(Applausi)*, difficilmente lo farà adesso perché si è cambiata la *governance* della RAI, ma non è questo il tema che mi interessa. è che questo tema dello Stato di diritto lo sento tornare spesso, da parte di esponenti della sinistra di vario genere, parlamentari e opinionisti, e a me - lo dico con onestà, colleghi - suona come un incitamento alla Commissione europea. È come se una parte della sinistra,

Voi vi rendete conto di quanto questo sarebbe grave? Vi rendete conto di quanto sarebbe grave chiedere un intervento esterno, bloccando all'Italia le sue risorse e i suoi diritti, semplicemente perché non si è in grado di battere questo Governo facendo opposizione? *(Applausi)*. È su queste cose che bisogna capirci. È su queste cose che secondo me, colleghi, si supera il limite,

mi ero appassionata nella replica, ma non mi vedrete mai paludata, come magari vi aspettereste. *(Applausi)*. Penso che dovrò preoccuparmi di più quando non riuscirò a mettere la stessa passione in quello che faccio. Ci divideremo sempre e, per carità, non mi si può dire né potrei mai chiederlo io - che non ho fatto sconti dall'opposizione - di non fare l'opposizione come va fatta e come ritengo che vada fatta, con decisione, senza peli sulla lingua. Non lo chiederei mai.

Chiedo al ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

e della direzione che il Governo Meloni percorre nel solco del più alto interesse nazionale e del rispetto del mandato elettorale, a differenza di chi poche ore fa in quest'Aula invece ha esaltato Carola Rackete,

Anche in quest'occasione, nel Consiglio europeo di domani, l'Italia, diversamente dal passato, si appresta ad essere rappresentata ai tavoli europei in un modo diverso, a cui non eravamo più abituati da diversi anni, fatto di concretezza e di carattere politico, che rispecchia fedelmente le aspettative che milioni di italiani hanno riposto nel programma della coalizione

a quella delle opposizioni. Signor Presidente, grazie finalmente ad un Governo politico, oggi possiamo andare in Europa con la testa alta e la schiena dritta, senza servilismi, non sbattendo sterilmente i pugni sul tavolo, ma affermando con pragmatico buon senso le solide ragioni del nostro interesse nazionale su tutti i *dossier* e gli argomenti all'ordine del giorno. Voglio quindi aprire questo mio intervento con un ringraziamento, non certo formale, al Presidente del Consiglio per averci testimoniato con le sue comunicazioni una vera passione per l'Italia, anche rivendicata poc'anzi, e l'impegno del Governo alla ricerca di soluzioni vere alle enormi sfide che stanno attraversando il nostro Paese e l'intera Europa. Stiamo parlando di sfide epocali su temi estremamente complessi. Mi riferisco cioè alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, alla politica industriale dell'Unione europea e alla crescita, al mercato unico e alla competitività delle imprese, alla sicurezza e alla difesa europea, alle questioni riguardanti le migrazioni e le relazioni esterne. In merito a questi *dossier* fondamentali, il nostro Paese, tornato di nuovo protagonista dell'iniziativa politica europea, è destinato giocoforza a recuperare centralità nello scacchiere mediterraneo, grazie alla determinazione e alla credibilità che il presidente Meloni, dall'inizio del suo mandato, anche per esempio con l'idea del piano Mattei, poc'anzi citato, è riuscita a rivendicare a livello comunitario e internazionale. La nostra vocazione atlantista, la nostra immagine e la nostra autorevolezza internazionale, la nostra lealtà rispetto agli impegni assunti e la nostra coerenza non solo vengono confermate al più alto livello, ma addirittura si rafforzano con atti e provvedimenti parlamentari univoci di una coalizione compatta e senza grigie ed opache zone d'ombra. Collega Spagnolli - anche se non ci si deve rivolgere all'Assemblea e ai colleghi - voglio ricordarle che lei parla della nostra unità di coalizione come unico valore di vittoria, quando è stato eletto sindaco solo grazie alla parte tedesca della mia città che le ha dato il consenso, altrimenti non sarebbe mai stato eletto. Tutto questo si traduce - diciamocelo chiaramente - anche per noi in un vantaggio concreto, perché è sotto gli occhi di tutti come la nostra ritrovata affidabilità istituzionale spinga i *partner* dell'Unione europea, nonostante gli auspici delle opposizioni, a dimostrare in concreto maggiore disponibilità nei nostri confronti e ad affiancarci e sostenerci nel fronteggiare le drammatiche emergenze economiche o

essere messi al margine dell'Europa. Era questo forse il vostro auspicio. Non tocca certamente a me ricordare quanto sia stato difficile per l'Italia, negli anni scorsi, praticamente abbandonata nella gestione dei flussi migratori, fare di questa emergenza, che il presidente Meloni ha definito strutturale, ed è vero, una priorità dell'agenda europea. A qualche collega voglio ricordare che, sì, è vero purtroppo noi abbiamo attratto l'immigrazione soprattutto con certe cooperative. E non voglio qui stare a ricordare, solo per dignità umana, la cooperativa del collega della Camera Soumahoro, Per lunghi anni, l'*affaire* immigrazione è stato solo e soltanto un problema cinicamente scaricato sull'Italia. Oggi comincia, viceversa, un nuovo cammino. I primi risultati si possono già vedere. Le conclusioni assunte nelle sedi degli altri Consigli sono state alla base della presentazione, da parte della Commissione europea, di un nuovo piano piano per la gestione delle frontiere esterne europee, in particolare con riferimento al Mediterraneo centrale. Concordiamo, quindi, con la visione che il nostro Primo Ministro ha espresso, in questa sede ed anche in occasione dei recenti bilaterali con la Francia e la Germania: è centrale il partenariato con il Mediterraneo, non solo con il Nord Africa, con particolare riferimento a Tunisia e Libia. Come non possiamo che condividere l'intesa avuta recentemente con la presidente del Parlamento europeo Metsola, secondo cui la priorità va data alla difesa dei confini e, in tale ottica, alla dimensione esterna, a partire dall'intesa UE con la la Tunisia, che è perfettamente riuscita. Tragedie come quella di Cutro e purtroppo, recentemente, anche quella consumatosi al largo delle coste della Grecia, che il presidente Meloni, con la consueta umanità, ha ricordato, ci insegnano che i flussi migratori non sono e non possono essere un problema solo ed esclusivamente dell'Italia, come qualcuno vorrebbe. Un adeguato bilanciamento fra i principi di solidarietà e responsabilità deve continuare ad essere quel *fil rouge* capace di unire e non certo dividere, per garantire la sicurezza della nostra Nazione, che ci ha reso tanto amati all'estero. Perché sicurezza non è arroccamento. Fermezza non è disumanità. È piuttosto l'accoglienza illimitata e non dignitosa ad essere disumana e rinnovo, appunto, il riferimento alla cooperativa di Soumahoro. La sicurezza, al contrario, ha a che fare con la certezza di valori economici, sociali, culturali, politici, geopolitici, che sono la forza di un'identità che non vive sulla difensiva, Italia ed Europa, ma vive nella visione dello sviluppo: uno sviluppo che si crea nel solco della civiltà europea con un nuovo paradigma, basato non più sullo scontro di civiltà, ma sulla cooperazione, lavorando sulla dimensione esterna. Tradotto in politiche vuol dire che, al contrasto all'immigrazione illegale, occorre sempre affiancare un'azione concreta, lungimirante e coraggiosa, di promozione, per esempio, dell'immigrazione legale. Una maggiore collaborazione con i Paesi di origine e di transito assicurerà di poter prevenire il traffico illecito dei migranti. Per questo fa bene e ci rende orgogliosi il presidente Meloni a richiamare gli organismi dell'Unione europea ad agire secondo meccanismi di concreta solidarietà e condivisione e a non soggiacere a velati ricatti. Siamo fieri del lavoro che è stato fatto finora, presidente Meloni, ma non basta e lo sappiamo. Per questo auspichiamo che, nell'imminente Consiglio europeo, si facciano significativi passi avanti. Non vogliamo che nel Mediterraneo la speranza di chi parte si trasformi in sonno eterno per mano degli scafisti senza scrupoli, gestori di un *business* spietato che gioca d'azzardo con la vita di migliaia di persone. L'Europa tutta deve assumersi impegni, essere più Grazie a tutti e una scia di morte e di distruzione. Su questo conflitto non ci sono e non ci possono essere dubbi di sorta. Per la maggioranza che sostiene questo Governo è ben chiaro chi sia l'aggressore e chi sia l'aggredito; chi ha violato le regole del diritto internazionale e chi sta esercitando il sacrosanto diritto alla difesa del territorio nazionale e delle proprie libertà, che non vanno mai date per scontate. L'Italia, come membro dell'Alleanza atlantica, non farà mai venire meno il sostegno economico, militare ed umanitario finché lo scenario bellico lo richiederà. Al tempo stesso, riteniamo che l'Europa, nel suo insieme, debba farsi carico di individuare e aprire percorsi che possano far intravedere la possibilità di un cessate il fuoco senza piegare la testa. Il presidente Meloni ha citato Borsellino. Io posso citare una celebre frase di Giovanni Falcone, che tutti dovremmo ricordare in quest'Aula. Come ben definito nella risoluzione di maggioranza, va riaffermato il principio che per raggiungere una condizione di pace durevole è essenziale aprire una mediazione tra le due parti in conflitto e che l'unica via per evitare ulteriori sofferenze al popolo ucraino è l'immediato cessate il fuoco, in preparazione di una pace giusta basata sul ripristino della legalità internazionale. L'Italia non può abdicare al suo tradizionale ruolo di esportatore di pace, come ci insegna appunto Papa Francesco.

contrario e lei lo ha detto in maniera inequivocabile. Se non avessimo aiutato gli ucraini, oggi vivremmo in un mondo molto più insicuro, con una guerra molto più vicina a casa nostra, in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte. A chi conviene un mondo così? Vorrei che qualche collega dell'opposizione rispondesse. Colleghi, il caos sul fronte russo cui abbiamo assistito nelle ultime ore, con un tentato *putsch* che ci farebbe probabilmente cadere dalla padella alla brace, non può che confermare che stiamo dalla parte giusta e che quella intrapresa è la giusta direzione.

Presidente, affronterò innanzitutto due argomenti toccati nelle comunicazioni della presidente Meloni, ovvero l'immigrazione e la guerra. Devo dire subito che nelle argomentazioni sull'immigrazione che ho ascoltato non c'è, dal mio punto di vista, nulla di nuovo. La difesa dei cosiddetti confini esterni sarebbe stata assunta come priorità dall'intera Europa, grazie alle pressioni del Governo italiano. A queste parole, però, poi seguono i fatti, che purtroppo sono quelli che abbiamo visto. Sono purtroppo l'ennesima strage nella quale sono morte 600 persone due settimane fa al largo delle coste greche, la più grave strage degli ultimi decenni, successiva di poche settimane a quella di Cutro. Vorrei quindi chiedere alla Presidente del Consiglio cosa significa esattamente "difesa dei confini esterni": guardare da un'altra parte mentre i barconi affondano? Mantenere e anzi rafforzare le condizioni che già fanno del Mediterraneo un immenso cimitero? E poi difesa da chi? Dalle persone che scappano? Dalle donne e dai bambini ci dobbiamo difendere? È certamente giusto coinvolgere l'Europa, ma credo con un obiettivo opposto, l'abbiamo detto tante volte e lo dico anche stasera: serve e non è più rinviabile una grande missione europea come fu Mare Nostrum. *(Applausi)*. È fondamentale coinvolgere l'Europa, ma per costruire canali di accesso legali e io penso che l'unica strada concreta e realistica per contrastare l'immigrazione clandestina sarebbe soltanto questa, evitando peraltro lo dico alla Presidente del Consiglio - questa sorta di criminalizzazione che ho sentito anche stasera dei migranti economici, come se la fame, la sete o i cambiamenti climatici non fossero essi stessi motivi sufficienti per scappare e per migrare. Anche sulla guerra devo dire che la posizione del Governo italiano è quella di sempre, la più estrema che c'è nell'Europa occidentale. stati liquidati, peraltro, in poche parole dalla Presidente del Consiglio anche gli ultimi recenti eventi di pochi giorni fa, quando una compagnia di ventura decisamente famigerata era a 200 chilometri dalla capitale dello Stato con il più folto arsenale nucleare del mondo. Ebbene, mi sembrerebbe sufficiente per dire quanto alto sia il rischio di una

qualche giorno fa è quello che tutti gli analisti, compresi quelli del Pentagono, considerano il più pericoloso, e cioè, l'implosione di una delle principali potenze nucleari del mondo, l'eventualità di una Federazione Russa frammentata e contesa da diversi signori della guerra. Chiariamoci, l'abbiamo detto tante volte: qui non si tratta certamente di voler difendere Putin, peraltro fino a ieri alleato con la Wagner; noi ci auguravamo la caduta di Putin molto prima di chiunque altro in questo Parlamento *(Applausi)*, e anzi ne denunciavamo la sua ispirazione antidemocratica quando tanti di voi, oggi al Governo del Paese, lo lusingavano. Ci auguriamo la caduta di Putin perché al suo posto si affermi una Federazione Russa democratica, pacifica e solida, non perché quel Paese diventi il campo di battaglia per eserciti rapaci, armati da ordigni nucleari. Non è evidentemente questa la sola minaccia innescata dalla guerra: gli allarmi nucleari sono all'ordine del giorno, da Taiwan alla frontiera tra le due Coree; i focolai di tensione che potrebbero sfociare in una guerra totale si moltiplicano, e qui naturalmente nessuno contesta

la situazione che abbiamo denunciato fin dall'inizio della guerra, pur indicando, per l'appunto, senza ambiguità, le responsabilità dell'aggressione. Sto parlando del rischio di una *escalation* i cui effetti si diffonderebbero sull'intero pianeta. Il punto, Presidente, è che l'Europa non sta facendo nulla per provare a porre fine alla guerra. Se si insiste nel confondere la pace con la sconfitta militare della Russia e se pensiamo che tutto vada risolto sui campi di battaglia e non sui tavoli di trattativa, ci comportiamo esattamente come quei sonnambuli che già una volta nel 1914 portarono l'Europa e il mondo nell'abisso. Dicevano esattamente le stesse cose che dite voi oggi. *(Applausi)*. Abbiamo addirittura sentito qualche giorno fa che il cessate il fuoco sarebbe un errore e un vantaggio per Putin. Penso invece che il cessate il fuoco debba essere il primo obiettivo per cui dovrebbe spendersi l'Italia, perché è evidentemente condizione essenziale per intavolare possibili trattative di pace; dovrebbe levarsi una voce diversa dal solo rullare dei tamburi di guerra. Quella voce, fatti salvi i tentativi, a mio avviso straordinari e preziosi, della Santa Sede, potrebbe e dovrebbe provenire solo dall'Europa, che invece non è mai apparsa così marginale. E il compito dell'Italia dovrebbe essere esattamente quello di spingere l'Unione europea in quella direzione, e invece ci distinguiamo per le posizioni più estreme e più radicali tra i Paesi occidentali. Inviare armi sempre più potenti non significa difendere l'Ucraina, ma significa spingere il mondo verso il precipizio, innalzare le spese militari sino al 2 per cento del PIL, il che equivale a dire che la diplomazia passa solo per le armi, destinare i fondi del PNRR alla produzione di munizioni significa lanciare davvero un messaggio devastante. Vorrei dire con grande chiarezza che non basta nascondersi dietro l'impegno a non adoperare in Italia le risorse del del PNRR, non solo perché spesso gli impegni lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto perché alle parole bisognerebbe essere conseguenti con i fatti. A Strasburgo bisogna avere il coraggio di votare contro quelle scelte che sono pericolose, miopi e drammaticamente dannose. Avrei ancora tre argomenti da trattare ma ne cito solo una per concludere. economia davvero in poche battute. Lei, Presidente, parla di rialzo dei tassi, ma se fosse conseguente rispetto alle critiche alla BCE, dovrebbe fare solo una cosa: tassare gli extra profitti delle banche, delle aziende, delle società energetiche che in questi anni si sono enormemente arricchite, mentre milioni di italiani si sono indebitati anche a causa, come sappiamo,

Le assicuro che glielo diciamo senza nessun aiuto esterno, senza bisogno di nessun aiuto esterno, ma glielo diciamo - spero - non in solitudine, ma anche in quelle piazze che io sono convinto presto si riempiranno. Grazie, presidente cui la Presidente del Consiglio ha dato lettura questa mattina alla Camera dei deputati è stata molto articolata e ne ho apprezzato la volontà di esprimere non solo la posizione di Capo di Governo, ma anche quella della persona e principalmente della donna che ha l'onere e l'onore di ricoprire la più alta carica di Governo. Quel famoso tetto di cristallo, che lei stessa dichiarò di aver infranto quando si presentò alle Camere per chiedere la fiducia, è fatto di un materiale particolare, perché se viene infranto tende a ricostituirsi e ogni volta sembra essere sempre più duro. Questa metafora, signora Presidente del che sono consapevole - e penso di condividere con lei questa consapevolezza - che il ruolo delle donne in politica è fondamentale. Dopo questa premessa ci tengo a dirle che ho apprezzato il suo operato nelle missioni del 6 e dell'11 giugno con la presidente della Commissione europea Von Der Leyen e il *premier* olandese Rutte per giungere alla definizione di un pacchetto europeo a sostegno di Tunisi. Esprimo soddisfazione per l'inserimento di questo punto nell'agenda di politica estera del Consiglio europeo. posso confermare che il tema della stabilità dei Paesi del Nord Africa è fondamentale, non solo per la sicurezza del nostro continente con riferimento alle politiche migratorie, ma anche per la tutela dei pescatori siciliani, spesso oggetto di assalti e financo di provvedimenti di sequestro delle navi ad opera delle autorità dei Paesi costieri africani. In questi casi più volte si è reso necessario l'intervento dello Stato italiano per la liberazione degli equipaggi che vengono trattati come predoni del mare, quando la loro unica colpa è quella di essere andati a pescare nelle acque territoriali italiane e comunque nel limite della fascia di mare internazionale. In questo, signora presidente del Consiglio Meloni, approvo ogni intervento volto a favorire una politica comunitaria a tutela dei diritti degli italiani che lavorano sul mare e che sul mare trovano le risorse per l'economia siciliana

pongono gravissimi problemi per la stessa isola e la spingono al limite della sostenibilità. Sia chiaro che non è in discussione il dovere di accogliere e prestare soccorso ai migranti; ciò che l'Italia deve rivendicare è proprio, come dice lei, l'importanza del suo ruolo e della sua posizione geografica, che da estremo confine meridionale dell'Europa deve trovare proprio in questa condizione le ragioni per ribadire la centralità del suo ruolo e la sua autorevolezza per difendere le sue legittime posizioni. In tal senso, l'inclusione permanente dell'Unione africana nel G20, a favore della quale si è espresso questo Governo, costituisce una scelta che merita condivisione, perché consentirà l'ingresso di una nuova e autorevole voce, cioè quella dei Paesi africani, nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide globali. Questo Consiglio europeo è chiamato ad esprimersi ancora una volta sulla guerra in Ucraina. È molto complicato esprimersi e addentrarsi in un'analisi di quanto accaduto lo scorso fine settimana, anche perché troppi elementi sono ancora sul piano delle ipotesi; tuttavia, più le unità della Wagner si avvicinavano a Mosca (come seguivano in una diretta quasi convulsa con i telegiornali che davano gli aggiornamenti), più ci è apparsa giusta la posizione assunta dall'Italia dall'inizio del conflitto. Come abbiamo già detto ieri in quest'Aula nella discussione sulle missioni internazionali, in un quadro internazionale così fitto di incognite, turbolenze e potenziali minacce per la pace e la stabilità, è essenziale che l'Italia resti saldamente ancorata alla sua dimensione europea e ai patti dell'Alleanza atlantica. Su questo, signora presidente del Consiglio Meloni, le sue parole e i suoi atti non hanno mai lasciato spazio a dubbi. Abbandonare l'Ucraina al proprio destino avrebbe significato rinnegare i principi fondamentali del diritto internazionale che sanciscono la sovranità territoriale di ogni Stato. Questo impegno, però, non deve mai perdere la tensione e la speranza per giungere quanto prima alla fine delle ostilità. Proprio oggi il presidente della CEI, cardinal Zuppi, è a Mosca. È un tentativo, quello della Santa Sede, che va guardato con rispetto e attenzione, e ci auguriamo che da questa iniziativa possano nascere dei corridoi umanitari, per mettere fine a uno dei crimini più odiosi di questa guerra, quello dei bambini strappati alle loro famiglie e deportati in Russia. Anch'io, come madre, come lei, provo un vero e proprio orrore per questo che è a tutti gli effetti un crimine di guerra, e pertanto la esorto sinceramente, signora Presidente, ad adoperarsi con ogni mezzo per il ripristino di quelle garanzie minime di soccorso e di solidarietà internazionali che in questo conflitto sembrano sembrano essere state spazzate via da una strategia bellica che ha colpito con crudeltà i civili e, fra essi, i più indifesi: le donne, i bambini e gli anziani. Sulla politica economica, signora Presidente, ben venga l'intervento per la fine dell'austerità e l'approccio che lei ha definito "a pacchetto" sui temi delle regole del Patto di stabilità, del completamento dell'unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria. Condividiamo con lei la preoccupazione che l'aumento dei tassi, intrapreso dalla Banca centrale europea, si riveli una soluzione semplicistica, che non è in grado di risolvere le ragioni della crisi inflazionistica, con il conseguente aumento dei prezzi. pur ritenendo che la ricetta della BCE non sia adeguata alla cura, non possiamo dimenticare che sul fronte interno ci sono questioni non risolte, che bloccano l'economia, come la questione del superbonus e del *bonus* 110 per cento, per le quali aspettiamo ancora dal Governo che ci dica come le vuole risolvere, restituendo la liquidità alle imprese che in questi strumenti hanno creduto e che adesso si trovano con opere incomplete e senza le risorse economiche per andare avanti, mentre le banche si trovano a gestire crediti cartolari, dei quali non se ne fanno nulla. Concentriamoci anche sul PNRR: avviare un confronto con l'Europa per una rinegoziazione o, in generale, per semplificare le informazioni e le procedure per i finanziamenti europei, concedendo flessibilità nello studio dei fondi europei, per favorire e finanziare gli investimenti in settori strategici, cioè il famoso *step* che lei ha citato oggi, non è certamente un'eresia. Il punto, tuttavia, è cosa si chiede. Ben venga tutto quello che possa rafforzare la transizione ecologica, la competitività del sistema produttivo e il contrasto alle diseguaglianze territoriali, ma non dimentico che la settimana scorsa la maggioranza alla Camera dei deputati ha bocciato un ordine del giorno che chiedeva al Governo di rispettare gli impegni presi sugli asili nido. E questo è un pessimo segnale, unito al fatto che ancora non è chiaro come il Governo vuole vuole riscrivere il PNRR. Se non è chiaro al Parlamento, fatico a capire su quali basi si possa avviare questa discussione in Europa. Per concludere, signor Presidente del Consiglio, pensiamo che l'autorevolezza e il rispetto,

al percorso europeo della Moldova), sia quando si tratta di tradurre in atti politici le proprie esigenze su questioni nazionali, come quelle sui migranti, sulle politiche umanitarie e sul PNRR. Il comportamento, cioè, di un Paese che sia fieramente e convintamente europeista e che nell'Europa e dall'Europa troverà gli strumenti per affermare la propria autorevolezza, nello scenario internazionale, garantendo la stabilità e la crescita economica.

l'intervento della Presidente del Consiglio è, come sempre in questi casi, sospeso tra due registri. Da un lato c'è il tono più istituzionale, tipico di chi si accinge per la quarta volta a un impegno anche molto importante, persino un po' burocratico, come quello del Consiglio europeo, e dall'altro c'è quello tipico della nostra Presidente, che ama molto, in particolar modo in sede di replica, rispondere punto per punto, anche con toni che talvolta scendono un po' più nel campo dello scontro politico, in alcuni casi anche della propaganda e direi del dibattito da *talk show*. Credo che siano questi i momenti in cui la Presidente si diverte di più e anche noi talvolta ci divertiamo. Sarebbe bello replicare punto per punto, ma sono certo che non mancheranno occasioni in cui potremo, nelle sedi dei *talk show*, dialogare, discutere e rinfacciarle tutte le considerazioni, signora Presidente, che anche lei giustamente rinfaccia a noi. Ciò anche perché chi governa ha sempre un problema di rapporto complicato con la coerenza: lo abbiamo avuto tutti. Ce l'ha in particolar modo la Presidente del Consiglio, perché ha fatto della coerenza la sua carta vincente alle elezioni. Ed è normale che in alcuni momenti, essendo il Governo l'arte del compromesso, essendo il Governo il luogo in cui si compongono opinioni diverse, questa coerenza venga meno. Presidente, lei ieri ha fatto due ottime scelte (lei e i suoi colleghi del Consiglio dei ministri). e avviato l'*iter* per la nomina del Governatore della Banca d'Italia nella persona di Fabio Panetta. *(Applausi)*. Bravi, farà sicuramente meglio di Visco (anche perché peggio è difficile), ma soprattutto è una nomina che va nella direzione giusta, quella di ridare autorevolezza alla Banca d'Italia. Lei però non può venire stamattina in Aula e dire che la Banca centrale europea ha sbagliato tutto, perché Fabio Panetta in questi anni era a Francoforte,

mi piacerebbe, punto punto, mettermi a discutere con la Presidente del Consiglio, anche con un po' di sana autoironia. Per esempio oggi la Presidente ha detto una cosa giustissima (me la sono segnata): ha detto che la fermezza è la prima forma di prudenza (si riferiva alla politica estera). Io sono d'accordo con il Governo su questo. Non altrettanto lo era l'attuale Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione e quando c'era un altro Presidente del Consiglio, del quale eviterò di citare il nome (era il 2016), che ella definiva un "idiota" (ma era una citazione affettuosa, dostoevskijana direi), perché schierava le truppe della NATO in Lituania. Io quell'ex Presidente del Consiglio lo conosco e le garantisco che non se l'è presa a male; però, insomma, come si cambia vale per tutti. Allora, se dobbiamo fare di questo luogo un luogo di dibattito da *talk show*,

Ma, in ogni caso, questo dibattito tra di noi per me lascia il tempo che trova. Potrei impiegare i miei dieci minuti a replicare punto punto; alla fine torniamo a casa e ci mandiamo un messaggino su chi ha fatto la battuta più bellina, però siamo punto e a capo. Perché? Perché la mia opinione, della quale, signor Presidente, per suo tramite vorrei mettere a conoscenza il Parlamento, è che la situazione dell'Europa sia drammatica. Io vengo da una cultura diversa da quella di tanti di voi, amici e colleghi della destra, perché sono un convinto europeista, che non è mai stato un sostenitore dell'Europa delle Nazioni. Invito tutto il Parlamento a leggere uno straordinario intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Mantovano, che in una sede per me importante, quella di una rivista che fa la differenza e che si chiama "Tempi", ha fatto una riflessione culturale interessantissima, arrivando a delle conclusioni diverse dalle mie, ad esempio su Ventotene. Invito chi ha tempo a leggere questo intervento di Mantovano. Perché dico questo? Perché chi parte da questa lettura, che non è la mia, e chi invece parte dalla lettura di Ventotene e degli Stati Uniti d'Europa (il sogno nel quale noi portammo Merkel e Hollande a dialogare, perché l'Europa per noi ripartiva da lì), entrambi dobbiamo prendere atto che la situazione politica dell'Europa è drammatica. Se non partiamo da questo giudizio, che è profondamente diverso da quello dell'Europa di dieci anni fa, restiamo attaccati ai nostri stereotipi e ai nostri pregiudizi ideologici, dividendoci in sovranisti e non sovranisti, senza avere uno sguardo su quello che sta accadendo. Mi spiego e vado rapidamente a chiudere. L'Europa ha una crisi demografica senza precedenti. È dai tempi della crisi dell'Impero romano che una civiltà non ha una crisi demografica così significativa Noi siamo mezzo miliardo di persone (anche meno, da quando se n'è andato il Regno Unito); gli altri sono sette miliardi e mezzo. E gli altri cambiano. Rispetto a quando io stavo in quei banchi lì, c'è una Cina che è diversa da prima. Vi abbiamo richiamato a una riflessione e io sono d'accordo con la Presidente del Consiglio, quando dice che noi siamo dentro *One Belt One Road*, ma altri fanno più affari di noi. Dieci giorni fa il nuovo Primo Ministro cinese se n'è andato a Berlino e ha fatto degli accordi, mi pare per una ventina di miliardi, con i tedeschi. Allora, anche su questo o L'Europa è unita o non lo è. È un tema interessante da affrontare. Fatto sta che c'è una Cina prima Xi Jinping e dopo Xi Jinping; c'è un'India (un miliardo e mezzo di persone, più dei cinesi) prima Modi e dopo Modi; c'è un Brasile che è cambiato rispetto al Brasile di due anni fa, perché la visione terzopolista di Lula, che porta Dilma Rousseff a fare la presidente della banca indicata dai cinesi, la banca dei Paesi dei BRICS, è un elemento di novità che non va sottovalutato. Il Medio Oriente vede nella *leadership* saudita più giovane rispetto a quelle precedenti un cambio radicale, non solo per il Medio Oriente, ma anche per i Paesi africani, dove i Paesi più popolosi, a cominciare da Nigeria, Etiopia ed Egitto, vivono le difficoltà che sappiamo. In questo quadro, come se non bastasse, gli Stati Uniti hanno una debolezza strutturale, che è la debolezza della loro democrazia, e vi sono stati due unici elementi di novità dall'Europa in questi in questi ultimi dieci anni. Il primo è la Brexit: non propriamente un fatto positivo per l'Europa, ma nemmeno per il Regno Unito, se è vero - com'è vero - che qualcosa sta cambiando. Lo dico perché anche in questo Parlamento in tanti applaudirono la vittoria di Farage nel 2016; qualcuno era persino compagno di banco di Farage al Parlamento Europeo. Dall'altro lato la vicenda ucraina. Noi condividiamo la linea del Governo, ma diciamo anche che siamo in una situazione in cui, dopo ciò che è successo in Ucraina, nulla sarà più come prima per il nuovo disordine globale e per l'Europa, perché quando l'Ucraina entrerà dentro l'Unione europea - ed è bene che ci entri doppio della Germania; il doppio no, ma è più grande della Germania. È un Paese che cambia radicalmente le regole del gioco in Europa e noi vogliamo che prima possibile vi sia la fine della guerra e l'Ucraina entri nell'Unione europea. Noi siamo dalla parte giusta, dalla parte degli ucraini, ma diciamo anche che questo porterà una serie di modifiche strutturali. Di fronte a queste modifiche strutturali, la mia impressione è che non ci sia sufficiente consapevolezza nelle *leadership* europee del fatto che stiamo rischiando di perdere il treno europeo. Non è un problema di dividerci tra di noi, di farci le battutine, di farci le polemiche sullo spazio, sulle biotecnologie, sulle *startup*, sulle infrastrutture, persino sulle università (oggi è uscita l'ennesima classifica) o sulla cultura e lo sport.

anche perché, se vuole mantenersi coerente con i principi con cui ha vinto le elezioni (di questo dobbiamo prendere atto, essendo un dato di fatto oggettivo), dobbiamo avere l'intelligenza politica di sfidarla su temi che siano un po' più elevati rispetto a quelli che talvolta mettiamo in campo. Questo vale anche per lei, perché quando lei arriverà al Consiglio europeo non rappresenterà più Fratelli d'Italia, ma rappresenterà fratelli, sorelle, nipoti, papà: rappresenterà tutta l'Italia. Se questo è vero, signor Presidente del Consiglio, noi sappiamo che lei avrà un grande compito nei prossimi anni, contro la nostra volontà, perché avremmo voluto che lei non vincesse le elezioni. Ma lei sia all'altezza di questo compito, ci rappresenti, sapendo che quello che si sta discutendo non è più un dibattito interno tra noi e voi, è l'idea di che tipo di Europa avremo domani, perché il rischio è che l'Europa diventi quel pessimo incubo burocratico che sostituisce il sogno politico e diventa, purtroppo (lo faccia dire a chi crede di essere un cittadino europeo, crede di essere convintamente dalla parte degli Stati Uniti d'Europa), Uniti d'Europa), la più grande occasione perduta anche dal nostro Paese. Buon lavoro, signora Presidente. Signor Presidente, la situazione internazionale e gli accadimenti intorno a noi rendono sempre più centrale una risposta europea sui grandi temi temi e l'Italia deve continuare a fare la sua parte, come sta già autorevolmente facendo da alcuni mesi. Ci sono due modi per presentarsi in Europa e sedersi al tavolo dei ventisette: adottando una posizione subalterna con un approccio di inferiorità che somiglia molto alla sindrome di Stoccolma; il secondo, quello che stiamo sperimentando dall'ottobre scorso, quando cioè per la prima volta dopo undici anni si è insediato un Governo politico votato dagli italiani, un Governo di centrodestra, è di porsi da pari a pari di fronte ai nostri partner europei. Uguale dignità, uguale rispetto, uguale credibilità, ma soprattutto uguale autorevolezza nel dare le carte, né più né meno degli altri Stati. È proprio come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, che capì forse per primo quanto avere solide relazioni internazionali e positive relazioni interpersonali fosse indispensabile per governare meglio un grande Paese come l'Italia. Presidente Meloni, lei ha parlato diffusamente di immigrazione. La sua linea e la linea di questo Governo sulle politiche migratorie, i contributi, le sollecitazioni all'Europa, sono andati a segno. Grazie all'azione convinta e testarda, nello stesso tempo anche seria e credibile, di questo Governo, oggi in Europa è cambiato il paradigma. Avevamo sottolineato a più riprese che i confini dell'Italia in realtà sono i confini dell'Europa e che dunque il tema dell'immigrazione andava affrontato in modo globale, in una logica europea e con la volontà da parte dell'Unione europea di intervenire in Africa, a partire proprio dalla Tunisia. di dire che soltanto un cieco, una persona in malafede potrebbe negare che questo cambio di approccio vi sia stato, fin dal Consiglio europeo del febbraio scorso, passando dalla missione a Tunisi, e per finire con l'impegno della Commissione a stanziare nel prossimo bilancio pluriennale ingenti risorse per la cosiddetta dimensione esterna delle politiche migratorie. Mettere in sicurezza la Tunisia ed evitare il suo collasso politico, economico e sociale è la vera urgenza: se la pentola a pressione dovesse saltare, ci ritroveremo migliaia di immigrati irregolari, pronti a salpare dai porti tunisini verso l'Italia e da lì provare a proseguire il loro viaggio della speranza verso l'Europa settentrionale. Ben venga dunque la sottoscrizione di un accordo Unione europea-Tunisia, che nasce proprio dalla lungimiranza e dall'insistenza del Governo italiano. La rotta è tracciata ed è giusta; la via tracciata in Europa è quella del Governo italiano e dobbiamo andarne fieri, con buona pace degli scafisti, dei mercanti di uomini che sono i veri responsabili - quelli sì -, i veri assassini dei disperati che muoiono in mare e la cui condotta deve essere stroncata, come abbiamo fatto, per esempio,

abbiamo tutti seguito con apprensione gli avvenimenti degli ultimi giorni con la marcia su Mosca dei mercenari della brigata Wagner, accompagnata da tanti aspetti che non conosciamo del tutto e che non è facile ovviamente decifrare. I fatti però, non la propaganda, dimostrano che il gigante è debole e vulnerabile, sperando che questa fase possa portare ad un deciso dialogo per avviare i negoziati di pace, che ovviamente tutti auspichiamo, ma che non possono essere penalizzanti per una Nazione aggredita come l'Ucraina, che deve tornare ad essere davvero libera, davvero indipendente. La pace giusta e duratura si ottiene con i negoziati, sì, ma è impossibile se una delle due parti è sorda o cieca. In questo quadro, bene fa dunque il Governo ad assicurare il massimo sostegno al popolo ucraino: un supporto politico, economico, umanitario militare che ovviamente permetta al Paese di difendersi. Dobbiamo lavorare a questo esito anche perché un mondo pacificato è un terreno più fertile per la crescita economica. Viviamo ancora tempi difficili, con un'inflazione che continua a mordere e rispetto alla quale sono fondamentali gli interventi del Governo per sostenere famiglie ed economia; che la signora Lagarde, dai palazzi di Francoforte, vorrebbe che noi interrompessimo, proprio mentre la BCE annuncia un imminente ulteriore rialzo dei tasti di interesse. Noi lo diciamo da europeisti convinti e anche nel rispetto dell'autonomia della BCE: questa linea è suicida e proseguire questa cura da cavallo, che rischia di tradursi in una mannaia, manderà sul lastrico decine di migliaia di famiglie e imprese, provocando un impoverimento collettivo. Presidente Meloni, so di non doverla convincere in merito. Le chiedo, però, di esercitare tutto quanto in suo potere per invertire la rotta, perché non possiamo costruire in Italia, per poi vedere i nostri sforzi annullati da una miope politica monetaria europea. Abbiamo ascoltato le sue repliche, alla Camera e anche qui in Senato. Il Governo sta subendo pesanti pressioni sulla ratifica del MES. Noi riteniamo che la questione non possa e non debba essere affrontata da sola. È necessario inquadrarla in una cornice più ampia, ovviamente, prima di ratificarla acriticamente. Deve includere, per esempio, la modifica del Patto di stabilità, affinché esso non sia un ritorno alla rigidità, quella che per anni ha ha badato alla stabilità, con pessimi risultati, e ben poco alla crescita. Durante il Covid-19, la sospensione del Patto di stabilità ha ridato fiato all'economia e spinta alle imprese. Dobbiamo insistere affinché vengano scorporate le spese per ambiente, transizione verde, digitale e difesa.

Qui sta tutta la differenza tra un'Europa che muore di austerità e un'Europa che rilancia su crescita e competitività. Noi di Forza Italia, che dal 1994 siamo in campo con questo spirito e con queste parole d'ordine, non abbiamo dubbi su quale Europa puntare. Presidente, tra i tanti temi di politica estera che affronterete c'è, finalmente, il grande tema del rapporto con la Cina: un rapporto difficile, controverso, che abbiamo lasciato correre forse troppo. Ci siamo ritrovati totalmente in condizioni di dipendenza per alcune materie prime e per alcune tecnologie. Parliamo di due approcci, quello europeo e quello cinese, in cui c'è assoluta necessità di *standard* e di regole comuni nell'interesse dell'Europa stessa, proprio per evitare che essa venga fagocitata dall'espansionismo senza regole di Pechino. Per quanto riguarda noi, lo dicevamo nel 2019 e lo ribadiamo oggi: sottoscrivere il *memorandum* sulla Via della seta è stato un errore strategico che ha visto l'Italia essere il primo e unico Paese dell'Europa occidentale a farlo. Continuiamo a ritenere che, alla scadenza dello stesso, l'Italia non abbia alcun interesse a rinnovarlo perché, come sosteneva il nostro presidente Berlusconi, che già ne intravedeva i pericoli, le opportunità si sono rivelate di gran lunga inferiori ai rischi. Quindi, affidiamo nelle mani del Governo il negoziato migliore possibile, che ci consenta, da un lato, di riaffermare i nostri valori in continuità con i nostri alleati occidentali e, dall'altro, di non penalizzare le nostre imprese. Infine, presidente Meloni, voglio cogliere l'occasione, anche se si tratta di temi che non sono proprio all'ordine del giorno del Consiglio europeo, per ribadire una posizione ferma e decisa di contrarietà a tutti quei *dossier*, intrisi di ideologia ultra ambientalista, che hanno trasformato una grande opportunità come la transizione verde in un incubo per famiglie, cittadini e imprese. Auto elettriche, case *green*, imballaggi, nutri-score e quant'altro: sono tutte normative pensate con arroganza dal commissario Timmermans e totalmente scollegate dalla realtà! ora stanno anche cercando di accelerare, perché hanno paura che quel centrodestra di Governo, che sta dando ottima prova di sé in Italia, possa prendere forma anche in Europa e mandare a casa le sinistre anche nelle istituzioni della democrazia europea.

credo di dover ringraziare il Presidente del Consiglio per il suo intervento. anche noi non vorremmo vedere un Presidente del Consiglio, per citare le sue parole, impaludata. E non l'abbiamo vista impaludata, oggi come in diverse altre occasioni. Noi vorremmo, però, che il Presidente del Consiglio e il Governo evitassero delle sgrammaticature istituzionali vergognose, come ad esempio quelle fatte oggi nell'intervento di replica dal Presidente del Consiglio che, da Presidente del Consiglio, in vista di un Consiglio europeo, attacca una forza di opposizione con parole inaccettabili. Credo, infatti, che quando il Presidente del Consiglio va in Europa rappresenti il mio Paese e rappresenti anche tutti quegli italiani che non la pensano come il Presidente del Consiglio, ma avrà il nostro supporto quando difenderà gli interessi dell'Italia in Europa. Ora invece assisto ad attacchi strumentali, con parole inaccettabili e risponderò puntualmente alle domande che il Presidente del Consiglio ha posto alla mia forza politica in quest'Aula. Ritengo però surreale dover rispondere delle dichiarazioni di un non iscritto al MoVimento 5 Stelle che liberamente, da sociologo e da cittadino, fa le dichiarazioni che ritiene. *(Applausi)*. Ritengo profondamente sbagliata la posizione di chi dice che è meglio vivere in una dittatura che sotto le bombe in una guerra, perché la libertà è un principio che va difeso in modo totale. Rispondo anche sulla questione di che cosa comporta la sospensione dell'invio delle armi. Noi la riteniamo come l'unico elemento, oggi, di potenziale discontinuità in un processo che da oltre un anno e quattro mesi non sta portando ad alcun progresso sul fronte della pace.

che sta davvero cercando di affrontare il tema della guerra e della pace nel modo corretto e coerente. Oggi c'è una missione di pace fondamentale e noi vorremmo che il nostro Governo si schierasse a fianco del Santo Padre da questo punto di vista. Sul ruolo della Chiesa non serve scomodare certamente un precedente storico importante come quello del 1962, con Giovanni XXIII, con il ruolo che ebbe la Chiesa in quel momento, ma credo che quelle parole vadano riviste oggi, nella situazione attuale, perché sono assolutamente contemporanee.

oppure viene sconfessato dal Governo, dalla sua forza politica, dalla Presidente del Consiglio? Faccio anche un'altra domanda, perché ho sentito, in risposta all'intervento del collega Lorefice, dire che rinunciare alla propria capacità di difesa in ordine alle spese militari europee non è mai gratis, perché c'è sempre qualcun altro che deve difenderti. Allora chiedo qual è il prezzo della difesa che stiamo facendo in Ucraina in questo momento? Perché se non è gratis la difesa, ad esempio, degli Stati Uniti verso l'Europa, non è gratis neanche la difesa che l'Occidente sta facendo in questo momento in Ucraina. A che cosa porterà quella follia che, secondo me, è l'ambizione del pareggiare le forze militari in campo? Significa dotare l'Ucraina delle armi nucleari? E questo a cosa porta? Se la domanda che mi è stata posta è a che cosa porta rinunciare all'armamento, io chiedo a che cosa porta continuare ad armare? Quello che mi dispiace è la banalizzazione che si è fatta, nell'intervento del Presidente del Consiglio, di problemi molto complessi, che citava in parte il senatore Renzi. Renzi. Ciò che stiamo vivendo in Europa in questo momento, frutto anche di un diverso atteggiamento cinese degli degli ultimi anni, con l'espansionismo economico e quindi con la Cina rivolta al mercato esterno, con una stagione come quella di Trump che ha portato invece gli Stati Uniti a guardare al proprio mercato, America First, quindi al protezionismo americano interno che ha cambiato completamente il paradigma, ha in qualche modo messo al centro l'esigenza di avere un'Europa più forte anche all'interno dell'Alleanza atlantica, dove dobbiamo avere il coraggio di dire quello che pensiamo veramente. La Presidente del Consiglio non è stata chiamata dal Presidente degli Stati Uniti e io non ne godo, non ne sono contento, anzi avrei preferito vedere riconosciuta la centralità del mio Paese nell'ambito europeo, ma non è colpa nostra se questo non è accaduto. Mi auguro che l'autorevolezza del nostro Governo porti nuovamente gli americani a considerarci veramente autorevoli sui temi europei. Ma veniamo ad altri elementi. Ho dimenticato un passaggio che, però, non voglio tralasciare: aver citato Borsellino, quella sì, è davvero una vergogna inaccettabile Dopo che il Presidente del Consiglio è andata in quelle terre a parlare di pizzo di Stato in riferimento alle tasse del nostro Paese, ci viene a chiedere conto della questione della lotta alla mafia? A noi? la banalizzazione viene proposta anche sul tema della Via della seta, che il Governo Conte I, assieme alla Lega, ha sottoscritto all'interno di un *memorandum*. La banalizzazione è questa: il principio che chi ritiene che non ritiene che non sia impossibile a prescindere parlare di rapporti commerciali con un Paese in espansione come la Cina diventa filo cinese. Ho portato in Consiglio dei ministri un *golden power* per bloccare l'operazione di acquisizione da parte di Syngenta di Verisem, primo *golden power* totale di blocco di un'operazione di una società cinese che voleva acquisire una società sementiera italiana perché ritenni che quella fosse un'operazione strategica ma le cose nel mondo accadono e o le guidiamo o le subiamo. Nel porto di Trieste c'è una concessionaria che ha ceduto il 50,01 per cento del proprio capitale al porto di Amburgo, che oggi a sua volta ha ceduto il 25 per cento a Cosco, che è una società cinese. Le cose accadono e bisogna guidarle, altrimenti le subiremo.

mi piacerebbe avere un Governo che credibilmente ponga le questioni di un ritorno spaventoso all'austerità e alle regole europee che hanno fatto del male al nostro Paese, ai parametri di Maastricht, al 3 per cento, al rapporto debito-PIL,

Abbiamo bisogno di avere un *carnet* di strumenti contro l'austerità e le possibilità di investimento in cui qualsiasi Stato membro può scegliere gli attrezzi migliori per la propria economia. Ma qual è l'autorevolezza di un Governo che chiede non austerità in Europa e la applica in Italia tagliando lo stato sociale *(Applausi)*, facendo soldi sui più poveri e occupandosi esclusivamente di chi ha già di più? il PNRR continuo a vedere uno scaricabarile sul Governo precedente. La chiudo banalmente: tre forze politiche della maggioranza attuale erano parte di quel Governo che ha scritto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e oggi volete prendere le distanze da ciò che avete contribuito a scrivere! Presidente, ho cercato di rispondere anche alle sollecitazioni del Presidente del Consiglio; non riesco ad affrontare tanti altri temi che avrei voluto citare. Sull'immigrazione, Presidente, attendiamo il blocco navale. Concludo, Presidente. Avevo un qualche imbarazzo sulle modalità di conclusione di questo intervento, ma me l'ha tolto, per suo tramite - la ringrazio - il senatore Scurria, che ha chiesto se abbiamo mai visto un Governo così. Grazie a Dio no! E speriamo di non vederne

egregi membri del Governo, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, presidente Meloni, nell'annunciare il nostro voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, in questa dichiarazione di voto intendiamo soffermarci su tre punti principali contenuti tra i temi che verranno trattati nel Consiglio europeo di domani e dopodomani: il tema dell'immigrazione, il tema economico e, naturalmente, la questione legata alla guerra Ucraina-Russia. Sul tema dell'immigrazione, signora Presidente del Consiglio, il Governo italiano si sta muovendo molto bene con le recenti missioni fatte proprio a Tunisi, per cercare di garantire la stabilità politica ed economica di questo Paese. È un nuovo modo di muoversi per cercare di contrastare l'immigrazione, cercando anche di dare stabilità al Nord Africa, anche perché se non si aiuta e non si dialoga col Governo tunisino, se quel Governo dovesse cadere, come qualcuno ha auspicato, quale sarebbe l'alternativa? Ricordiamoci l'instabilità che è seguita ad altre cadute di governo nel Nord Africa e soprattutto alle conseguenze che poi ha portato. Bisogna insistere con l'Unione europea, come sta facendo il Governo italiano, e anche col Fondo monetario internazionale proprio per finanziare la Tunisia, anche perché se l'Occidente non dovesse aiutare e sostenere la Tunisia, abbiamo visto che già la Cina si sta proponendo come alternativa e naturalmente questo significherebbe che se non aiutiamo noi Tunisi, rischiamo di lasciare un Paese centrale nella politica del Mediterraneo in mano alla Cina e naturalmente, di conseguenza, anche alla Russia.

prevalenti nell'Unione europea, figlie di un certo capitalismo senza regole, che spinge per un'immigrazione incontrollata solo per far proliferare manodopera a basso costo (altro che salario minimo), devono lasciare spazio al fatto che la sicurezza dei confini è una questione di sicurezza nazionale. *(Applausi)*. Questo è ciò che dobbiamo ribadire. Il nostro ministro Salvini ha dimostrato nei fatti, quando era Ministro dell'interno, essere pronto a battersi per difendere i confini nazionali e, anziché processarlo per questo, bisognerebbe proprio far capire che la sicurezza dei confini è una questione di sicurezza nazionale.

ci stiamo accorgendo che anche l'Unione europea stenta un po' a intervenire, quindi l'aiuto della NATO da questo punto di vista può essere molto importante. È quindi bene che il Governo prosegua su questa strada. Sui temi economici,

nell'Unione europea non sono le stesse che ci sono state negli Stati Uniti. Infatti, l'aumento della domanda è stato reale negli Stati Uniti d'America e per questo motivo il rialzo dei tassi della Federal Reserve di fatto ha funzionato, anche se non con la rapidità attesa. In Europa non era la domanda a crescere, ma l'offerta a restringersi per ragioni geopolitiche che hanno fatto diventare l'energia Il rincaro di gas ed elettricità a catena hanno fatto aumentare i costi di produzione anche di altri settori, in testa quello alimentare. Vanno trovate altre strade, perché andando avanti di questo passo, oltre a deprimere l'economia, rischiamo di far pagare un prezzo troppo alto

A tal proposito rendiamo noto che proprio la Lega oggi ha presentato una mozione per chiedere al Governo di introdurre, laddove sia fattibile (noi crediamo di sì), dei meccanismi che consentano di sospendere se non proprio il pagamento delle rate, almeno il differenziale determinato dai rialzi del tasso di interesse,

citando il tema della guerra tra Ucraina e Russia. Nei giorni scorsi abbiamo registrato che il mondo ha trattenuto il respiro, sia per il timore che le rivolte interne alla Russia possano far cadere nelle mani sbagliate le testate nucleari, sia per il rischio che Putin stesso, messo in un angolo, diventi ancora più pericoloso. Si registrano una Bielorussia sempre più dentro le dinamiche putiniane, dispiegamento delle atomiche russe sotto il controllo di Mosca sul territorio bielorusso ed è al via anche la costruzione di un campo militare capace di ospitare 8.000 mercenari della compagnia La Polonia ha già rafforzato i controlli al confine con la Bielorussia. La Germania dispiegherà in Lituania, da quello che abbiamo letto, in modo permanente, una robusta brigata di 4.000 soldati. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di recente ha dichiarato, a proposito del nucleare russo, che la minaccia di usare le bombe tattiche è reale. Giorno dopo giorno sembra ci si avvicini ci si avvicini di più a un coinvolgimento diretto nella guerra, che ha come teatro proprio il territorio europeo. Alcuni analisti poi - che sia vero o meno - si sono addirittura spinti a prefigurare che potrebbe non essere escluso un futuro impiego diretto di soldati della NATO. Il rischio, dunque, è una guerra totale, oppure un Afghanistan europeo, come ha sostenuto di recente anche il governatore Luca Zaia. e dopodomani, i Paesi dell'Unione europea dovrebbero riflettere attentamente su ciò che sta accadendo, il che non significa cambiare posizione sull'Ucraina, che deve essere sostenuta. Lei, signora Presidente del Consiglio - questo magari la sorprenderà, perché lo dico io - sicuramente ha fatto la politica giusta, quella che bisognava fare e che avrebbe dovuto fare qualsiasi Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. Molto probabilmente l'avrebbe fatta anche il presidente Conte, se avesse vinto le elezioni. A maggior ragione, adesso ancora di più va sostenuta, alla luce anche della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si è tenuta nei giorni scorsi a Londra... automaticamente) ...*che ha visto la partecipazione di 60 Paesi, proprio per un anticipo sugli aiuti necessari a disegnare il futuro post-bellico di Kiev. Come però ha dichiarato proprio il ministro Crosetto, oggi ancora più di ieri serve il massimo sforzo da parte di tutti per una soluzione diplomatica, promuovendo ad esempio a livello europeo ogni iniziativa utile in grado di supportare e sostenere la missione diplomatica della Santa Sede, tenuto conto del ruolo universalmente riconosciuto al Capo di Stato vaticano. Ciò cercando di superare anche - e sto veramente chiudendo - quel convincimento secondo cui auspicare un cessate il fuoco e una tregua significhi essere putiniani, perché così fotografiamo la situazione reale, avvantaggiando la Russia, e questo significherebbe quasi legittimare l'invasione. No, non intendiamo questo. Quando parliamo di cessate il fuoco e di tregua, ciò significa lavorare per fermare questa guerra, a determinate condizioni, che possono anche prevedere il fatto che la Russia possa - anzi debba - sostanzialmente arretrare rispetto a quello che ha fatto, che però si possono trovare anche aprendo dei canali diplomatici, esclusivamente in un'ottica di ripristino della legalità internazionale. *(Applausi)*. Per dirla con una frase che si legge su una importantissima rivista di politica internazionale, in America naturalmente: è il momento di sviluppare una visione di come finirà questa guerra.

avrà pensato a delle distanze siderali sull'Europa, tra la maggioranza e l'opposizione, che probabilmente ci sono, perché anche dalle dichiarazioni di voto finali dei diversi Gruppi si percepiscono alcune distanze. Questo poi sarà però smentito dei fatti, perché il via libera dato dal ministro Fitto, già a Montecitorio, su alcune proposte fatte dai Gruppi di opposizione dà il senso della distanza che c'è, signora Presidente, tra i contenuti della risoluzione europea e la propaganda politica. *(Applausi)*. Propaganda, signora Presidente, che le confesso, a nome del Partito Democratico, non mi sarei aspettato con un tasso così alto proprio su temi così delicati. Ma voglio entrare nel merito delle questioni che lei ha sollevato e ricordare a noi tutti, ai colleghi, che abbiamo discusso e che ci esprimeremo, con questo voto, su questioni importanti inerenti al conflitto russo-ucraino, sulla politica industriale, sulla competitività del nostro Paese, sull'economia, sulla sicurezza e sulla difesa, sulla migrazione, sulle relazioni esterne e su altri punti. Cioè sulla carta d'identità della Repubblica italiana in Europa; e quella carta d'identità non cambia con la propaganda. Lo dico, signora Presidente, perché il Consiglio europeo discuterà anche delle relazioni con la Cina, dopo che il 20 giugno la Commissione europea ha presentato una comunicazione, che lei conosce bene, dedicata alla sicurezza economica, che fa seguito a quanto è emerso al vertice G7 di Hiroshima del maggio scorso e al discorso tenuto il 31 marzo dalla presidente von der Leyen. Sull'Ucraina il Consiglio europeo farà nuovamente il punto sulla guerra. La posizione del Partito Democratico è molto chiara, cristallina, limpida e non si presta a nessuna interpretazione particolare. Il numero di rifugiati ucraini in Europa ammonta a 6 milioni e in Italia ne abbiamo solo 183.000; potevamo fare molto di più, possiamo fare molto di più. Lo dico perché c'è un pezzo di Europa che si è messa sulle spalle, molto più di noi, il dramma dei rifugiati ucraini e lo dico perché ucraini e lo dico perché su questo tema, quando noi vi chiediamo, dopo aver sostenuto l'azione del Governo e l'azione dei Governi europei, di adoperarvi in sede europea e internazionale per un negoziato, a cui ha fatto riferimento il collega Delrio prima, che consenta una soluzione diplomatica europea, volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, tutto questo non è alternativo al sostegno all'Ucraina e non è alternativo alla linea coerente che l'Europa sta avendo al fianco del popolo ucraino. *(Applausi)*. Non è alternativo, è complementare e rafforza la credibilità dell'Europa, dentro la quale l'Italia non è solo braccia, ma è braccia e cuore. Signora Presidente, braccia e cuore; deve spiegarlo ai Gruppi parlamentari cui fanno riferimento i tre partiti oggi maggioranza in Italia, perché alcuni di questi Gruppi non considerano l'Italia, in questa Europa, né cuore, né braccia. Vale per gli ultra-nazionalisti a cui fa riferimento il Gruppo Lega in Europa e vale per i conservatori e riformisti (è un ossimoro, lei lo sa) che sono i nazionalisti a cui appartiene il Gruppo Fratelli d'Italia; così come Forza Italia fa lo sforzo, dentro i popolari europei, di tenere tutti insieme. Perché ribadisco questo concetto? Lo ribadisco perché proprio la differente posizione in Europa dei tre Gruppi che in Italia sono maggioranza sta trascinando il nostro Paese sul terreno dell'incoerenza sull'economia e sui migranti. Veniamo all'economia. Sono molto preoccupata - ci dice lei, presidente Meloni - del fatto che il Patto di stabilità potrà tornare alla fine del 2023 e sul PNRR non ho condiviso il metodo, non ne condivido la indebita i nostri figli ed è stato approvato senza dare al Parlamento la possibilità di approfondirlo. Signora Presidente, queste sono le sue parole, qualche mese prima che diventasse Presidente del Consiglio. Le do una notizia: il Patto di stabilità rischia di tornare, rischia di tornare, se lei non fa alcune scelte chiare, che dovrà fare con il suo Gruppo anche in Europa. Non solo se non le fa come Governo italiano, ma se non portiamo alcuni Paesi ad affrontare temi centrali che la Commissione ha posto sul tavolo, signora Presidente del Consiglio. Io non penso che sia molto patriottico criticare la Commissione e non assomiglia all'interesse nazionale criticare, oltre alla Commissione, un commissario italiano, per di più con una responsabilità importante agli affari economici. *(Applausi)*. Io non penso che sia molto patriottico, signora Presidente; penso che sia un errore, penso che sia il tentativo di trascinare, facendo propaganda, le contraddizioni che sono dentro quei tre Gruppi parlamentari in Europa, nella dinamica tutta italiana. Ma questo gioco prima o poi finisce. In ogni caso, mentre il gioco si allunga in Europa, il danno è solo italiano, è solo italiano, mentre noi avremmo bisogno di certezze. Nel nostro Paese vi è uno straordinario impegno delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e dei nostri territori.

Presidente del Consiglio, noi abbiamo un terzo delle Province italiane che hanno più pensionati che popolazione attiva. Quei territori coincidono - le do una notizia - con il Mezzogiorno, con le aree interne e con le aree di montagna, anche quelle ricche del Nord.

e imprese. Oltre alla propaganda sulla natalità, rispetto alla quale noi abbiamo preferito i fatti (ricordo l'assegno unico e ricordo tutte le politiche di sostegno alla natalità) forse dovreste prendere atto che c'è un pezzo d'Italia che ci chiede coraggio e quel coraggio va fatto atterrare in Europa. Invece no, continuiamo con la propaganda. senatore Misiani nel suo passaggio - di *credit crunch*, una fase in cui le politiche industriali segnano il passo, il portafoglio ordini diminuisce, l'edilizia che ha tirato negli ultimi trimestri è in grande frenata, mentre ci sono queste condizioni, voi che fate? Come se foste dei passanti, signora Presidente, criticate la Banca centrale europea e ci sta, perché fa una politica monetaria probabilmente non condivisibile. Ma voi non siete degli opinionisti, non siete non siete colleghi del povero De Masi che oggi avete fatto diventare oggetto del nostro dibattito pubblico. Signora Presidente del Consiglio, lei deve assumersi la responsabilità di dirci quali sono le politiche anti-inflazionistiche e le politiche industriali che mettete in campo per far sì che gli errori eventuali della BCE possano essere superati. Non basta criticare la BCE.

non lo molliamo l'osso fino a quando non sapremo cosa dicono le schede progetti. Evitiamo di fare propaganda su alcuni investimenti.

il Partito Democratico, non siamo ricattabili. Tiratele fuori le carte sui progetti che non vi piacciono. *(Applausi)*. Ditelo con chiarezza, non continuate a dirci che ci sono progetti che forse avevano delle caratteristiche. Tirateli fuori, non siamo condizionabili, vogliamo conoscere le schede progetto progetto per progetto e poi giudicheremo, giudicheranno i territori se è giusto o sbagliato. Rispetto a questo non ci preoccupa, ministro Fitto, la terza rata. Ci preoccupa la quarta rata, la quinta e la sesta rata, ma ci rivedremo e sono convinto che la sua disponibilità sarà sempre molto grande. rivolgendomi alla presidente Meloni, che finora è stata molto brava a nascondere le contraddizioni politiche all'interno della sua maggioranza. In Europa, i tre partiti fanno parte di famiglie politiche contrapposte e, a causa di queste divisioni interne, l'Italia appare ai margini del dibattito che oggi è in atto sulla *governance*, sul MES, sulla riforma del Patto di stabilità e anche sugli interventi del PNRR. Ma voglio dirle una cosa, cosa, signora Presidente del Consiglio: i nodi arrivano sempre al pettine e a quel punto il re è nudo; in questo caso il Governo è nudo di fronte alle responsabilità politiche e alle responsabilità della storia, e verrà fuori tutta l'incoerenza di questa maggioranza, qui e BOCCIA). Il PD è sarà sempre dalla parte del rafforzamento delle istituzioni europee. Se dopo gli insulti e la propaganda, anche in parte sentita in questo dibattito, il suo Governo sosterrà un rafforzamento dell'Europa, noi ci

puntualizzando che siamo contrari sul punto connesso alla Tunisia, limitandosi a rimettere questo tema sul tavolo del presidente La Russa, che è l'unico che può consentirci in questo caso di votare per parti separate la proposta di risoluzione

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, voglio ringraziare, non tanto da esponente di Fratelli d'Italia, né tantomeno da senatore della Repubblica italiana, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governo che guida per quello che sta facendo in questi mesi; lo sta facendo con un lavoro incessante, con grandissima determinazione e sta dando all'Italia una credibilità che non conosceva. Lo fa per dare più forza alle posizioni italiane in consessi sovranazionali, che spesso e volentieri vedevano nell'Italia semplicemente un Paese che seguiva le indicazioni e i *Diktat* che arrivavano

Oggi l'Italia è protagonista e porta un proprio contributo all'Europa che è fatto di proposte, di idee, di sensibilità e anche di umanità; quell'umanità di cui, secondo la descrizione di chi siede sui banchi di quella che oggi è l'opposizione, ma che per tanti anni è stata la maggioranza in questo Parlamento,

per l'appunto gli ideali dell'umanità eravate voi, ossia quelli che hanno governato nell'ultimo decennio senza aver preso alcun tipo di provvedimento efficace per contrastare ad esempio

sfumata accusa all'operato dei nostri militari e alle nostre forze dell'ordine, ma mai una parola di condanna nei confronti di coloro i quali lucrano sull'immigrazione. *(Applausi)*. chi ha guadagnato dall'immigrazione non sono solo gli scafisti. Forse anche perché, guardando al *cui prodest*, chi ha guadagnato da un'immigrazione clandestina senza regole in Italia negli ultimi decenni sono state non solo le organizzazioni criminali, che hanno potuto sfruttare la disperazione di chi arrivava dal Sud del mondo, ma qualche volta anche qualche cooperativa e qualche organizzazione legittima, qualcuno che ha costruito un'impresa e ha costruito guadagni sulla disperazione di chi arrivava dal Sud

Per garantire questo diritto, dobbiamo costruire rapporti e collaborazioni con l'Africa, che consentano

venga dunque, finalmente, la presa di coscienza da parte dell'Europa, grazie all'azione del Governo italiano, del fatto che non si difendono i confini esterni del continente, se non lo si fa tutti assieme, e che non si difende la sicurezza, la sicurezza, ma soprattutto la dignità, delle persone che, venendo in Europa, cercano di migliorare le loro condizioni di vita, dandole in pasto agli scafisti e condannandole, nella migliore delle ipotesi, ad essere sfruttate nel nostro mondo e, nella peggiore delle ipotesi, ad affondare drammaticamente nel Mediterraneo. Apprezziamo il sostegno che l'Unione europea finalmente ha deciso di dare e darà anche alla Guardia costiera libica, nel quadro del piano d'azione per il Mediterraneo centrale. da parte del MoVimento 5 Stelle e della sinistra, in particolare del Partito Democratico, evidentemente ci si dimentica di quali furono le posizioni quando c'erano altri Governi alla guida dell'Italia. E ci si dimentica, forse, che nella Commissione europea siede anche il commissario Gentiloni. Allo stesso modo, guardiamo con grande favore a un accordo di partenariato con la Tunisia, per rafforzare la cooperazione e gli scambi commerciali tra l'Europa e Tunisi. La Tunisia, nei primi mesi del 2023, ha superato la Libia in termini di flussi migratori verso l'Italia e la difficile situazione economica e sociale, potenzialmente esplosiva, rischia di avere conseguenze catastrofiche per il nostro Paese e per l'Europa. il presidente Meloni ed il Governo italiano a chiedere a tutti i livelli che le organizzazioni sovranazionali aiutino la Tunisia e la rafforzino anche economicamente in un quadro di questo tipo, dato che è parte integrante del piano Mattei, quel progetto ambizioso e visionario che mira a ripensare il rapporto tra Europa e Africa favorendo lo sviluppo, la stabilità e la crescita economica dei Paesi africani e a trasformare l'Italia in un *hub* energetico di primo piano. Questa è l'idea che abbiamo. Senatore Delrio, nel suo intervento prima ha detto alcune cose inesatte. Riferendosi ad alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ha detto che lo speronamento non ci fu. fu. Dispiace ricordarle, invece, che lo speronamento c'è stato e che Carola Rackete è stata assolta per il riconoscimento di una esimente, come mi ha ricordato il collega, avvocato senatore Balboni, che esclude la punibilità, ma non il fatto. È stata assolta, ma non perché il fatto non sussiste! In ogni caso, è davvero vergognoso che alcuni colleghi di questa Istituzione si indignino per opinioni di un Ministro e non abbiano provato vergogna grande senso di offesa nel momento in cui una nave battente bandiera straniera speronava una motovedetta della Guardia di finanza! *(Applausi)*. Ecco perché siamo diversi: certo che lo siamo,

modo certamente lei ha detto che ci sono cose che noi non abbiamo detto. È vero, ci sono tante cose che voi non avete detto. Abbiamo ascoltato il vostro silenzio complice, dal punto di vista politico, quando con il *green deal* avete permesso che venissero colpite le imprese europee a vantaggio degli interessi del Paese di un altro Continente, come la Cina oppure quello che non avete detto e non avete fatto per difendere gli interessi delle catene produttive italiane ed europee; sul vostro fallimento, poi, sulla globalizzazione e sulla liberalizzazione dei mercati, c'è stato un silenzio assordante, ma voi parlate con una narrazione una narrazione della quale ormai siete diventati vittime, fantasiosa sulla quale avete cercato e continuate a cercare un consenso che drammaticamente non vi arriva, nonostante cerchiate di ampliare i vostri campi d'azione. Ecco perché oggi, con questo Governo, ci poniamo in modo diverso in Europa. Va bene, presidente Meloni, il programma STEP, che certamente è un primo passo per la costituzione di un fondo sovrano europeo, ma è giusto adoperarsi con

altrimenti invece di permettere alle nostre imprese e alle nostre aziende di svilupparsi e di crescere vivremo un periodo di stagnazione. Visto che Visto che ormai abbiamo esaurito il tempo e non voglio prendere troppi rimproveri da parte del Presidente,

Ci aspettavamo nel merito un'opposizione battagliera, piena di contenuti da proporre e invece, come dicevo prima, siete vittime di una narrazione che continua a vedervi sconfitti, perché è falsa. Gli uccelli del malaugurio non piacciono agli italiani, soprattutto quando toppano sistematicamente tutte le loro previsioni, men che meno hanno successo tra gli italiani ogniqualvolta si va alle elezioni.

non è e non potrà essere più solo una somma o un insieme di regole, così come spesso viene percepita. L'Europa è una comunità di popoli, è Ha parlato esattamente quanto gli altri; anche il senatore Boccia ha avuto un prolungamento del suo tempo.

non ha fatto ridere molto, non l'abbiamo capita! *(Ilarità).* Ricordo che il ministro per gli affari europei, onorevole Fitto, ha espresso i seguenti pareri: ha accettato

il Governo ha espresso parere contrario sulle premesse e parere favorevole sugli impegni 1, 2, 3 e, previa riformulazione, anche sul 5, nonché favorevole sul 6 e 7 e, previa riformulazione, anche sull'8.

Anche se non ci sono contestazioni in proposito, voglio comunque dare lettura della valutazione regolamentare: ai sensi del combinato disposto degli articoli 102, comma 5, e 105 del Regolamento, sulla base dei pareri formulati dal Governo e delle richieste pervenute alla Presidenza, invito l'Assemblea a esprimersi intanto per alzata di mano sulle proposte di votazione per parti separate, per ciascuna risoluzione, del complesso dei punti con parere favorevole del Governo e, successivamente, del complesso dei punti sui quali è stato espresso parere contrario. Ove non diversamente indicato - attenzione! - riterrò accolte dai proponenti le richieste di riformulazione da parte da parte del Governo, prima enunciate, finalizzate all'espressione del parere favorevole. Non si procederà alla votazione per parti separate per le risoluzioni sulle quali il parere del Governo è unitariamente favorevole o contrario.